Comunico che, in data 16 luglio 2020, è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la pubblica amministrazione*: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»

penso che sia già in distribuzione. Ci troviamo in un contesto di crisi finanziaria senza precedenti e da mesi il Governo sta approntando tutte le contromisure per reggere l'urto di questo 2020 all'insegna del coronavirus. Ovviamente gli istituti di credito in questa fase si trovano costretti ad alzare i livelli di attenzione per limitare i rischi di insolvenza, l'accesso ai finanziamenti è divenuto sempre più difficile anche per società di grandi dimensioni. Tra esse, c'è il segmento pesantissimo delle grandi aziende che lavorano nel contesto del trasporto aereo. Le compagnie più importanti, infatti, da sempre sfruttano forme di finanziamento particolari per imbastire le loro flotte e per l'acquisizione di aeromobili spesso si fa leva su contratti di *leasing* o finanziamenti specifici. Tra questi, quelli su scala internazionale diventano sempre più competitivi, purtroppo però le nostre imprese spesso si trovano impossibilitate ad accedervi a causa dell'inadeguatezza e della farraginosità del nostro sistema giuridico. La lentezza della giustizia italiana, gli strumenti di garanzia previsti dal nostro ordinamento hanno determinato un progressivo allontanamento da parte dei finanziatori di aeromobili dal nostro Paese, dato che non consentono al finanziatore di poter rapidamente riprendere possesso dell'aeromobile, mettendo in difficoltà le compagnie aeree italiane nell'accesso ai più vantaggiosi sistemi di In questa fase di crisi finanziaria globale, il *gap* che rischiano di dover affrontare le nostre aziende dell'aerotrasporto rischia di diventare insormontabile. In verità, la questione è sul tavolo della politica già da circa vent'anni. Per ovviare al problema, nel 2001 l'Italia ha firmato la convenzione di Cape Town, relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e con essa il protocollo relativo alle garanzie internazionali su beni mobili per le questioni inerenti al materiale aeronautico. Sia la convenzione che i protocolli, all'epoca, dovevano avere la finalità di offrire un quadro normativo omogeneo per la registrazione delle proprietà, degli interessi

di finanziamento dei beni aeronautici, aeromobili o parti di essi, attraverso la creazione di una garanzia internazionale particolarmente forte a favore dei creditori (venditori a credito, organismi finanziari che hanno finanziato tali beni) che accorda loro la prelazione assoluta su tali beni in un registro internazionale. La convenzione è entrata in vigore il 1° marzo 2006 ed è stata firmata da ben 81 Paesi, mentre il protocollo riguardante gli aspetti inerenti al materiale aeronautico è entrato in vigore il 1° marzo 2008 ed è stato ratificato inizialmente da 8 Paesi, ai quali se ne sono successivamente aggiunti altri, per un totale di 65 Paesi. Nel 2009 è stato ultimato l'*iter* di adesione dell'Unione dell'Unione europea. L'Italia, pur essendo una firmataria della prima ora sia della convenzione, sia del protocollo, non ha mai proceduto alla ratifica della convenzione. Ciò ha portato gli operatori del settore a individuare strumenti contrattuali *ad hoc* per disporre degli aeromobili senza quasi mai procedere col loro acquisto. Ciò spiega perché oggi non ci sono aeromobili registrati in Italia presso ENAC, dato che la gran parte risultano registrati all'estero nei Paesi che hanno ratificato la convenzione. Il recepimento della convenzione di Cape Town nel nostro sistema giuridico consentirà, appunto, agli operatori di ridurre i rischi finanziari attraverso l'introduzione di criteri efficienti ed armonizzati a livello internazionale per la tutela delle banche finanziatrici o delle società di *leasing*, come per esempio il diritto di rivendicare la proprietà del velivolo o il diritto del creditore ipotecario di accedere al bene ipotecato. Nella pratica, la convenzione prevede che, al momento di acquistare un aereo, i vettori di uno Stato aderente al relativo protocollo possano ottenere dai fornitori condizioni finanziarie notevolmente migliori di quelle normalmente applicate dal mercato. fronte di tali vantaggi per il vettore, il creditore in caso di insolvenza o fallimento del cliente potrà facilmente recuperare quanto a lui dovuto, in virtù dei rimedi previsti dalla convenzione e dall'annesso protocollo. Proprio grazie ai predetti rimedi e alla conseguente possibilità di ripossesso immediato del bene aeronautico che la convenzione e l'annesso protocollo riconoscono al creditore

o al concedente in un contratto di *leasing*, i finanziatori hanno maggiori possibilità di assicurare, all'atto della conclusione del contratto, condizioni più flessibili e meno onerose. Il protocollo si applica solo e soltanto se il cosiddetto *obligor*, ovvero il soggetto passivo dell'operazione, cioè il vettore aereo, appartiene ad un Paese che ha ratificato l'accordo. Se sussiste questo presupposto, chi presta il finanziamento (*lessor*) si si affretta a iscrivere la transazione su un registro telematico internazionale situato nel Paese aderente alla convenzione e in quel momento diventa il creditore privilegiato di quell'aeromobile. Insomma, l'intero segmento non potrà che avere benefici abnormi: tutti i costruttori aeronautici nazionali, ad esempio, potranno beneficiare di un aumento delle vendite e dei livelli occupazionali grazie alle maggiori opportunità di finanziamento per i loro clienti con conseguenti vantaggi per i passeggeri, una riduzione del costo di finanziamento per le compagnie aeree avrà inevitabili riflessi sulle tariffe applicate ai passeggeri. Se sin qui la convenzione non è stata approvata, lo si deve principalmente al fatto che è caratterizzata da meccanismi che possono discostarsi dai tradizionali principi del nostro ordinamento in tema di garanzie a favore dei creditori che appaiono meno snelli di quelli dei Paesi di *common law*, su tutti quelli del sistema anglosassone. Proprio per superare tali ostacoli, la convenzione ha previsto un meccanismo di ratifica suscettibile di consentire agli ordinamenti di *civil law* come il nostro di potervi aderire con alcune riserve garantendo, al contempo, la massima diffusione della disciplina internazionale e l'armonizzazione delle regole nel settore del trasporto aereo. Con la ratifica, l'Italia potrebbe avanzare le dovute riserve a talune disposizioni della convenzione affinché essa, una volta ratificata, non si ponga in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento. Questo consentirebbe al nostro Paese di poter vedere le proprie flotte registrate in Italia, nel

la modifica delle norme del codice della navigazione. L'articolo 760 richiede, in caso di cancellazione dell'aeromobile dal RAN, un'attesa del velivolo in Italia di sessanta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione di tale richiesta, per consentire ad eventuali interessati di far valere le loro ragioni sullo stesso entro detto termine. Tuttavia, senza la ratifica sarà impossibile recepire i vantaggi previsti dalla convenzione in altra maniera nel nostro ordinamento. Nel mercato italiano, i finanziamenti di aeromobili, sia che si tratti di *leasing* finanziario o di *dry lease*, abbiano costi più alti, perché i vettori aerei operanti in Italia non possono accedere alla regolamentazione finanziaria relativa alle garanzie internazionali iscritte nel registro telematico, e laddove ciò avvenga sono costretti a registrare, per espressa richiesta del finanziatore (*lessor*), gli aeromobili in Paesi che hanno ratificato la convenzione e il protocollo anziché nel registro aeronautico nazionale il mancato recepimento da parte dell'Italia dell'articolo XI del protocollo sul materiale aeronautico rappresenta uno dei maggiori ostacoli che i *lessor* e le imprese costruttrici di aeromobili

all'avvio dell'*iter* di autorizzazione alla ratifica di cui al precedente impegno, a provvedere al conseguente riordino e adeguamento delle disposizioni contenute nel codice della navigazione in relazione alle procedure di registrazione e cancellazione degli aeromobili dal registro aeronautico nazionale, nonché alla normativa nazionale in materia d'insolvenza e di regime delle garanzie reali, oltre che delle pertinenti disposizioni processuali. Ha facoltà di parlare il senatore Mallegni - che invito cortesemente a recarsi al banco del relatore - per illustrare la mozione n. 270.

cercherò di essere meno formale e più improntato alla sostanza del provvedimento di cui stiamo discutendo. La questione è interessante e importante, perché, in particolare in questo momento in cui abbiamo di fronte un mercato dell'aviazione civile in grande difficoltà, mi parrebbe indispensabile addivenire alla sottoscrizione e alla ratifica di questa convenzione di Città del Capo.

fortunatamente si è aggiornata, perché, se ci limitassimo a offrire garanzie e tutele per l'acquisto di aeromobili, oggi saremmo fuori dal mondo.

però che rinuncio all'intervento, onde non creare disagio ai colleghi che si stanno facendo gli affari loro - correttamente - e di conseguenza vorrei che continuassero. Quindi, io mi asterrei dal proseguire l'intervento e spero che voterete la mozione che Forza Italia ha presentato.

Mi permetterà la Presidenza di divagare leggermente per soffermarmi sul concetto di solidità economica dal punto di vista imprenditoriale e non necessariamente con il sostegno pubblico. riteniamo necessaria la presenza dello Stato (ossia che il pubblico sia un elemento essenziale e importante della compagine societaria delle imprese, in particolare di quelle di bandiera), però ci siamo un po' fatti prendere la mano,

compagnia. La breve *liaison* con il concetto dell'internazionalità delle compagnie, la solidità e la sottoscrizione della convenzione mi impone di dire: attenzione, offriamo servizi e garanzie e obblighiamo a una solidità economica, però cerchiamo di fornire a chi opera nel mercato dell'aviazione (parlo delle imprese e dei privati) la possibilità di ottenere garanzie - queste sì

che carica sulle spalle dei cittadini - dal più piccino al più anziano - centinaia e centinaia di milioni di euro per finanziare

braccia aperte. La Ryanair arriva negli scali più strani del nostro Paese e raccoglie quattrini a piene mani:

che viene - anche giustamente - criticato nei confronti della compagnia di bandiera, viene erogato costantemente e mensilmente a compagnie private che hanno sede in Stati esteri, che non pagano le tasse nel nostro Paese e che portano via mercato al sistema dell'aviazione nazionale di Alitalia. Secondo uno studio di qualche giorno fa,

delle compagnie aeree che meritano, e non di quelle che speculano non lasciando nulla sul territorio nazionale.

delicato come quello della convenzione di Cape Town, una delle classiche convenzioni firmata dopo una conferenza a livello diplomatico per provare a uniformare normative diverse di Paesi diversi su questioni che implicano - come in questo caso - garanzie su beni mobili mobili anche di dimensione importante. Non a caso, il lavoro fatto dall'istituto per la salvaguardia e la difesa del diritto privato che si occupa di questi temi ha diviso in tre protocolli il suo lavoro: uno dedicato ai beni aeronautici, agli aeromobili; un altro legato al materiale rotabile, e un protocollo relativo ai beni spaziali. Le mozioni si indirizzano soprattutto sul protocollo in tema di beni aeronautici per una questione ben nota agli addetti ai lavori in Italia, quella concernente le garanzie internazionali sugli aeromobili; caso che riguarda da vicino anche le compagnie aeree italiane. La convenzione e i protocolli firmati dall'Italia non hanno mai avuto una ratifica, e ci sono delle motivazioni.

proprietà, interessi di sicurezza, locazioni e contratti condizionali di vendita, nonché diversi strumenti giuridici in caso di insolvenza per le convenzioni di finanziamento. Con la costituzione della garanzia internazionale, i finanziatori, attraverso l'iscrizione nel registro telematico internazionale, godono della possibilità di recuperare i beni aeronautici, ovvero gli aeromobili che, attraverso le loro organizzazioni, vengono dati in locazione. uno dei punti principali che riguarda anche il mercato italiano. L'Italia ha firmato la convenzione già da tempo, in particolare il protocollo concernente la parte aeronautica, nel dicembre 2001, ma non ha ratificato tali strumenti. Ciò comporta il rischio - in alcuni casi concreto,

alla regolamentazione finanziaria relativa alle garanzie internazionali iscritte nel registro aeronautico nazionale (RAN). Da questo punto di vista, le motivazioni per cui non si procede in questo senso sono dovute comprensibilmente che questa normativa ha subito l'influenza dei Paesi in cui vige un sistema giuridico caratterizzato dalla *common law* rispetto a realtà come la nostra caratterizzate dalla *civil law*. sia un tema sicuramente superabile per provare a costruire un contesto e un terreno per i nostri operatori tali da dare garanzia sia ai finanziatori che alle compagnie, anche perché è necessario uniformare e dare garanzie. L'Europa lo ha fatto solo parzialmente perché alcune riserve che si potevano mettere all'inizio,

opponibili. Da questo punto di vista, dobbiamo dare maggiori garanzie per poter uniformare il quadro normativo. una discussione e portare in Assemblea la ratifica. Quindi, vediamo di risolvere gli ultimi punti ancora in sospeso e di fare i necessari approfondimenti con tutti i Ministeri coinvolti, compreso il Ministero della giustizia, in modo da addivenire

adottare, all'interno del medesimo disegno di legge di ratifica, iniziative normative volte a innalzare le garanzie economiche necessarie a fondare una compagnia aerea in Italia e nella Comunità europea, prevedendo, tra l'altro, che una nuova compagnia aerea disponga di buona solidità finanziaria, da dimostrare anche, solo a titolo di esempio, tramite la proprietà di aerei; e al terzo punto che impegna ad attivarsi, per quanto di competenza e anche attraverso accordi internazionali, al fine di stabilire controlli efficaci sulle compagnie aeree che operano in Italia. È un tema

questi punti siano pleonastici e meritevoli di un approfondimento con altri strumenti. Da questo punto di vista, come ribadirà il senatore D'Arienzo

le mozioni al nostro esame intendono sollecitare il recepimento del trattato multilaterale di Città del Capo attraverso il quale si vuole creare un complesso di norme omogenee, di *standard* e di garanzie internazionali per quanto riguarda gli aeromobili e i motori, i beni mobili strumentali del settore aereo, ferroviario e spaziale. Una volta che tutti i Paesi che hanno sottoscritto il trattato lo avranno ricevuto nei rispettivi ordinamenti, esso avrà validità sui territori degli Stati aderenti. Il Trattato è importante specie in questo momento, perché riguarda uno dei settori - quello aereo - che più ha sofferto e soffre a causa delle chiusure agli ingressi e alle uscite dai vari Paesi nel mondo. Il Trattato intende dare una maggiore garanzia di stabilità finanziaria e, quindi, operativa al mercato di riferimento con - a caduta - garanzie per il settore del trasporto aereo e ferroviario e, pertanto, per gli ingressi degli stessi viaggiatori. La Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e i tre protocolli riguardanti il materiale aeronautico, il materiale rotabile ferroviario e i beni spaziali compongono il Trattato di cui chiediamo la ratifica. La Convenzione è del 2004 ed è già stata firmata da ventotto Paesi; il Protocollo sul materiale aeronautico invece è del 2006 e hanno già aderito quarantasei Lo scopo del pacchetto di disposizioni cui chiediamo di aderire, recependole con una legge italiana, è offrire un quadro normativo che semplifichi l'offerta di finanziamento di beni aeronautici mediante una garanzia internazionale. In assenza delle nuove disposizioni a garanzia, abbiamo un mercato italiano dove i finanziamenti di aeromobili hanno costi più alti, in quanto né i finanziatori, né i debitori possono accedere alla regolamentazione finanziaria relativa alle garanzie internazionali iscritte nel registro telematico internazionale. Il Trattato, al contrario, contiene diverse tipologie di garanzia sia per i finanziatori che per i debitori. Quella che riteniamo sia la più interessante per il settore dei nostri aeromobili ed elicotteri è la cosiddetta disciplina di efficacia e opponibilità ai terzi della garanzia iscritta nel registro internazionale ed anche la possibilità di applicare la Convenzione stessa e i mezzi immatricolati nel registro degli aeromobili di uno Stato contraente. Allo stesso modo, in caso di insolvenza del creditore, le procedure di restituzione del materiale aeronautico possono agevolare il settore in Italia. Il Trattato andrebbe quindi modificato e potenziato anche in funzione dei nostri interessi nazionali. Le compagnie aeree oggigiorno tendono ad utilizzare lo strumento della locazione finanziaria, il cosiddetto *leasing*, per i propri aeromobili e sempre meno a prenderli in proprietà. Pertanto, è persino possibile fondare una compagnia aerea avendo tutti gli aeromobili in *leasing*, condizioni molto semplificate che richiedono una capacità finanziaria certamente ridotta. Questo può essere anche visto come un elemento di criticità in un mercato, come quello dei servizi aerei, in cui si misurano grandi compagnie aeree fortemente strutturate. E per sfidare i colossi c'è il rischio che una società con una solidità finanziaria non adeguata sia poi costretta a chiudere dal confronto col mercato, con implicazioni evidenti sui posti di lavoro perduti, sul mancato versamento dei contributi, sull'attivazione degli strumenti pubblici di sostegno al reddito, sui fornitori e sui creditori, ma rilevando possibili ricadute negative anche sui passeggeri. Quindi, siamo certamente favorevoli a ratificare la Convenzione di Città del Capo e il relativo Protocollo in materia di materiale aeronautico attraverso gli opportuni strumenti di legge. Allo stesso tempo siamo a favore dell'innalzamento delle garanzie economiche necessarie a fondare una compagnia aerea in Italia e nell'Unione europea: disposizioni che si potrebbero inserire nella stessa legge di ratifica. Mai come in questo momento bisogna operare una distinzione netta tra operatori affidabili e meno affidabili, per cui diventano importanti le funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile per la verifica degli *standard* stabiliti - noi diciamo - a presidio della solidità delle compagnie aeree, ma intendiamo soprattutto a garanzia di chi viaggia in aereo e dei cittadini, su cui spesso ricade il conto del fallimento delle compagnie aeree.

ovvero «a favorire, in tempi rapidi, l'avvio dell'*iter* per la presentazione alle Camere del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della convenzione di Cape Town Per quanto riguarda i punti 2, 3 e 4 del dispositivo, esprimiamo parere contrario, perché si tratta di aspetti non attinenti alla Convenzione di Cape Town e che, per la loro rilevanza, meritano un approfondimento separato.

in particolar modo nel settore aeronautico, dove gli acquisti sono finanziati dalle aviolinee attraverso operazioni molto complesse e contratti di *leasing* che richiedono un sistema di diritti e garanzie a favore della banca finanziatrice o della società di *leasing*, diventa sempre più gravoso, anche a causa della lentezza dei vari processi e a volte dei vuoti normativi del nostro sistema giuridico, accedere a finanziamenti internazionali più competitivi, allontanando così un numero elevato di finanziatori di aerei. Per superare le suddette difficoltà, nel 2001 l'Italia ha firmato il Trattato internazionale nella conferenza diplomatica di Città del Capo, ma ad oggi la Convenzione e il relativo Protocollo aeronautico attendono di essere ratificati. Recependo finalmente la Convenzione nel nostro sistema giuridico potremo ridurre i rischi finanziari mediante l'introduzione di criteri unici per la tutela della banca finanziatrice o della società di *leasing*, come ad esempio l'introduzione di norme internazionali comuni per individuare la giurisdizione competente per la risoluzione dei conflitti, oppure il diritto di rivendicare la proprietà del velivolo o il diritto del creditore ipotecario di accedere al bene ipotecato. Finalmente i finanziatori, attraverso l'iscrizione nel registro internazionale unico completamente accessibile *online*, in cui si iscrivono i velivoli, il proprietario e le garanzie date alle banche su base dichiarativa e seguendo il principio della antecedenza, avranno una prelazione assoluta rispetto alle iscrizioni successive. Con la ratifica della Convenzione, i creditori potrebbero servirsi di una serie di misure finalizzate a far valere i propri diritti o interessi sull'aeromobile, incluse le operazioni per rendere più rapida possibile l'assunzione di provvedimenti cautelari senza la necessità di intervento giudiziario. Si avrebbe la garanzia di soddisfazione a livello generale dei requisiti specifici del settore aeronautico concedendo la massima fiducia a finanziatori e creditori impegnati nel garantire il credito nel settore.

internazionali con benefici generalizzati e diffusi. È importante e necessario avere un quadro giuridico unico di riferimento per le garanzie internazionali sui velivoli per rispondere correttamente alle esigenze ormai internazionalmente riconosciute e permettere a tutte le parti interessate al settore del trasporto aereo di godere di ampi e reciproci benefici. Ratificare la Convenzione significherebbe equiparare la nostra legislazione a quella di altri Paesi per attrarre banche e società di *leasing* aeronautico, le quali sicuramente preferiscono registrare i propri velivoli in Paesi coperti dalla Convenzione. Si incrementerebbe così l'operatività delle aviazioni civili nazionali e la competitività delle banche nazionali attraverso la riduzione di costi e rischi per i finanziamenti internazionali. Avremo anche la possibilità di sviluppare un contesto politico e legislativo favorevole per le società di *leasing* e le banche finanziatrici, con un rilevante incremento dell'occupazione e maggiori introiti fiscali. La ratifica in esame appare dunque necessaria per portare ossigeno alle aviolinee con una certa riduzione dei costi finanziari e un più ampio accesso alle fonti di finanziamento internazionali. Ancora, è fuor di dubbio che con la Convenzione ratificata tutti i costruttori aeronautici nazionali, grazie alle maggiori opportunità di finanziamento per i loro clienti con conseguenti vantaggi anche per i passeggeri, in quanto una riduzione del costo di finanziamento necessariamente influirà sulle tariffe aeree, potranno così aumentare non solo le vendite, ma - quello che è più rilevante - anche i livelli occupazionali con beneficio economico e sociale per tutto il nostro Paese. Per tutti questi motivi, il Gruppo parlamentare Italia Viva-P.S.I. condivide la mozione e dichiara il proprio voto favorevole.

perché in un momento delicato come l'attuale, con le banche di tutto il mondo, comprese quelle italiane ovviamente, che sono in sofferenza e hanno alzato l'attenzione sul tema del credito e dei rischi di insolvenza, l'accesso al credito è diventato punto essenziale per molte società, soprattutto quelle di grandi dimensioni. In riferimento agli aerei, che tradizionalmente si rifinanziano attraverso

di una serie di processi che limitano l'accesso delle aviolinee - sulle quali l'Italia ha delle esperienze molto significative - a finanziamenti internazionali più competitivi, rappresentano un problema per lo sviluppo in prospettiva delle società loro rifinanziamento richiede un sistema di diritti e di garanzie a favore della banca che finanzia o della società di *leasing* che nel nostro Paese sta comportando, a causa della presenza di una serie di ostacoli, situazioni addirittura paradossali. Per superare tali difficoltà si era pensato al Trattato che è stato firmato nel 2001 e che poi

delle banche o delle società di *leasing* - ad esempio - grazie al diritto di rivendicare la proprietà del veicolo o del creditore ipotecario di accedere al bene ipotecato, che sembrano due banalità assolute ma, ad oggi, l'attuazione dei principi previsti dalla Convenzione di Cape Town permetterà di semplificare e armonizzare le procedure internazionali garantirà benefici generalizzati e diffusi in particolare al nostro Paese. La creazione, finalmente, di un quadro giuridico di riferimento unico per le garanzie internazionali sui veicoli risponde ad esigenze riconosciute

il Trattato di Cape Town e questo ha creato un disequilibrio anche all'interno della stessa Unione europea, nell'ambito della quale alcuni Paesi come l'Irlanda fanno da padroni. sua ratifica da parte nostra ci permetterebbe di equiparare la nostra legislazione a quella degli altri Paesi che attraggono le aviolinee per i finanziamenti delle banche o delle società di *leasing* aeronautico. È più conveniente infatti registrare i propri velivoli - lo fa anche all'Italia - in questi Paesi, incrementando l'operatività delle operazioni altrove, anche se si tratta di beni nazionali. Dunque, l'approvazione della Convenzione aumenterebbe la competitività delle nostre banche e delle nostre società di *leasing* e ciò potrebbe comportare, ovviamente, una riduzione dei costi per le società aeree e rischi minori connessi ai finanziamenti internazionali. La ratifica del Trattato di Cape Town porta,

da parte dell'Italia, del Trattato di Cape Town permette di ridurre il rischio - finora è capitato e capiterà ancora - che si sono assunte le agenzie Sace e Simest nell'attività di finanziamento delle esportazioni italiane. Infatti, sia Sace che Simest sono particolarmente impegnate in questo momento e presenti sul finanziamento delle esportazioni di alcuni velivoli. In prospettiva, la ratifica del Trattato porterà l'Italia allo stesso livello di altri Paesi nel mondo ma, soprattutto, all'interno dell'Unione Europea; e potrebbe favorire i costruttori aeronautici nazionali, che potranno beneficiare, potenzialmente, di un aumento sia delle vendite che dei livelli occupazionali, grazie alle maggiori opportunità di finanziamento per i loro clienti. Questo potrebbe determinare anche una riduzione dei costi dei riflessi positivi sulle tariffe aeree. Quindi, la ratifica della Convenzione - così come diceva anche il collega, senatore Alfieri, che si è espresso nella fase della

Per chiudere questo processo, che va avanti da molti anni, si è dovuto attendere la riflessione, alla fine conclusa, finalmente, da parte dell'Unione europea, su chi avesse la titolarità a ratificare questo Trattato: se i Parlamenti nazionali o l'Unione europea stessa (la Commissione europea, nel particolare). Adesso che il nodo è stato sciolto, ovvero che spetta

benefici sia sui flussi di finanziamento sia sulla salvaguardia del nostro patrimonio industriale e - ci auguriamo - anche sulle tariffe per i passeggeri. Per queste ragioni positive, il Gruppo Partito Democratico sosterrà positivamente la mozione n. 133 (testo 2), a senatrice Lupo.

radente sulla nostra normativa. Negli anni Ottanta, in Italia, le compagnie aeree che volevano aprire ed effettuare l'attività di trasporto passeggeri e il trasporto merci, dovevano avere la disponibilità, all'interno della propria flotta, di oltre il 50 per cento di vettori in proprietà. Successivamente, la norma è cambiata e oggi ci ritroviamo con compagnie che aprono,

per poter aprire una compagnia aerea, con tutte le conseguenze del caso, a partire anche dai risparmi che molto spesso vengono effettuati nell'ambito della manutenzione e del controllo degli aeromobili.

Mi pare che ci troviamo anche qui di fronte a una situazione estremamente critica, proprio per l'insufficienza di garanzie; tant'è che negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a numerosi

di qualche concedente sia stato bloccato o pignorato. Questa è la situazione reale, che mette in grosse difficoltà i fornitori e tutta la conseguente catena e crea le situazioni di disequilibrio. Dobbiamo ancora segnalare all'interno della Comunità economica europea ci siano Paesi che hanno norme addirittura più elastiche rispetto

e mezzo di euro in tasse, in contributi INPS e in contributi al Fondo volo, che è il fondo

Secondo un rilevante studio uscito recentemente e pubblicato da un importante quotidiano nazionale, si è verificato che questione ottengono annualmente in Italia, dagli aeroporti italiani, circa 300 milioni di euro. è un fatto notorio - le tasse non vengono pagate in Italia e questo è un problema. La maggior parte dei passeggeri che proviene dall'Italia viene trasportata al di fuori dell'Italia stessa. Qui vorrei ricordare la situazione della British Airways, che è una grande compagnia aerea, avente un numero molto elevato di vettori internazionali; le compagnie *low cost* in buona sostanza si trovano ad aiutarla e ad incrementarne l'attività, mentre Alitalia si trova in difficoltà, soprattutto per la ragione che evidenziavo prima, e cioè la concorrenza sleale. In conclusione, riteniamo assolutamente

da poter effettuare i controlli adeguati su tutte le compagnie aeree operanti in Italia, in particolare su quelle nazionali che dovessero rivelarsi eccessivamente elastiche nell'applicazione delle norme. Infatti le Nazioni, che molto spesso - come detto all'inizio del mio intervento - hanno una legislazione a maglie molto larghe, si mettono in concorrenza con le nostre compagnie di navigazione, in particolare con Alitalia.

possa essere di grande interesse e soprattutto consentire all'Italia di mettersi sui binari giusti per poter recuperare economicamente quella forbice creatasi con le compagnie aeree di altri Paesi, che sono molto più strutturati rispetto al nostro.

per fare ciò. La procedura è ovviamente legittima, ma noi abbiamo preferito non depositare una mozione perché crediamo esistano delle vie molto più brevi per fare un'operazione

Qualcuno ha citato prima le compagnie *low cost*. Il mondo dei trasporti aerei, anche se non sono un esperto, è profondamente cambiato, come è cambiato anche il mondo dell'aerospazio. Quindi oggi non esistono più i grandi vettori, ma si parla di

l'oggetto del contendere è sicuramente estremamente importante, soprattutto in questo periodo. Veniamo da una crisi enorme, che non conosce pari da molti decenni, ed è chiaro che anche il settore in questione ha bisogno di una

permetterebbe di avere un quadro normativo omogeneo e, quindi, uno scenario giurisdizionale unico, che ovviamente è importante per la possibilità di attrarre investimenti per le nostre aziende, per le nostre aziende, ma anche, in maniera bidirezionale, per permettere ai nostri imprenditori di muoversi liberamente sul mercato internazionale. La mancata ratifica della Convenzione da circa vent'anni ha determinato il fatto che sul mercato italiano ovviamente abbiamo avuto, purtroppo, dei costi molto più alti e tutto ciò ha aumentato il rischio del settore sul mercato finanziario. È già stato detto che ci sarà una forte riduzione dei rischi finanziari per strutture

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, la mozione che ci apprestiamo a votare oggi riveste grandissima importanza, affinché il Governo possa dare seguito a quanto stabilito nel Trattato nel Trattato multilaterale adottato nel corso della conferenza diplomatica tenutasi a Città del Capo tra il 29 ottobre e il 16 novembre del 2001; un Trattato dai contenuti specifici di grande peso. Parliamo di garanzie internazionali su beni mobili strumentali, ovvero di norme uniformi che disciplinano la costituzione e gli effetti di una garanzia internazionale su determinate categorie di beni mobili strumentali. Il nuovo quadro giuridico internazionale mira - come indicato in una relazione della Commissione europea - a facilitare l'offerta di finanziamento dei beni aeronautici attraverso la creazione di una garanzia internazionale particolarmente forte a favore dei creditori, che accorda loro la prelazione

ma il cosiddetto Protocollo, quello che specificatamente tratta di aeromobili e motori aeronautici, entra in vigore solo dopo due anni, il 1° marzo 2006. A quella data era stato ratificato da otto Paesi (Etiopia, Irlanda, Malesia, Nigeria, Oman, Panama, Pakistan e Stati Uniti), ai quali poi si sono aggiunti successivamente altri Stati. Purtroppo l'Italia non ha ratificato né la Convenzione né il Protocollo aeronautico, pur avendo firmato entrambi i documenti in data 6 dicembre 2001. Questo, signor Presidente, ci è costato molto in termini economici, in quanto nel mercato italiano i finanziamenti ad aeromobili hanno costi elevati; i vettori aerei operanti in Italia non possono infatti accedere alla regolamentazione finanziaria relativa alle garanzie internazionali iscritte nel registro telematico e naturalmente ciò condiziona l'intero mercato. Come l'Italia, anche la Francia e la Germania hanno firmato la Convenzione e il Protocollo, rispettivamente nel 2001 e nel 2002, ma non hanno ancora provveduto a ratificarli. All'inerzia delle istituzioni italiane ha risposto la Commissione europea, presentando inizialmente due proposte di firma poi bloccate in seno al Comitato speciale dei rappresentanti permanenti, a causa di dissidi tra Spagna e Regno Unito. Nel frattempo, a partire dal 2004, nuovi Stati hanno aderito all'Unione europea e il 1° marzo 2006 la Convenzione di Cape Town e il Protocollo sul materiale aeronautico sono entrati in vigore, rendendo del tutto obsoleta la proposta di firma avanzata dalla Commissione europea e rendendo altresì necessario l'avvio di un procedimento Il procedimento di adesione da parte dell'Unione europea si è concluso il 29 aprile 2009 e la Convenzione e il Protocollo sono entrati in vigore nell'ordinamento europeo il successivo 1° agosto. Nonostante tale adesione, le limitazioni restano diverse. La disciplina soprarichiamata relativa alla garanzia internazionale sui beni strumentali e la prelazione garantita al finanziatore che provvede all'iscrizione di tale garanzia nel registro telematico non è ancora applicabile. È giunto il momento di ovviare a queste condizioni che risultano controproducenti per il nostro Paese. La citata Convenzione e il Protocollo aeronautico introducono un nuovo quadro giuridico relativo alle garanzie internazionali sui beni strumentali, sui relativi diritti e alla definizione in tale ambito La Convenzione specifica il campo di applicazione dello strumento finanziario; favorisce le debite definizioni; fissa i prerequisiti formali per la costituzione di garanzia internazionale, disciplinando la loro efficacia nei confronti di terzi e stabilisce i mezzi di ricorso giudiziali in caso di inadempienze alle previsioni della stessa. Secondo la Convenzione di Cape Town, i vettori di uno Stato aderente al relativo protocollo che acquistano un aereo possono giungere con i loro fornitori a condizioni finanziarie nettamente migliori rispetto a quelle normalmente applicate dal mercato. Insomma, è una svolta decisiva. A fronte di tali vantaggi per il vettore, il creditore, in caso di insolvenza o fallimento del cliente, potrà facilmente recuperare quanto a lui dovuto in virtù di rimedi previsti dalla Convenzione e dall'annesso Protocollo: un aspetto anche questo che va preso in massima considerazione. Più in particolare il Protocollo disciplina le modalità di restituzione a favore del finanziatore del materiale aeronautico che costituisce la garanzia del creditore per il caso di insolvenza del debitore. Tra le misure di maggior rilievo va menzionata la possibilità del creditore di ottenere, in caso di inadempimento e purché siano presenti determinate condizioni, la cancellazione dell'aeromobile dal registro nazionale di immatricolazione o l'esportazione e il trasferimento fisico del materiale aeronautico dal territorio nel quale esso si trova. Appare del tutto evidente che un vettore che impiega aeromobili registrati in un Paese aderente alla Convenzione, sia in forma di *leasing* sia nel caso di proprietà da parte di una propria una propria controllata, può sfruttare l'adesione del proprio Paese al Protocollo, ottenendo delle migliori condizioni. A fronte di ciò, c'è la garanzia in capo a chi eroga il finanziamento di avere maggiori certezze, che gli permettano di rivalersi immediatamente, qualora ciò si renda necessario. Tra gli Stati a noi geograficamente più vicini, alla Convenzione e al Protocollo hanno aderito la Repubblica di Malta e la Repubblica di San Marino,

Cape Town del 2001, in quanto tale recepimento servirebbe ad uniformare, a vantaggio tanto del creditore quanto del debitore, la disciplina della registrazione della proprietà, del finanziamento e delle garanzie relative alle transizioni internazionali aventi ad oggetto specifici beni, come gli aeromobili, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

Signor Presidente, da ligure è un onore illustrare la mozione presentata dal mio Gruppo sulla gestione delle autostrade, sul blocco della rete autostradale che la mia Regione subisce quotidianamente, con ingenti danni economici, e sui dubbi che riguardano l'accordo siglato nel Consiglio dei ministri in data 15 luglio I dubbi sull'accordo riguardano principalmente l'uscita di scena di Atlantia e il subentro di Cassa depositi e prestiti. Siamo preoccupati per il debito di Aspi, che si aggira intorno ai 10 miliardi di euro, cui dovrà far fronte chi subentra ad Atlantia, cioè Cassa depositi e prestiti. Ricordiamo che Cassa depositi e prestiti si finanzia principalmente con il risparmio postale degli italiani, quindi, a meno di chiarimenti, ad Atlantia andranno gli utili e agli italiani i debiti.

«Premesso che la società Autostrade per l'Italia SpA gestisce 2.857 chilometri di rete autostradale in Italia sulla base della Convenzione unica sottoscritta in data 12 ottobre 2007 con l'allora ente concedente ANAS SpA; nella rete autostradale gestita da Autostrade per l'Italia SpA rientra il tratto autostradale della A10 Genova - Savona, su cui insiste il viadotto Polcevera (anche noto come ponte Morandi), crollato il 14 agosto 2018, con la conseguente morte di 43 persone; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sua qualità di autorità amministrativa concedente, ha avviato un procedimento volto ad accertare eventuali inadempimenti del concessionario Autostrade per l'Italia SpA agli obblighi scaturenti dal rapporto concessorio in essere; contestualmente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha avviato le indagini volte a individuare eventuali profili di responsabilità penale connessi al crollo del ponte e ai decessi da esso cagionati; la Convenzione unica del 2007 disciplina, *inter alia*, l'accertamento di gravi inadempimenti del concessionario, la decadenza della concessione e le ipotesi di recesso, revoca e risoluzione della Convenzione; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto n. 386 del 2018, ha nominato una commissione ispettiva, la quale ha elaborato una relazione tecnica, sulla base della quale il Ministero ha prospettato alla società concessionaria la risoluzione della Convenzione per grave inadempimento agli obblighi assunti, in relazione a quanto peraltro previsto dalle citate disposizioni della Convenzione unica del 2007; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto n. 119 del 2019, ha altresì istituito un gruppo di lavoro chiamato a verificare le possibili implicazioni giuridiche delle condotte o delle omissioni della società Autostrade per l'Italia SpA, con riferimento al perimento del viadotto Polcevera; tale gruppo ha concluso i suoi lavori con l'approvazione della relazione in data 28 giugno 2019; l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, dispone il subentro di ANAS SpA nella gestione di strade o autostrade in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione delle relative concessioni, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario»...

giusto nei confronti di chi invece vuole ascoltare. *(Commenti)*. Avete poco da recriminare: chi non vuole ascoltare, può benissimo uscire. *(Applausi)*. Ho il diritto di illustrare una mozione che interessa un'intera Regione che in questo momento è al collasso. «Nel corso della seduta n. 56, tenutasi nella notte tra il 14 e il 15 luglio 2020, il Consiglio dei ministri ha deliberato di definire la controversia con Autostrade per l'Italia SpA accettando le proposte transattive presentate da quest'ultima; tali proposte prevedono in sintesi: un nuovo assetto societario della stessa Autostrade per l'Italia SpA, con l'immediato passaggio del controllo di essa ad un soggetto a partecipazione statale individuato in Cassa depositi e prestiti (CDP), nonché l'uscita di Autostrade per l'Italia dal perimetro dell'attuale controllante (Atlantia) e la sua contestuale quotazione in borsa; la realizzazione di investimenti compensativi da parte di Autostrade per l'Italia per 3,4 miliardi di euro, la riscrittura della Convenzione unica, il rafforzamento del sistema dei controlli a carico del concessionario, l'adeguamento alla disciplina tariffaria introdotta dall'Autorità di regolazione dei trasporti e l'inasprimento delle sanzioni per violazioni da parte del concessionario. Considerato che: a quasi due danni dal crollo del Ponte Morandi, non si è giunti ad alcuna decisione in ordine alla revoca o mantenimento in essere della concessione autostradale in capo alla società Autostrade per l'Italia SpA; in meno di due anni si è provveduto alla costruzione del nuovo viadotto, che sarà inaugurato nelle prossime settimane, grazie allo speciale regime normativo previsto dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109; la perdurante situazione di stallo tra Governo e la società Autostrade per l'Italia SpA ha portato al blocco di tutti gli investimenti privati sulla rete autostradale in concessione per 14,5 miliardi di euro, nonché ad una totale paralisi della viabilità ligure: da molte settimane, infatti, l'Autostrada dei Fiori (A10) e l'Autostrada dei Trafori (A26) sono interessate da ispezioni e lavori di manutenzione dei viadotti e delle gallerie, il perdurare dei quali è causa di code e rallentamenti su tutta la rete viaria ligure, con pesanti disagi per i cittadini e imprese e perdite per oltre 1 miliardo di euro al mese per il sistema logistico nazionale; i disagi sulla viabilità della Liguria si sono riverberati sul volume dei traffici del porto di Genova e Savona, con un crollo pari a circa il 30 per cento negli ultimi due mesi, impegna il Governo: ad attivarsi affinché la società Autostrade per l'Italia SpA realizzi idonei investimenti sulla rete autostradale in concessione a seguito del crollo del Ponte Morandi, e realizzi in particolare gli interventi infrastrutturali richiesti dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova per il territorio e il sistema portuale liguri; a garantire l'effettiva realizzazione degli investimenti compensativi da parte di Autostrade per l'Italia SpA in tempi certi, quale precondizione essenziale alla conclusione dell'accordo transattivo citato in premessa; ad addivenire ad una risoluzione della controversia insorta con Autostrade per l'Italia SpA priva di oneri per lo Stato; a provvedere alla tutela di tutti i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti, siano essi gli azionisti, i creditori, i fornitori e i 6.923 dipendenti di Autostrade per l'Italia SpA, nonché al pagamento di indennizzi dovuti alle imprese a compensazione dei danni economici eventualmente patiti; a provvedere, nel caso di assunzione del controllo di Autostrade per l'Italia SpA da parte di Cassa depositi e prestiti, alla tutela degli investitori istituzionali e di tutti i soggetti il cui risparmio gestito costituisce la maggiore fonte di finanziamento di CDP; a riformare a riformare la normativa vigente in materia di concessioni autostradali, nei termini di semplificazione e chiarezza normativa, prendendo a riferimento, per quanto compatibili, le *best practice* riferibili ad altri regimi concessori». Ho concluso, Presidente.

in dichiarazione di voto in maniera più generale sull'argomento che si presta a molte riflessioni, anche di ordine politico, come è facilmente intuibile. La nostra mozione, in realtà, riprende un argomento che avevamo già sviluppato quasi quasi un anno fa, quando era esplosa la questione del Ponte Morandi nonché la questione della desecretazione del regime di concessionario, e cioè degli accordi tra lo Stato e le società private che avevano preso in gestione la rete autostradale. Emergeva una stranezza che, peraltro, era facilmente riscontrabile da parte di chiunque frequentasse o frequenti come utente la rete autostradale. Mi riferisco alla lievitazione abnorme e ingiustificata dei costi

perché ci sono delle *royalties* che lo Stato ha autorizzato da parte della società private nei confronti dei gestori di questi servizi commerciali. Si tratta di un regime assolutamente illiberale, ingiustificato e totalmente monopolistico, naturalmente sulle attività commerciali che sono costrette a imporre prezzi che le escludono dal mercato e dalla competizione. All'interno del mercato libero italiano, pertanto, c'è una sorta di regime costruito

cento. Non siamo dinanzi a un regime concessionario, ma a una cuccagna che lo Stato ha autorizzato nei confronti di privati. Accanto alla cuccagna di Stato, che si alimenta di pedaggi che aumentano ogni anno molto più dell'inflazione senza gli investimenti che dovrebbero essere associati; accanto alla strozzatura delle attività commerciali e di un regime totalmente illiberale e accanto al fatto che questi poveri

Il regine autostradale non può essere in contrasto con le leggi italiani e le altre attività che si svolgono al di fuori della rete autostradale. La conclusione che il Governo ha annunciato su questa vicenda, di cui parlerà il collega Fazzolari fra qualche minuto, è una soluzione che non ci convince. Presidente, circa tre giorni, prima della conclusione, il *premier* Conte su esplicitato in maniera solenne due concetti: lo Stato non sarà mai socio di Benetton e la revoca è la strada maestra. La revoca non c'è stata; non c'è stata la risoluzione del contratto; i Benetton sono ancora soci dello Stato. I Benetton ci sono, mentre la revoca non c'è. Se i Benetton usciranno da autostrade, lo faranno con il portafoglio gonfio in tempi che nessuno è ancora in grado di determinare, ma che si annunciano

Un accordo è un atto scritto; ci saranno un documento e un piano industriale; ci sarà un accordo scritto tra le parti: ci vuole un atto ufficiale sottoposto al controllo del Parlamento e su cui il Parlamento possa esprimere un proprio parere. Noi ad oggi - lo chiedo anche al rappresentante del Governo - non abbiamo un pezzo di carta dal quale dedurre i tempi e i modi di questo passaggio da Benetton a Cassa depositi e prestiti e per la realizzazione - per quanto abbiamo potuto capire perché, ripeto, non abbiamo pezzi di carta e dati ufficiali - di una *public company*, di cui lo Stato dovrebbe essere indirettamente il controllore.

costino molto di più di quanto il mercato chiede e molto di più di quanto anche il buonsenso possa immaginare. Questo è un regime che non può continuare; lo Stato deve intervenire perché alla fine chi paga il prezzo di tutto questo è ancora una volta l'utente dell'autostrada, che deve far fronte a un servizio indispensabile gestito in maniera monopolistica, ma i monopoli, anche di Stato, devono essere vietati.

Prima di illustrare la mozione vorrei fare un breve passaggio preliminare: oggi infatti ci troviamo in quest'Aula a trattare il tema autostrade perché il Governo e la maggioranza hanno sicuramente messo a segno un punto importante. C'era chi dava per giuridicamente impossibile o tecnicamente sbagliata la risoluzione del contratto di concessione avanzata all'indomani degli approfondimenti tecnici che hanno riguardato i fatti tragici verificatisi con il crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018. Oggi invece possiamo affermare chiaramente che la parte privata evidentemente non la riteneva così impossibile, altrimenti non avrebbe accettato di arrivare ad una transazione con lo Stato che ribalta il modello di gestione delle autostrade sin qui seguito. Venendo nel merito della discussione, ripercorro velocemente quanto accaduto dall'agosto del 2018 fino ad arrivare al grande risultato ottenuto oggi. È noto a tutti che, all'indomani del crollo del viadotto Polcevera insistente sul tratto autostradale della A10 Genova-Savona, il Ministero delle infrastrutture ha avviato verifiche per accertare eventuali inadempimenti degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio in essere in forza della convenzione unica del 2007 da parte di Autostrade per l'Italia. È stata nominata successivamente una commissione ispettiva tecnica, a cui è stato chiesto di individuare le possibili cause del crollo del viadotto. La commissione, il 14 settembre 2018, ha ultimato le attività depositando una relazione tecnica. La Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali del medesimo Ministero, con nota del 16 agosto 2018, ha formalmente avviato nei confronti della concessionaria la contestazione di gravissimo inadempimento degli obblighi di manutenzione e custodia in oggettiva considerazione del collasso dell'infrastruttura, delle vittime accertate e degli ingenti danni riportati ai beni anche di soggetti terzi. Quanto accaduto con il crollo del ponte Morandi ha avuto echi e riflessi sull'intera rete autostradale affidata in concessione, innanzitutto facendo venir meno la fiducia da parte del concedente, cioè lo Stato, che che rappresenta l'interesse generale di tutti nell'accordo con il concessionario privato, in particolare degli utenti di tutta la rete autostradale. In un tale contesto e vista la gravità dell'inadempimento della società concessionaria appariva pienamente plausibile l'opzione della risoluzione della convenzione e l'estinzione anticipata del rapporto concessionario con ASPI. Visti però gli elementi di complessità della questione, anche sotto il profilo giuridico, è stato successivamente istituito un gruppo di lavoro per procedere ad un approfondimento sull'ipotesi di soluzioni alternative alla risoluzione. È infatti doveroso ricordare che dalla prima convenzione del 1997, recentemente considerata illegittima dalla Corte dei conti, si sono succeduti ben venticinque anni di norme di favore per il concessionario e per il settore in generale, norme culminate con l'approvazione per legge dell'ultima convenzione avvenuta nel 2008 grazie all'allora governo di centrodestra, con dentro la Lega e l'attuale *leader* di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. È un fatto che venticinque anni di norme di favore, con l'avallo di una politica compiacente, potevano e potrebbero rendere molto insidioso un contenzioso con il concessionario, aggiungendo al dramma di quarantatré vite umane spezzate la potenziale beffa di una maxi-esborso a carico dello Stato. Si è giunti quindi, a seguito di attente e ponderate verifiche ed analisi, con il concerto tra tutte le amministrazioni interessate, alla soluzione individuata nel Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, durante il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha svolto un'informativa sullo stato di definizione delle procedure di grave inadempimento nei confronti di Autostrade per l'Italia SpA (ASPI). Nell'informativa sono state esposte le possibili alternative sulla definizione della vicenda. Durante la riunione sono state trasmesse da parte di ASPI due nuove proposte transattive riguardanti, rispettivamente, un nuovo assetto societario di ASPI e nuovi contenuti per la definizione transattiva della controversia. Va da sé che le proposte sono il frutto di un costante *pressing* che lo Stato è riuscito ad esercitare tenendo sempre ferma l'opzione della revoca. La proposta prevede specifici punti qualificanti riguardo al futuro assetto societario del concessionario, ovvero: misure compensative ad esclusivo carico di ASPI per il complessivo importo di 3,4 miliardi di euro; riscrittura delle clausole della convenzione al fine di adeguarle al decreto-legge n. 162 del 2019 (cosiddetto milleproroghe); rafforzamento del sistema dei controlli a carico del concessionario; aumento delle sanzioni anche in caso di lievi violazioni da parte del concessionario; rinuncia a tutti i giudizi promossi in relazione alle attività di ricostruzione del ponte Morandi, al sistema tariffario e all'accettazione della disciplina tariffaria introdotta dall'autorità di regolazione dei trasporti. In vista della realizzazione di un rilevante piano di manutenzione e investimenti, contenuto nella stessa proposta transattiva, Atlantia e ASPI si sono impegnate a garantire: l'immediato passaggio del controllo di ASPI ad un soggetto a partecipazione statale (Cassa depositi e prestiti); la cessione diretta di azioni ASPI a investitori istituzionali di gradimento di CDP; la scissione di Atlantia con l'uscita di ASPI dal perimetro di Atlantia e la contestuale quotazione di ASPI in Borsa. Il Consiglio dei ministri, a seguito di quanto emerso in seno al Consiglio medesimo, ha ritenuto di avviare l'*iter* previsto dalla legge per formale definizione della transazione. Il tempo trascorso dalla tragedia è servito ad arrivare alla migliore soluzione possibile, quella che maggiormente tutela l'interesse pubblico. Come ha detto il presidente del Consiglio Conte, ci interessa la sostanza e non gli *slogan* e la propaganda dell'opposizione. Grazie all'accordo, avremo tariffe più eque e trasparenti, più efficienza, più controlli e direi meno vite spezzate. Questo Governo ha affermato un principio, in passato troppo spesso calpestato: le infrastrutture sono un bene pubblico prezioso che deve essere garantito in modo responsabile garantendo sempre la sicurezza. stati premiati il lavoro di squadra, la fermezza del Presidente del Consiglio, il grande impegno dei Ministri, la collaborazione fattiva di tutte le forze di maggioranza anche nei passaggi più difficili. La mozione vuole dunque impegnare il Governo: a dare seguito a quanto deciso in sede di Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 in merito alla transazione di cui si è detto, chiarendo le tempistiche e la scansione temporale delle fasi di attuazione previste per la definizione della transazione con Autostrade per l'Italia (ASPI), fermo restando la risoluzione unilaterale della convenzione con ASPI in caso di mancato completamento dell'accordo transattivo, anche tenendo conto che le società coinvolte nell'accordo sono composte da una pluralità di azionisti; a garantire una costante e stringente vigilanza sull'operato del concessionario ASPI durante tutte le fasi di implementazione dell'accordo in relazione agli obblighi scaturenti dal rapporto concessorio e dalla transazione, in ragione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti; a garantire, in particolare, la realizzazione da parte del concessionario degli interventi essenziali per la messa in sicurezza e l'adeguamento tecnologico della rete autostradale, tenuto conto della necessità di ristabilire pienamente la tutela dell'interesse generale alla sicurezza come come obiettivo imprescindibile dell'azione pubblica e del rapporto concessorio, nonché il mantenimento degli attuali livelli occupazionali di Autostrade per l'Italia anche dopo la conclusione positiva dell'accordo transattivo in esame. in esame; 4) a garantire una migliore attuazione dei programmi di manutenzione delle infrastrutture affidate in concessione e un più efficace monitoraggio degli interventi realizzati, nonché ad assicurare e salvaguardare la trasparenza nell'azione delle società concessionarie o, in generale, del gestore dell'infrastruttura, anche mediante obblighi di puntuale e periodica pubblicazione di tutti gli atti e i dati idonei a permettere un controllo sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

dichiarazioni con annunci di revoca, ora si passa all'acquisto con fondi pubblici. L'acquisto viene descritto, almeno sui per il crollo del ponte Morandi e purtroppo per le vittime. La domanda che però ci poniamo, nella valutazione che

I soldi degli italiani, il risparmio postale è ben investito nella scelta politica di nazionalizzare Autostrade per l'Italia? Non corriamo il rischio che diventi un'altra Alitalia o come molte delle società a partecipazione statale di antica memoria? Il grande tema di questi giorni, oggi attuale ma anche per i prossimi giorni perché al momento non abbiamo ancora visto il cosiddetto memoriale che dovrebbe definire le modalità dell'accordo, è quanto costerà

o comunque del tutto appaiato, a quanto sarà fatto per i cosiddetti altri soci o soci preferiti. Non può esserci, in questo caso, un doppio peso tra il prezzo d'acquisto da parte di Cassa depositi e prestiti e i *partner*, i soci preferiti. Vi rendete conto, colleghi, che questa è un'operazione che è stata un po' confusa e in alcuni passaggi anche, se vogliamo, violenta, più violenta nelle dichiarazioni che nei fatti.

convinta a cedere - spontaneamente o spintaneamente dipende certamente dal prezzo - o lo Stato che dovrebbe fare e valutare l'interesse pubblico.

vi parla vorrebbe uno Stato che concentrasse i propri fondi più su scuola, ospedali, giustizia e difesa, ma ho il massimo rispetto per quella che può essere anche una scelta politica che però impone automaticamente nuovi CDA e relative vendette politiche. Noi ribadiamo: se c'erano colpe, dopo due anni dovevano essere chiarite e doveva esserci, nel caso, la revoca. Ora, però, si pongono alcune questioni. come vorrà il Governo indirizzarsi rispetto alla qualità delle future scelte aziendali? Con un comunicato stampa si dice già che si modificano le tariffe,

non vorrei che, su una dichiarazione di questo tipo, pagassero le autostrade quelli che le autostrade non le usano. Io vorrei che ci fosse questa valutazione da parte del Governo. Altro elemento che io ritengo rilevante è all'immagine di Paese e di politica anche industriale. I Benetton e gli altri soci hanno hanno guadagnato certamente moltissimo in Autostrade per l'Italia. Benetton, però, è anche un grande marchio nazionale, in particolare nel settore tessile. Qual è il danno d'immagine che il nostro Paese ha con un'operazione di questo genere? Io vorrei ricordare che, nel nostro Paese, sono stimati in 400 miliardi gli investimenti esteri su società che operano nel nostro Paese. Come leggeranno gli investitori esteri questo comportamento? Noi abbiamo già, come tutti voi, colleghi, sapete, un deterrente agli investimenti nel nostro Paese, che è il tempo della giustizia. D'altra parte, se dopo due anni non abbiamo ancora

Si fideranno ancora della parola degli italiani? Potremo dire che gli italiani hanno una sola parola? Dobbiamo porceli questi problemi. Naturalmente, dobbiamo porceli come Parlamento, indipendentemente da quello che deve fare, da parte sua, il Governo. Vengo Vengo ora a Cassa depositi e prestiti. Quest'operazione fa il paio con il decreto rilancio approvato settimana scorsa in quest'Aula. Signor Presidente, si sta utilizzando Cassa depositi e prestiti come un bancomat. Cassa depositi e prestiti è stata, nella storia di questo Paese, la banca che ha finanziato le opere pubbliche di Comuni e Province e le opere pubbliche in generale. Essa ha l'obbligo e il dovere di gestire bene il risparmio fiscale e, quindi, di investirlo in operazioni redditizie. redditizie. Può darsi che il sistema autostradale possa essere un'operazione redditizia. Non sappiamo quali saranno, invece, quelle del decreto rilancio, ma su questo poniamo la massima attenzione. attenzione. Su questa incertezza complessiva si legge sui giornali che la revoca non è ancora esclusa, anche perché non abbiamo ancora il documento finale. Serve forse a rassicurare i mercati? È un elemento che rassicura i mercati?

della comunicazione dell'accordo. La domanda è: va bene così? Non è, forse, turbativa di mercato? È poi possibile sapere chi ha comprato e chi ha venduto in quei due giorni, nei quali il Presidente del Consiglio e altri comunicavano l'intenzione di revoca e il titolo crollava? fa parte di quella stessa trasparenza cui hanno diritto gli italiani rispetto agli atti secretati degli accordi di Autostrade con il Ministero dei trasporti. Su questi temi, signor Presidente, noi poniamo la questione:

caducazione o di decadenza della concessione, come disse il buon Conte del Grillo che, un po' come la proverbiale sveglia che segna l'ora giusta due volte al giorno pur stando ferma, anche lui ogni tanto una cosa giusta Perché è importante fissare questo termine? Perché la concessione doveva decadere in conseguenza di una palese inadempienza e quindi, come tale, nulla sarebbe stato dovuto nei confronti del concessionario, cioè il concedente non gli doveva nulla. Se il concessionario avesse avuto qualche cosa di cui lamentarsi, il tribunale sarebbe stato la la prima domanda è: perché si è usato a un certo punto solo il termine «revoca»? Malafede? Diciamo che statisticamente, se tutti cominciano a parlare di revoca, il dubbio viene. Questo è il primo errore gravissimo che è stato fatto. Il secondo errore è stato quello di personalizzare la vicenda. Devo dire che questo l'ha fatto un solo partito: non l'ha fatto il PD, non l'ha fatto Italia Viva, non l'ha fatto la Lega, non l'ha fatto Fratelli d'Italia e non l'ha fatto Forza Italia. L'errore è consistito nel trasformare una questione di principio, cioè una palese inadempienza, in un fatto personale: ce l'abbiamo con l'azionista di maggioranza e vogliamo che esca. Questo i politici non lo devono fare, perché devono sempre agire secondo l'interesse pubblico e non secondo l'odio personale verso qualcuno. Ma andiamo avanti e vediamo un pochino, nel caso particolare, l'operazione finanziaria, quella formalizzata il 14 luglio. Com'è la situazione attuale? La situazione attuale è che l'88,06 per cento di ASPI è detenuto, in via diretta o indiretta, dalla famiglia Benetton, tramite la controllante Atlantia; il 5 per cento da Silk road fund (i cinesi) e il resto da una cosa che si chiama Appia investments Srl, che contiene Allianz e altri. L'operazione che si vuole mettere in campo funziona così: si farà un aumento di capitale dedicato, con iniezione di soldi pubblici, che non toglierà una sola azione al controllante ma semplicemente diluirà la sua quota. Quindi lo Stato metterà soldi freschi tramite la Cassa depositi e prestiti. Se allora lo scopo era estromettere il controllante si rilevava la sua quota azionaria; se non lo si fa è perché si mette nero su bianco che bisogna ricapitalizzare Autostrade. Poi vedremo perché bisogna ricapitalizzare. La seconda fase sarà che Atlantia dovrà cedere una parte delle sue quote, ma non al pubblico, bensì a degli investitori istituzionali che, contrariamente a quello che si pensa, non sono pubblici sono tipicamente fondi di investimento, cioè raccoglitori di risparmio privato. Se quindi l'operazione doveva essere quella di riportare in mano pubblica un bene pubblico come le concessioni, mi sa che non sta funzionando così.

quota. In questa operazione Atlantia non metterà quindi un centesimo; sarà una ricapitalizzazione e un'iniezione di fondi in Autostrade per la quale Atlantia non "caccerà" niente. luogo, si parla di uno scorporo con quotazione di autostrade, cioè di un'operazione di puro mercato. Lo Stato in questo momento non fa lo Stato ma si comporta come un operatore di mercato. Questo scorporo dovrebbe avvenire cedendo quote azionarie (se quoti vuol dire che metti delle azioni). Bene, queste azioni saranno quote di Cassa depositi e prestiti (*pro quota* per tutti) o sarà un altro aumento di capitale, quindi altri soldi raccattati sul mercato? Io credo la seconda delle due, perché resta il fatto che Autostrade per l'Italia ha tanti debiti (circa 10 miliardi di euro), che naturalmente andranno ridistribuiti *pro quota*; quindi una parte dei debiti Atlantia non li avrà più e li metterà in carico allo Stato.

almeno farei così, perché è l'unica operazione logica per qualcuno che vuole disimpegnarsi dall'investimento. Perché poi la quotazione? Per rimettere in mano al mercato ciò che tanto faticosamente si voleva riportare al pubblico? Bello! Si dichiara una cosa e poi se ne fa un'altra; il cattivo mercato che vuole la remunerazione del capitale. Quindi anche questa è un'operazione che apparentemente non ha senso. Ma non solo; in questo momento sono bloccati circa 15 miliardi di euro di investimenti sulla rete.

il controllante attuale non spenderà più per ricapitalizzazioni e per manutenzioni e i debiti pro quota, mi sembra che superiamo abbondantemente i 10 miliardi Tutto a fronte di 3,4 miliardi di euro di risarcimenti compensativi per non dover più parlare di altro. A me sembra che questo sia un grosso affare da parte di qualcuno che voleva liberarsi della propria quota. Tanto che va detto

per parlare anche di un'altra importante concessione in mano al gruppo Atlantia e quindi alla famiglia Benetton di cui si parla molto di meno. Mi riferisco cioè alle concessioni aeroportuali di ADR, ADR, Aeroporti di Roma, che riguarda le concessioni di Fiumicino e Ciampino, che sono anch'esse delle concessioni di beni pubblici pubblici costruiti con i soldi degli italiani e dati in concessione a dei privati con delle clausole particolarmente generose. generose. Volevo aprire una parentesi sul punto perché trovo alquanto bizzarro che mentre il Governo fa la voce cattiva con Atlantia e con i Benetton, dicendo che cose scandalose non saranno più permesse, nel frattempo sembra tramare nell'ombra per fare favori ai Benetton sulle concessioni aeroportuali di Roma. alcune questioni specifiche: nel cosiddetto decreto rilancio, un decreto-legge fatto per affrontare la grande emergenza del coronavirus, per fronteggiare la crisi economica che si abbatte e si abbatterà sull'Italia per aiutare chi è in ginocchio, all'ultimo momento la maggioranza ha introdotto un emendamento nel quale prevede la proroga di due anni di tutte le concessioni aeroportuali, compresa la concessione di Aeroporti di Roma che scadeva addirittura nel 2044 - già questa è una bestemmia - e che grazie al citato decreto-legge, per fronteggiare la crisi del coronavirus, verrà posticipata al 2046. O meglio, non verrà posticipata: è stata posticipata al 2046. Visto che in quest'Aula «Il Fatto Quotidiano» viene usato come fonte di diritto, come abbiamo visto fare prima a colleghi del MoVimento 5 Stelle, ebbene la fonte di diritto «Il Fatto Quotidiano» dice che questa proroga di due anni equivale a un regalo di un miliardo di euro alla famiglia Benetton.

pubblica il piano Italia veloce; un piano con le grandi opere che il Governo intende realizzare e velocizzare. Tra queste grandi opere, nell'elenco pubblicato il 12 giugno e presentato agli Stati generali di Villa Pamphilj, appare anche il raddoppio del sedime aeroportuale di Fiumicino, perché viene espressamente inserita la dicitura «realizzazione quarta pista e adeguamento dell'area dell'area aeroportuale», che è esattamente quella riportata nel *master plan* di Fiumicino, che prevede il raddoppio del sedime aeroportuale. In spregio al buonsenso e a quanto stabilito in ogni sede dai tribunali italiani, e cioè che il sedime aeroportuale di Fiumicino non può essere raddoppiato perché va a incidere su una riserva naturale di massima tutela, nonostante quindi legge e la Costituzione non prevedano la possibilità di farci sopra una colata di cemento, il Governo, che "abbaia alla luna" contro i Benetton, nel piano Italia veloce inserisce il raddoppio del sedime aeroportuale di Fiumicino.

è più che sufficiente portare il traffico dagli attuali 40 milioni a 80-100 milioni di passeggeri, come si vorrebbe fare, in quanto Fiumicino ha già tre piste attive, oltre a quelle di rollaggio.

di cinque piste. Si può dire che non c'è nulla di losco, se non fosse che per fare il raddoppio del sedime aeroportuale di Fiumicino vengono destinate le risorse

indicata dal piano realizzato nel 2012. Invece viene eliminato il terzo aeroporto del Lazio e vengono incentrate tutte le risorse su Fiumicino, in modo da creare un grande mostro per continuare a permettere speculazioni ai soliti noti, a discapito anche delle nostre riserve naturali, a discapito del trasporto aereo e anche di Alitalia, perché tutti sanno benissimo che concentrare le compagnie *low cost* a Fiumicino ha comportato la morte attuale di Alitalia. Questo è il pacchetto che era stato realizzato. Non a caso, il 12 giugno viene pubblicato il piano Italia veloce e il 25 giugno il Governo decide di annullare la risposta in Aula a una mia interrogazione a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia proprio sulla riserva naturale del litorale romano. A seguito di questo, sale la polemica sui *media*, che titolano in diversi articoli «regalo ai Benetton»

il piano Italia veloce, facendo scomparire quello del 12 giugno e pubblicandone uno nuovo datato 7 luglio, nel quale scompare momentaneamente il raddoppio di Fiumicino;

c'è chi ha l'anello al naso, va bene che c'è gente che gira con la sveglia al collo, ma non proprio tutti gli italiani sono sprovvisti di un collegamento Internet e della possibilità di andare a verificare le modifiche che sono state apportate a un sito Internet e vedere che, beccato con le mani nella marmellata a fare l'ennesimo regalo ai Benetton, il Governo ha dovuto fare marcia indietro e ritirare il riferimento al raddoppio dell'aeroporto di Fiumicino. Poi in fase di dichiarazione di voto ci esprimeremo nello specifico sulla situazione delle concessioni autostradali, però se questo è il *modus operandi* non andiamo molto lontano. Se quando i riflettori vengono accesi su un'anomalia si cerca di fare qualcosa senza disturbare troppo, ma poi, appena possibile, continuano i regali, non andiamo lontano. Pertanto, almeno su questo per l'ennesima volta Fratelli d'Italia ha sventato un'ignobile speculazione sull'area della riserva naturale del litorale romano. Speriamo che qualcuno non ci riprovi.

tutti gli italiani che hanno visto le immagini del crollo del ponte di Genova e hanno saputo delle numerose vittime che ci sono state. da questa vicenda sta venendo fuori un'operazione che non risolve nessuno dei problemi e ne crea degli altri. Per due anni si è parlato della revoca delle concessioni Per due anni si è parlato della revoca delle concessioni su questi 3.020 chilometri di autostrade. Più della metà delle autostrade italiane è racchiusa in questa concessione che a suo tempo fu data senza nessuna procedura competitiva, solo con operazioni finanziarie, dove coloro che avrebbero dovuto mettere i capitali sono stati piuttosto bravi a prenderli e non a mettercene

e si è arrivati a questa sorta di compromesso per cui forse (perché qui siamo soprattutto all'annuncio) ci sarà la del tutto opinabile soddisfazione di vedere la famiglia Bénetton (o Benettòn come la filologia suggerisce si dovrebbe pronunciare questo nome) fuori dall'azionariato di Atlantia, e dunque di Autostrade per l'Italia, però a caro prezzo. E chi mette i soldi per comprare le loro quote azionarie, atteso che l'esproprio evidentemente non dovrebbe essere previsto, anche in base alla Costituzione che tutela l'impresa privata? I soldi dovrebbero metterli gli italiani, cioè i contribuenti italiani. Dunque,

dà una cifra molto grossa a coloro che sono stati indicati come i principali colpevoli. Intanto sarebbe opportuno vedere tutte le collaborazioni che ci sono state anche a livello ministeriale, perché bisogna ricordare che tutte le autostrade italiane sono proprietà dello Stato e non dei concessionari, concessionari, i quali hanno dei contratti che dovrebbero onorare; la maggior parte delle volte lo fanno, quando non lo fanno poi di solito vengono premiati, come abbiamo visto con la vicenda della tratta Il fatto di mettere soldi dei risparmiatori italiani in un'azienda è veramente folle, in questo periodo: lo Stato italiano ha bisogno di soldi per i mille interventi che ci vengono chiesti, in particolare in questo periodo di crisi. Cosa si fa? Anziché intervenire a sostegno delle piccole, medie e grandi aziende, aziende, che hanno bisogno di fare investimenti per stare al passo con la concorrenza internazionale; anziché sostenerle in questo momento difficilissimo, in cui hanno problemi drammatici di liquidità, dove si mettono i soldi di Cassa depositi e prestiti? Per pagare la famiglia Benetton, in modo che qualcuno abbia la soddisfazione di dire: «I Benetton sono stati cacciati via dalle Autostrade». A quale prezzo? Non lo sappiamo: calcoli ragionevoli, che sono in corso, ci parlano di cifre molto, ma molto alte. Non si capisce veramente la logica, dunque. non sarebbe più logico fare quello che i principi della concorrenza e della convenienza per i cittadini suggerirebbero, ossia di fare una gara, come se ne sono fatte tante per società pubbliche,

tutela dell'occupazione, l'efficienza nella gestione di quest'azienda e di questa grande attività), in modo che non vada in passivo. Autostrade per l'Italia, infatti, ha avuto profitti enormi e un margine operativo lordo

per mettere su una società statalizzata (si ritorna alla vecchia IRI, che fu fondata durante il fascismo e poi in seguito ha fatto molte

dei maggiori azionisti di Autostrade di uscire dall'azionariato? Si faccia una gara, perché le autostrade sono proprietà dei cittadini italiani *(Applausi)*, non dei signori che gestiscono Cassa depositi e prestiti. Che razza di criterio è

chi è buono e chi è cattivo; ma esistono dei principi di concorrenza e non sono principi astratti bensì per la convenienza: avete presente come sono cambiati i prezzi della telefonia da quando c'era il monopolio a quando c'è la concorrenza?

perché subito dopo salterà fuori che la cifra da dare ai famosi azionisti è troppo alta e perché quest'accordo è talmente vago che in realtà non è tale. Più che altro si è trovato l'accordo sul comunicato stampa da fare alla fine del Consiglio dei ministri. Qui ci vogliono invece soluzioni serie, in quanto bisogna tutelare l'occupazione e una realtà finanziaria e imprenditoriale che è molto importante per il Paese, indipendentemente da come può essere stata gestita e dalle carenze che ci sono state. Bisogna tutelare tutti gli aspetti, nell'interesse

dunque soluzioni efficienti al passo con i tempi e non soluzioni stataliste che probabilmente servono per collocare qualche amico su qualche poltrona in qualche consiglio di amministrazione. Infatti, si riducono i parlamentari ma si aumentano i posti per persone parassitarie non elette da nessuno, che fanno il danno del Paese.

incrementare le proprie entrate in estrema difficoltà. È evidente che i tempi di percorrenza delle nostre autostrade siano fuori da ogni controllo.

doveva andare fino a Bolzaneto e fare un giro tipo Asterix. Avete presente quando Asterix girava e non trovava una via d'uscita? Ecco, si doveva rientrare e si perdeva un sacco di tempo. C'è un aspetto che fa ancora più specie.

10 ottobre, con sotto il parcheggio delle aziende pieno, con la coda che io ho fatto decine e decine di volte su quel tratto, probabilmente non saremmo a contare le 43 vittime - che sono un disastro, fosse anche una soltanto - ma sarebbero molte di più.

800 milioni di euro; sembrava un grande evento industriale, e poi cos'è accaduto? Che l'evento industriale si è trasformato in un quasi un quasi fallimento della Piaggio. Quindi, il problema che noi ci poniamo in questo momento, reale, tangibile,

È evidente che l'annuncio che CDP poteva entrare all'interno della *governance* ha fatto in modo che le azioni

rispetto a chi oggi non ha manutenuto le autostrade italiane. Colleghi, stiamo parlando del tratto - che io faccio più spesso - che va da Ponente a Levante, ma il tratto che va da Voltri verso la Lombardia è parecchio messo male. Se arrivo ad Arenzano e sono in coda perché la gente sta per andare a Milano, e non riesce a uscire perché c'è una sola carreggiata con i tir che vanno a 20 all'ora, questo è un grosso problema. La situazione che è venuta a generarsi ha di fatto immobilizzato la mia terra dal punto di vista economico. Le perdite non si contano: si parla di un miliardo di euro al mese. Ciò vale

soprattutto, di mettere al centro dell'attenzione puntuale e precisa gli investitori istituzionali della CDP (che non devono essere messi in condizione di avere delle perdite),

i cittadini liguri che hanno subito il crollo del ponte Morandi, le mareggiate che hanno devastato le nostre coste il crollo del ponte sulla A6 chiedono e, anzi, pretendono di sapere chi paga i debiti dei Benetton. Lo vogliamo sapere. Non lo vuole sapere Ripamonti o la Lega: credo lo vogliano sapere gli elettori di tutti i partiti che si chiamano cittadini italiani.

perché noi abbiamo almeno tre profili da recuperare e da coltivare per quanto riguarda questa gigantesca questione che si può definire in vari modi: «rottura di civiltà inferta alla Liguria», «situazione di dolore sanguinante che ha riguardato la città di Genova», ma anche, in termini più generali, «condizione delle principali infrastrutture dell'Italia» dopo che, per un certo numero di anni, la distrazione e la superficialità non hanno voluto prendere atto che le infrastrutture italiane per la mobilità tradizionale avevano superato la loro vita tecnica. C'è un luogo in Italia che si chiama Consiglio superiore dei lavori pubblici. In un Paese nel quale purtroppo è valso solo il Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio superiore dei lavori pubblici stabilì nel 1968 che le infrastrutture per la mobilità hanno come vita tecnica cinquanta

Sarebbe servito che, a un certo punto, questo tema dovesse e potesse entrare nell'agenda del Paese, ma anche in quella dell'ordinamento europeista,

È accaduto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha rivisto la vita tecnica delle infrastrutture e sul nuovo adesso serve garantire cento anni di vita, esattamente il doppio. Ciò chiama a una sfida che non è quella del "parlatoio" della politica, ma del Parlamento della politica. Non si tratta di organizzare il buttare qui e lì delle parole giusto per marcare un'esistenza di partito, partito, ma di curare un'agenda di priorità che abbia risorse finanziarie e da ieri finalmente abbiamo risorse finanziarie all'altezza. Si tratta di concepire procedure.

ma attenzione a immaginare ovunque, per ogni dove e per ogni banco di scuola, un commissario: poi si svilisce il ruolo del commissario che serve per necessità. necessità. Dobbiamo sapere, allora, che in questo momento c'è una grande questione che riguarda la Liguria, Genova e l'insieme dei territori dell'Italia. La terza corsia dell'autostrada è una priorità per fare in modo che lungo le strade non si coltivino le morti, perché nel momento in cui ci siamo candidati abbiamo accettato di essere operatori della vita, non operatori della cultura della morte come allo stato attuale, se non si dà luogo ad una sveglia che sospenda la lotta politica purché si determini il conflitto e generi invece una cantierizzazione al futuro di ciò che serve all'Italia. Lavoro all'ANAS e ho curato per anni l'agenda delle cose da fare di uno dei migliori dell'ANAS, l'ingegner Michele Minenna, uomo nato con gli stivali nei cantieri e uomo che ha concepito le migliori infrastrutture realizzate in Italia, uno che lamentava negli anni lontani e passati che la Direzione generale per la vigilanza autostradale dovesse avere risorse umane e tecnologiche, altrimenti la piramide è sbagliata, tanto da fare con niente o poco per vigilare. Anche questo è il tema di Genova, delle sue infrastrutture, della Liguria e dell'Italia. C'è un contenzioso *dossier-*partita riguardante il profilo giuspenalistico di cui si occupano i magistrati e mi sembra con serietà. Finalmente li vorrei vedere con questo rigore ovunque in Italia; solo il merito e non la scomparsa della verità davanti alla verosimiglianza. Poi c'è una questione contrattuale di cui si sta occupando anche il Governo con risolutezza, perché l'idea di quella questione selettiva contrattuale è oggettivamente intelligente. Infine c'è una questione gestionale, che non è ancora affrontata, perché dire che se ne occupa l'ANAS non significa dire che se ne occupa la gendarmeria di Stanlio e Olio. Serve organizzare numeri, competenze e adeguatezza di competenze, perché non ci vuole nulla a determinare un chilometro di strada come un chilometro di lastre per la morte. Ecco perché il dibattito di oggi deve essere fertilità delle procedure decisionali, normative e amministrative che servono. Per troppo tempo abbiamo pensato che ci pensasse lo Spirito Santo. Conosco con

Financo questo è mancato in alcuni anni lontani e passati. Vivo in una Regione dove la mancanza del PEF, il nuovo piano economico finanziario, non consente alle gallerie abruzzesi (ma è il tema di tutte le gallerie italiane) di ritrovare resistenza e sicurezza. C'è una grande questione che riguarda anche le gallerie. Qui abbiamo un Sottosegretario che non è un tirocinante preso a caso, ma è un professore universitario di ingegneria che ha fatto anche libera professione e mi può venire incontro sul fatto che le opere d'arte in Italia hanno tutte bisogno di ritrovamento di capacità di funzionamento. Nel decreto-legge Genova il ministro Toninelli ha previsto una norma che non è entrata nel patrimonio di soddisfazione della classe dirigente: è una norma che prevede finalmente il catasto delle opere d'arte in Italia, che non sono le opere dell'estetica o le opere della bellezza, ma le opere della complessità realizzativa, i nodi che possono mettere a rischio il funzionamento di una struttura. Gallerie, ponti, viadotti: finalmente abbiamo il quadro - lo dovremmo avere oggi, perché è nata anche una direzione generale dedicata a questo - che ci fa capire, anche presuntivamente, quanto ci serve l'anno prossimo, quanto fra tre anni e quanto fra sei anni. Serve però organizzare un flusso di attenzioni. Ecco perché l'iniziativa del dibattito di oggi fa bene e serve che venga versato in atti presso il Ministero delle infrastrutture. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete riservato, sperando

il risultato di un'azione politica di governo si deve valutare sulla base delle condizioni date e sulla vicenda le condizioni date sono le seguenti: una convenzione una convenzione in atto, approvata nel 2008 da un Parlamento nel quale nessuno degli attuali componenti della maggioranza votò in maniera favorevole; fu invece votata da personalità importanti e da partiti che oggi sono all'opposizione. Quella convenzione era favorevole al concessionario sia per le condizioni generali e, ancor di più, per la clausola di risarcimento in caso di rescissione. Contemporaneamente, tenuto conto quindi di una convenzione di questo tipo, c'era e c'è la necessità di intervenire, dato il tragico e inaccettabile episodio di Genova e l'evidente insufficienza di monitoraggio e manutenzione che in questi anni vi è stata, anche in virtù della convenzione a cui prima facevo riferimento. La soluzione trovata evita il rischio di un contenzioso soccombente per il Paese per un importo che poteva variare tra i 7 e i 23 miliardi; evita i rischi di perdita di posti di lavoro, di impoverimento di *know-how* di una società; evita le difficoltà nel subentro del nuovo concessionario; allo stesso tempo, garantisce l'accettazione delle tariffe stabilite dall'ART. Lo dico ad un collega che sulle tariffe prima è intervenuto quasi fossero tariffe vessatorie: sono tariffe che vengono fuori da un calcolo fatto dalla *Authority* di regolazione dei trasporti. Non solo, vi è l'accettazione di un meccanismo per la remunerazione degli investimenti solo dopo che essi siano stati fatti e non prima, perché la convenzione, tanto favorevole e vantaggiosa, prevedeva persino che potessero essere pagati gli investimenti prima che essi venissero fatti e magari anche quando non venivano fatti. Non succederà più. prevedono 14,5 miliardi di euro di nuovi investimenti; 7 miliardi di euro per manutenzioni, quanto mai necessarie, come ricordato un attimo fa dal senatore d'Alfonso, che ringrazio; 3,4 miliardi di euro di risarcimenti in vari attraverso un meccanismo finanziario il cui *driver* principale è Cassa depositi e prestiti, consente di determinare un'uscita graduale e totale dell'attuale proprietà (altra priorità priorità del dibattito di questa fase). Ecco, se un risultato va valutato nelle condizioni date, ritengo di poter dire che nelle condizioni date il Governo e la maggioranza hanno conseguito un ottimo risultato, forse il miglior risultato possibile.

vorrei approfittare di questa circostanza per provare a guardare in modo un po' più vasto la questione, sperando il Parlamento voglia considerare il tema delle concessioni nel suo insieme e non guardare sempre solamente al dettaglio. Il 14 agosto 2018 è crollato il ponte Morandi, provocando 43 morti e 566 sfollati, un enorme danno economico e un enorme danno di immagine per l'intera Nazione. è emersa una situazione inaccettabile che riguardava le concessioni autostradali, ma in generale le concessioni in Italia, con ricavi enormi per i concessionari, manutenzioni non fatte, investimenti non fatti e accordi capestro in base il concessionario, anche se non rispetta la propria parte di contratto, non è sottoposto a nessuna penale né situazione particolare, anzi, qualora lo Stato volesse revocare la concessione per inadempienza, dovrebbe riconoscere al concessionario tutti i mancati ricavi dal momento della della revoca fino alla fine della concessione. Una situazione completamente folle, della quale le responsabilità sono molte e sono diluite negli anni, ma una cosa è certa:

A seguito di una situazione così grave, in tutto il mondo, dalle Isole Samoa al Cile, dal Sudafrica all'Islanda avrebbero revocato le concessioni autostradali. In Italia no. In Italia le concessioni autostradali sono rimaste in capo allo stesso concessionario responsabile, non sappiamo se penalmente ma sicuramente in qualità di concessionario, del crollo del ponte. Il Governo ha deciso Il Governo ha deciso di lasciare il *dossier* nel cassetto e di non affrontarlo, salvo poi ritrovarsi, a ridosso della necessità di apertura del nuovo ponte di Genova, a doverlo assegnare a qualcuno e a dover fare, quindi, un Consiglio dei ministri durante

Sembrerebbe di no, perché i titoli di Atlantia, principale azionista della concessione, che erano crollati a seguito di una paventata revoca annunciata dal Governo, sono poi schizzati verso l'alto e ritornati ai livelli precedenti la dichiarazione, quando l'accordo è stato chiuso. Quindi è difficile pensare che gli investitori del pianeta abbiano male inteso il nuovo accordo e che abbia ragione chi sostiene che l'accordo penalizza in modo particolare gli attuali azionisti. Più probabile pensare che l'accordo sia molto vantaggioso per gli attuali azionisti. era l'occasione per affrontare il tema delle concessioni anche con una visuale storica. Permettetemi questo parallelismo: caduta la contrapposizione tra i blocchi, abbiamo assistito, in Unione Sovietica alla nascita degli oligarchi, cioè dei privati ai quali veniva assegnata, in virtù di particolari rapporti con la politica, la concessione dello sfruttamento

Una forma di capitalismo talmente malata che lo stesso Putin, all'inizio del suo secondo mandato nel 2004, dichiara guerra agli oligarchi, dicendo i pozzi di petrolio sono dei russi e non proprietà privata dell'oligarca. In Italia, finita la contrapposizione tra i blocchi, e con la debolezza della politica, è accaduta esattamente la stessa cosa.

i pozzi di petrolio nostrani, con le autostrade date ai Benetton e la svendita dell'Eni e di Telecom, un fenomeno nel quale il parallelismo è totale. Nel periodo di concessione delle autostrade, autostrade, l'utile incassato e in gran parte tramutato in dividendi per gli azionisti è di 10 miliardi. Il patrimonio stimato di Abramovich è di 10 miliardi: questo è. Noi abbiamo consegnato i nostri pozzi di petrolio alle *lobby* e ai potentati economici italiani, con accordi che non andavano a premiare l'interesse pubblico, ma andavano semplicemente a fare *extra* profitti per i soliti noti. Questo era il problema che noi avremmo dovuto, come Nazione, affrontare il giorno dopo il crollo del ponte Morandi, cosa che non abbiamo fatto.

indirizzare, però, tutte le colpe di quanto accaduto alla singola proprietà sembra quasi il gioco di chi vuole non affrontare il problema, drammatico, delle concessioni in Italia, che non riguardano solo quelle tratte autostradali, ma anche altre, che riguardano interamente le nostre infrastrutture strategiche, che riguardano gli aeroporti, che riguardano tutto questo sistema malato di privatizzazioni fasulle, che hanno dato sistemi di monopolio su beni pubblici per far fare profitto ai privati. Questo avremmo dovuto affrontare e questo il Governo non ha affrontato e questo il Governo continua a non affrontare. Che cosa avremmo dovuto fare? Azzerare tutte le concessioni. Revoca della concessione di autostrade, ma non solo: azzeramento di tutte le concessioni presenti in Italia e nuova gara, con regole che che rispettino il nostro Stato di diritto, perché la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, la Corte costituzionale, in diverse fasi, hanno dichiarato che le attuali concessioni esistenti in Italia non rispettano le basilari norme del diritto italiano. Non esiste un contratto di diritto civile che prevede che uno dei due contraenti possa non rispettare la sua parte di contratto. banalmente le concessioni sono nulle; banalmente, le concessioni autostradali possono essere revocate, cosa che non è stata fatta. Fratelli d'Italia aveva presentato, nel 2018, una risoluzione, chiedendo, in base alle infrastrutture strategiche, di introdurre il principio di tutela dell'interesse nazionale. Dispiace che l'allora ministro Toninelli abbia espresso parere contrario e che la risoluzione sia stata bocciata. Abbiamo provato a ripresentare tale principio anche con questa mozione: Fratelli d'Italia chiede che, in sostanza, con le nostre infrastrutture e con le nostre concessioni, avvenga ciò che avviene in tutto il resto del mondo e che mette in atto chiunque voglia tutelare il proprio interesse. In primo luogo, chiediamo la proprietà pubblica delle infrastrutture strategiche; è il caso di Autostrade, ma non è il caso, ad esempio, della rete di telecomunicazioni. Chiediamo inoltre la gestione pubblica o privata delle infrastrutture di proprietà pubblica, ma con la clausola di salvaguardia dell'interesse nazionale. Se il Presidente mi concede soltanto 30 secondi, provo a sintetizzare Chiediamo che per una concessione privata ci sia un vantaggio oggettivo e certificato per lo Stato rispetto alla gestione diretta dello Stato, chiediamo che sia garantita la sicurezza nazionale attraverso l'obbligo per i gestori di avere la sede legale e fiscale in Italia, di risoluzione unilaterale da parte dello Stato in caso di gravi inadempimenti (questa dovrebbe essere una banalità) e chiediamo infine che ci sia l'obbligo, per il contraente, di reinvestire nelle infrastrutture non solo quello che è già previsto da contratto, tutto ciò che eccede il 15 per cento dell'utile netto (e andiamo a spiegare ai nostri imprenditori che un utile netto è accettabile del 50-60 per cento, come avviene per i nostri concessionari). Chiediamo che questo sia approvato. A nostro avviso, l'unica possibilità per mettere fine a questa vergogna del saccheggio sulle nostre infrastrutture strategiche è la revoca di tutte le concessioni e l'indizione di nuove gare sulla base di contratti seri e certi. I più bravi se li aggiudicheranno.

del Governo, oggi affrontiamo una questione particolare, che ha investito e ancora investe le sorti del nostro Paese su più fronti. In quasi due anni ci siamo ritrovati a dover rimettere in piedi non solo un'infrastruttura, quella del ponte Morandi, necessaria alla città di Genova e a tutta la Liguria, ma anche ad affrontare i risvolti di una crisi economica improvvisa, che, unita al blocco di un'arteria fondamentale di sviluppo anche per uno dei porti più importanti d'Italia, può risultare fatale per famiglie e imprese. A poche settimane dalla riapertura del ponte al pubblico, dobbiamo ancora discutere se sia più conveniente continuare a incastrare la macchina pubblica in un vortice infinito di burocrazia e tempi della magistratura oppure optare, oserei dire in modo più intelligente, per una riassegnazione chiara delle responsabilità e un alleggerimento rapido di quelle procedure che in questo momento bloccano l'intero Paese. È vero, abbiamo fatto passi da gigante, predisponendo in emergenza misure di velocizzazione per tante opere infrastrutturali fondamentali, come peraltro noi di Italia Viva avevamo già previsto con il piano *shock* presentato al Governo in tempi non sospetti. Ma ora, al di là di tutto, è il momento di dimostrare non solo all'Italia, ma a tutta l'Europa, che rinnovarsi e ripartire è possibile. Ora non possiamo più restare a casa, ma direi soprattutto che non possiamo più continuare, in maniera semplicistica, a insistere sul mandare a casa casa qualcuno, permettendo il protrarsi di situazioni volte a invocare unicamente la procedura di revoca della concessione ad ASPI, senza considerare null'altro. L'operazione forse sotto il profilo mediatico è sembrata efficace, ma poi, a nostro parere, non è risultata altrettanto soddisfacente durante le trattative di mediazione, limitando di molto la sua apparente forza. Colleghi, non abbiamo ancora, seppure possiamo immaginarlo, una definizione completa dello scenario burocratico che si potrebbe prospettare in caso di revoca della concessione. Ad oggi non si è velocizzato alcun procedimento e non sono stati realizzati nuovi investimenti e potenziamenti ai quali concessionario era tenuto. Fino a questo momento sono costanti solo le difficoltà dei cittadini e della Regione Liguria, che si trova sommersa da una situazione di estrema difficoltà nella programmazione dei lavori per il miglioramento delle proprie infrastrutture, bloccando così di fatto sia il trasporto delle merci, sia il turismo, e sommando a questi danni quelli provocati dall'emergenza epidemiologica Covid-19, che purtroppo sembra protrarsi più del dovuto. Mentre le proiezioni del PIL colano a picco, si continua da qualche parte con un tira e molla inutile, dando adito a uno scaricabarile pressoché infinito, piuttosto che mettere davanti alle proprie responsabilità chi finora aveva l'obbligo di manutenzionare e innovare le nostre arterie di asfalto. Scaricabarile, sì, perché non abbiamo una prospettiva immediata su cosa succederà in futuro sul tema delle concessioni o non vogliamo rendercene conto. A fronte di eventuali nuovi disagi che potrebbero colpire le nostre infrastrutture, consentiremmo ad un nuovo, ipotetico e presunto concessionario di spendere ulteriori soldi pubblici per riparare i danni cagionati da altri in precedenza, liberando così le tanto famigerate *lobby* da una responsabilità enorme, facendo quasi un favore a chi è stato negligente in passato. È necessario mettere mano ad un pacchetto di misure straordinarie che consenta all'economia intera di ripartire con lo sblocco, seppure nelle more degli accordi, degli investimenti già programmati e autorizzati da ASPI, affinché non si ritardi ulteriormente nella necessaria evoluzione delle nostre infrastrutture, che non possono più aspettare le lungaggini della burocrazia e le indecisioni della politica, che invece deve farsi carico di ogni decisione. Per evitare che questa emergenza economico-sanitaria si trasformi in un disastro economico e sociale e si vada oltre il 10 per cento di calo del PIL previsto dagli osservatori finanziari, il settore degli investimenti nelle infrastrutture deve essere adeguato, rafforzando l'impianto già previsto dei commissari straordinari, che gestendo direttamente le procedure con speciali poteri, come avvenne per Expo Milano 2015 e, più recentemente, è avvenuto con il ponte Morandi, ma che ora dovrebbero rientrare in una cornice normativa ordinaria, possano semplificare quella mole pachidermica di passaggi burocratici, consentendo un celere avvio dei lavori dei lavori con nuove opportunità occupazionali, che diano finalmente la possibilità al Paese di risollevarsi economicamente e dignitosamente. Lo abbiamo detto in tutte le salse in questi ultimi mesi: ce la faremo, ma ce la faremo solo davanti non ad un programma ambizioso, non ad una visione egoistica della politica, ma davanti a un futuro che è già presente ed è dato dalle opere già cantierabili autorizzate e finanziate. È un segnale importante da mandare al Paese per far comprendere che la politica oggi può e deve mettere da parte una discussione sostanzialmente sterile, come quella di una continua trattativa per nuovi concessionari, quando bisogna con serietà e mantenendo intatto qualsiasi livello di sicurezza, mettere di fronte alle responsabilità vere chi è già in grado di poter operare, pur attuando tutti i controlli e le verifiche possibili e intervenendo con ogni misura consentita dalle leggi vigenti. Sono troppe le opere ferme da tempo immemorabile nel nostro Paese ed è ora che il Governo intero possa finalmente dare una sterzata a questa corrente di immobilismo, partendo proprio dalla Liguria, liberando le difficoltà che affliggono la ripartenza e concedendo il via libera ad un progetto fondamentale per questa Regione. Mi riferisco qui all'adeguamento del nodo stradale e autostradale di Genova comprensivo della Gronda, per cui ci auguriamo si segua il progetto unitario previsto dalla convenzione, con anche l'immediata conclusione dei blocchi stradali che attualmente interessano la Regione. Si tratterebbe di 65 chilometri che servirebbero ad alleggerire il traffico in una zona fortemente sollecitata. Lo dico *in primis* a me stessa e poi a tutti i colleghi di maggioranza e di minoranza, con i quali lavoriamo senza sosta per far intravedere una speranza di futuro migliore ai nostri giovani: non sprechiamo altro tempo, vacillando sulle spalle di un mostro politico e burocratico che ha divorato i nostri conti pubblici e ha permesso il verificarsi di questi accadimenti tragici che in un Paese non dovrebbero esistere. Abbiamo tutti l'unico interesse di risollevare la nostra Italia, le famiglie, le imprese private e pubbliche e, non ultimi, i lavoratori che stanno dietro le quinte di queste grandi opere a rischiare la propria vita, uomini che non vorrebbero vivere di redditi di sostentamento, ma che chiedono dignità. Quella dignità che può venire solo dal lavoro, che se ben fatto e retribuito, li fa sentire orgogliosi di aver contribuito, ognuno nel proprio piccolo, al miglioramento della società. Non sprechiamo questi sacrifici e, in nome di quanti si adoperano per la crescita sana dell'Italia, chiediamo al Governo di valutare con attenzione e interesse e mettere in pratica le proposte della mozione di maggioranza oggi discussa, comprensiva delle istanze di tutti per il buon governo dell'Italia, e fiduciosi che anche le proposte di Italia Viva-PSI abbiano un adeguato riscontro, dichiariamo il nostro voto favorevole.

- sono anni che poniamo la questione del sistema delle concessioni autostradali nel nostro Paese - che stiamo parlando della gestione di un bene assolutamente pubblico, che ha costruito, in tutti questi anni di sistema delle concessioni profitti enormi in capo ai concessionari. Vorrei anche ricordare che addirittura abbiamo avuto il caso di concessioni (sono moltissime le concessioni) le cui convenzioni addirittura avevano gli *omissis*, cioè persino noi parlamentari non eravamo in grado di vedere e verificare tutte quante le clausole.

Sappiamo anche che, nel prosieguo del dibattito, molti di coloro che adesso si stracciano le vesti sull'accordo che è stato raggiunto

Per la verità, continuiamo a sentire gli accenti di una sorta di pregiudizio incredibile sulla presenza dello Stato nella gestione delle autostrade e anche un pregiudizio che è del tutto ideologico contro l'idea stessa di *public company.* Venendo al merito,

luogo perché sotto il profilo dell'assetto societario si profila l'immediato passaggio dal controllo di ASPI ad un soggetto partecipato, come la Cassa depositi e prestiti, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato da parte di Cassa depositi e prestiti e l'acquisto di quote partecipative da parte di investitori istituzionali, ma che devono essere anche questi di gradimento di Cassa depositi

Questi due anni sono stati contraddistinti da un contenzioso e da ricorsi. Questo anche rispetto all'intervento all'interno del decreto milleproroghe, perché vi era stato persino

transazione è quello delle misure compensative. L'altra cosa importante riguarda il tema della sicurezza, che è l'altro elemento del tutto scoperto sul sistema delle concessioni e in particolare nel caso di ASPI, che tra l'altro detiene una quota

dal punto di vista dei controlli e della sicurezza. Il rafforzamento dei controlli a carico del concessionario è certamente uno degli elementi fondanti di questo accordo, come anche l'aumento delle sanzioni in caso di violazioni, anche lievi, da parte

molto rispondente a quello che era necessario mettere in campo per la tutela dell'interesse pubblico. Anche sulle tariffe dei pedaggi c'è un

dal Consiglio dei ministri, ma di adoperarsi per continuare sulla strada di un controllo molto serrato di vigilanza sul concessionario, anche durante tutte queste fasi di transazione e di implementazione dell'accordo, e soprattutto di garantire immediatamente la realizzazione degli interventi essenziali per la messa in sicurezza. questo riguarda il caso ASPI, ma - per noi questo è molto importante - credo che questa transazione e tutta la discussione svolta anche in

oggi. Abbiamo solo ed esclusivamente il compito di guardare avanti e cercare di capire come portare a termine un'operazione strategica per la gestione di quelle concessioni.

che entrasse in carica questo Governo. Non è serio da parte di alcune forze politiche far finta di nulla o che queste cose cadano dal nulla, perché si dà la sgradevole sensazione che le scelte adottate a quel tempo siano state fatte non per cercare la verità, bensì per rispondere all'emotività del momento, che è la cosa più brutta.

di quella concessione. Da qui la soluzione che conosciamo e l'accordo di cui stiamo parlando. Quindi il teatrino della propaganda e questi messaggi

acquistare e vendere le azioni, coinvolgere tanti altri soggetti investitori istituzionali e quotarsi in borsa, quindi garantire anche una certa contendibilità, e magari in futuro anche fuoriuscire, penso sia difficile trovare una soluzione diversa e più conveniente per far funzionare questo sistema e garantire tutti coloro che investono adesso e investiranno in futuro. In certi momenti, come in quello che stiamo vivendo, misure straordinarie come queste probabilmente fanno il bene del Paese e di coloro che investono e devono attraversare queste autostrade. È sotto gli occhi di tutti che questa è l'occasione migliore per superare l'assetto che non ha garantito le cose alle quali sto facendo riferimento e che soprattutto garantirà un equilibrio che solo questo tipo di soluzione può In un determinato periodo o in presenza di determinate condizioni, come quelle che abbiamo visto su questa concessione, non è sbagliato che lo Stato intervenga entri nelle compagnie per avviare un lavoro diverso rispetto al passato; anzi, è proprio lo Stato a garantire un certo grado di affidabilità

lo Stato torna imprenditore e si dice che è il peggior segnale verso tutti gli imprenditori istituzionali. E perché mai? Si presuppone che tutti gli investitori si comportino come il concessionario negli ultimi anni?

l'affermazione più chiara ed evidente dell'interesse pubblico, che ritengo essere un fatto di valenza culturale in una fase storica come quella che stiamo vivendo. un'altra domanda alla quale bisogna dare risposta - stiamo buttando via i soldi degli italiani per un'operazione ideologica? Mi sono divertito anche stamattina a vedere le quotazioni negli ultimi anni di di ASPI. Faccio fatica a immaginare chi di noi non investirebbe visti quei risultati, che adesso saranno garantiti anche dallo Stato. È difficile perderci in un'operazione che garantisce un'elevata qualità Ma il fatto stesso che è lo Stato ad assumersi l'impegno di far funzionare nel migliore dei modi una concessione autostradale è già un buon investimento; non bisogna pensare soltanto alla remunerazione del capitale che, nel momento nel momento della quotazione in borsa, per quell'elevato livello di flottante che sarà in gioco, è nelle cose. Mi stupiscono alcune delle affermazioni fatte in quest'Assemblea, in cui non si riconosce il valore alto della collocazione sul mercato di azioni e quotazioni che riguardano un soggetto già di per sé remunerativo, ma garantito nella gestione dall'affidabilità e dalla credibilità dello Stato. Cassa depositi e prestiti (un soggetto disegnato in maniera molto negativa, nel cui statuto sono previste operazioni di questa natura quindi non è neanche un soggetto astruso a queste operazioni di mercato) farà certamente un intervento economico che sarà remunerato in un'infrastruttura in grado di funzionare anche grazie all'impegno dello Stato.

di un'operazione che garantisce tutti: non solo la prospettiva futura della concessione autostradale, ma anche tutti coloro che oggi hanno interessi economici nelle varie società di cui stiamo parlando e anche Atlantia. una garanzia che solo l'intervento dello Stato poteva dare. Tutto ciò è un valore di stabilità economica

Se tutto andrà nella direzione che auspichiamo, nella prossima primavera avremo questo nuovo soggetto che deterrà intorno al 30 per cento del capitale, qualificati investitori internazionali e un elevato flottante, al quale ho fatto riferimento, da parte di tanti investitori. La regia pubblica dell'operazione, l'assetto proprietario diverso, la sicura correttezza degli investimenti in sicurezza, il sistema di garanzia per gli utenti e la remuneratività degli investimenti sono valori che l'operazione garantirà e che saranno assunti certamente come buona gestione degli interessi degli italiani e - se permettete - anche dei loro soldi. Per questa ragione, il Gruppo Partito Democratico sosterrà

con un finale a sorpresa, tra l'altro: non si sa mai chi è l'assassino nei gialli o nelle *pièce* teatrali. Questa volta invece lo sappiamo: l'assassino è un pezzo della maggioranza e la vittima è l'altro pezzo. Anzi, vittime sono, come sempre, i cittadini italiani. In ambito politico, alla fine, bisogna anche semplificare per spiegare agli italiani quel che è successo. È evidente che la logica di statalizzazione del sistema produttivo è stato uno dei temi centrali della battaglia che, nel 1994, Forza Italia ha promosso nei confronti di quelle forze politiche che, fino al giorno prima, governavano il nostro Paese. La logica antistatalista

un'esclusiva funzione di controllo nell'ambito delle attività produttive, non una gestione in prima persona. Lo Stato deve essere l'elemento di garanzia; certamente può avere una partecipazione, ma la gestione e il controllo delle imprese devono essere affidati a chi fa impresa, quindi al privato. Lo Stato può esserne parte; può essere un elemento di garanzia, ma è il privato che deve opportunamente gestire il sistema produttivo del Paese. Da lì, Da lì, tutto quello che è accaduto nel passato, con la svendita dei gioielli di Stato oppure dei denti d'oro della nonna, come è accaduto dal signor Prodi

È evidente che quella non fu una privatizzazione; fu una regalia di imprese importanti che erano state assunte all'interno dell'Istituto di ricostruzione industriale, che aveva anche un senso quando fu realizzato. Aveva un fondamento; aveva una logica che in quel momento storico specifico funzionava.

crolla il ponte Morandi, decine e decine le vittime; tutti immediatamente pronti per responsabilizzare il gestore e, fermo restando che che la giustizia farà il suo corso, è evidente che è così. Tutti pronti per la revoca delle concessioni autostradali per giusta causa a un soggetto che le gestisce da decine di anni. Non solo. Qualche settimana fa, la Suprema corte dice che si è fatto bene a non affidargli la ricostruzione. Ho pensato

o, se li avessimo avuti, avremmo probabilmente vinto nuovamente per la revoca della concessione autostradale. Nel frattempo è successo

è lo *sponsor* storico di chi ha gestito le concessioni fino a ieri. L'ho detto simpaticamente al collega Cioffi anche poco fa.

3,4 miliardi di indennità per il crollo. ASPI deve pagare 3,4 miliardi e, nel frattempo, Cassa depositi e prestiti fa l'aumento di capitale di pari importo.

La logica delle concessioni autostradali deve essere necessariamente posta a salvaguardia, in quanto concessione e non regalo. La differenza fra regalo e concessione è sostanziale. La concessione si mette a gara;

i soldini dei libretti postali dei nostri concittadini e pensionati italiani non sarebbero stati buttati all'interno di un calderone che va a vantaggio esclusivamente di qualcuno e avremmo avuto la sicurezza

per ristoro e farli crescere del 25 per cento in una notte, a mercati aperti con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, riempiendo loro le tasche di soldi. Questa è una vergogna della quale siete responsabili e ancora una volta, cari cinquestelle, vi hanno buggerato. Sapete qual è la cosa più grave? Quelli buggerati sono gli italiani, che ancora una volta stanno a guardare la vostra incapacità di Governo. Noi voteremo contro

Presidente, gliene racconto una di ieri che ho vissuto personalmente: venendo giù da Milano per andare in Liguria il transito consigliato da Milano era andare a Torino e scendere giù dall'altra parte, perché non si poteva raggiungere Genova. Sto parlando di un'autostrada, la A26, che è il più importante collegamento fra la pianura Padana e ciò che sta oltre la pianura Padana, quindi la Mitteleuropa, la costa ligure, la Francia e la Spagna, perché il transito principale avviene attraverso quell'autostrada, che è impraticabile. La stessa cosa dicasi per la A10: i cancelli chiusi ormai da tanto tempo a ponente della città di Genova, da Genova aeroporto per arrivare fino ad Arenzano, impediscono il normale afflusso da ponente verso la città di Genova, cioè impediscono al porto di Genova di funzionare e alla città di Genova di ricevere quell'impulso turistico che aveva ricevuto in modo significativo negli ultimi anni. Siamo completamente a terra sotto tutti i punti di vista e i danni all'economia, al turismo, alla portualità e a ogni tipo di

ai turisti tedeschi e svizzeri che erano intenzionati a venire a Genova per visitare l'acquario, dove c'era scritto «per raggiungere Genova andare a Barcellona e prendere il traghetto». Era un cartello scherzoso,

quel quadro politico che ancora oggi è attuale. Mi riferisco a una sinistra che governava la città di Genova in alleanza con un partito dei Verdi,

Allora c'erano i verdi; oggi c'è qualcun altro. Devo però riconoscere al Partito Democratico un segnale di coerenza, una grande coerenza, dimostrata in tutti gli anni in cui le sinistre hanno amministrato la città di Genova e che è stata dimostrata nei dieci anni dell'amministrazione di sinistra Burlando della Regione Liguria: un totale congelamento; non si fa nulla; non si poteva dare una picconata da nessuna parte, perché se si va nella direzione di far crescere quella Regione, si va a rompere le scatole non si capisce bene a cosa o a chi. Ancora oggi

neanche. Guardate, oggi è anche la giornata giusta per discutere di questi temi. Questa mattina, signor Sottosegretario, il suo Ministro delle infrastrutture è a Genova e non è stato accolto tanto bene, non dalla politica, non da iniziative di partiti di centrodestra, della Lega o quant'altro. È stato accolto da manifestazioni spontanee tese a rimandarlo indietro, perché è una vergogna l'atteggiamento del Governo rispetto a scelte che devono essere fatte, ma che non arrivano mai. Genova oggi è ulteriormente bloccata per iniziative spontanee causate dalla presenza a Genova di un Ministro

in questo anno e più, per la ricostruzione del ponte. Io non finirò mai di ringraziare l'allora vice ministro Rixi, così come il Presidente della Regione e il commissario per quanto hanno fatto per la città, perché hanno sì avuto gli strumenti messi a disposizione a livello nazionale, ma hanno avuto il coraggio e la capacità di battere i pugni sul tavolo e di fare delle scelte.

Il modello Genova, quello che voi volete smontare bloccando ogni tipo di opera, è il modello dello sviluppo, della Gronda subito perché si può fare; è il modello del fare e del del no alla eccessiva burocrazia; è il modello della revisione del codice degli appalti. Questa è la riflessione

a raccogliere le macerie, per come è stato grande il fallimento delle sinistre a livello regionale e comunale. Mi avvio a concludere la mia dichiarazione di voto. Il Gruppo della Lega voterà a favore delle mozioni del centrodestra, quindi della nostra mozione, di quella di Fratelli d'Italia e di quella di Forza Italia. Ci dispiace, e lo dico con le braccia aperte, che il Gruppo di Italia Viva, che aveva presentato una mozione il cui dispositivo prevedeva di partire con i lavori della Gronda, abbia ritirato la mozione. Ancora una volta una vergognosa manovra all'interno della maggioranza, dove si ritira quello che si pensa pur di rimanere attaccati al carro, ad un Governo, ad una poltrona. *(Applausi)*. E sulla base di quella poltrona si sacrifica anche un'opera importante come la Gronda. Voteremo contro la mozione del Partito Democratico e dei 5 Stelle

che la Liguria è vissuta da questo Governo un po' come il margine dell'impero Conte, come il confine estremo. Abbiamo parlato in tre del Gruppo della Lega, tre liguri. Della maggioranza nessun ligure ha firmato una mozione e nessuno è intervenuto in quest'Aula. Forse perché i liguri di maggioranza si vergognano di cosa sta facendo questo Governo, di come si sta contrattando. Non sono neanche in Aula mentre stiamo parlando di questo tema. Ma con quale coraggio, poi, avranno la capacità o la volontà di presentare...

il calore di tutte queste dichiarazioni, vorrei ricordare a me stesso, perché l'Aula sicuramente ne è edotta, che mi sembra che De Gasperi sia morto. Mi sembra che sia morto anche Einaudi, se non ricordo male, quell'Einaudi che diceva che prima di deliberare bisogna conoscere, quindi prima di parlare bisognerebbe studiare, approfondire e sapere, quando si parla, di cosa si parla. quando si parla in questo modo bisognerebbe ricordare tante cose. Ne potremmo dire tante ma per iniziare vorremmo ricordare, per esempio, che nel 2008 le concessioni autostradali

fu detto che nella convenzione si inserivano gli articoli 9 e 9-*bis*, quel famoso articolo che prevedeva questa grande dilatazione dei compensi in caso di revoca,

Ma guardate un poco com'è strano il mondo, come sono strane le cose che succedono. E perché tante cose succedono? Prima ho sentito il senatore Mallegni parlare di

se si generano utili così elevati - perché sono utili enormi quelli previsti dalla concessione - è giusto che li incameri un privato o è giusto che vengano redistribuiti tramite il pubblico? Questo è il tema. Sono d'accordo - lo dice anche la nostra Costituzione - sul fatto che l'iniziativa privata è libera, ma il tema è quanto può e deve lucrare un privato.

249 miliardi, sono arrivate a 270 miliardi. Quindi raddoppiano i ricavi, le manutenzioni sono piatte e il costo del lavoro diminuisce. Che cosa significa tutto questo? Significa che quella concessione era un abominio. allora che deve intervenire lo Stato. Lo Stato deve essere forte, deve avere il coraggio di affermare la supremazia dei cittadini e degli utenti nei confronti di qualsiasi società privata che fa il suo interesse, quando l'interesse è troppo elevato. Nessuno dice che il privato non debba avere un utile, ci mancherebbe altro, ma, quando gli utili sono così stratosferici, c'è una sola possibilità, vale a dire che gli utili stratosferici li incameri il pubblico per redistribuirli,

Questo dovete dire a voi stessi, ne cito una sola. L'Agenzia del demanio è stata portata come eccellenza in Europa per lo sdoganamento direttamente a bordo: siamo più bravi. Sì, siamo i più bravi, possiamo insegnare al mondo queste cose e questo lo fa lo Stato, perché l'Agenzia del demanio è lo Stato. Vogliamo parlare delle privatizzazioni di quell'epoca? Vogliamo ricordarci che cosa è stato fatto con Telecom, quando Telecom è stata acquisita a debito due volte? Oggi Telecom ha 25 miliardi di euro di debiti.

possiamo tranquillamente parlare, e cominciata dalla relazione della Corte dei conti. Penso che della Corte dei conti, come al solito, ci dovremmo fidare, quando ci dice (leggo testualmente): «Anac ha rilevato che la spesa per manutenzioni rappresenta una bassa percentuale. Infatti, ammonta al 2,2 per cento di quella prevista dal piano economico-finanziario».

medesimi motivi la Sezione di controllo della Corte dei conti, nel 1997, ebbe a dichiarare illegittimo l'affidamento della più importante concessione». Quell'affidamento fu illegittimo e ci volle una legge per sanare quell'illegittimità. *(Applausi)*. È questo il tema di cui stiamo parlando oggi. Chi l'ha fatto? L'ha fatto Prodi? Quella cosa era illegittima, ragazzi; se non si faceva la legge, tutto questo non sarebbe successo. *(Commenti)*.

quell'opera portata avanti per lotti funzionali con l'avvio immediato del raddoppio dell'A7. Stiamo parlando del modo di fare - sì - la gronda, ma di farla bene. Questa è la differenza, caro Presidente. Dopo tanti anni sentiamo ancora oggi parlare di fare le cose come si diceva

la legge Galli del 1994, stabiliva che la gestione deve essere efficiente, efficace ed economica - questo diceva la legge, utilizzando tre parole importanti e corrette - noi dobbiamo fare in modo che, quando spendiamo i soldi, lo facciamo massimizzando l'efficienza. Questo significa aver rimesso mano alle analisi costi-benefici. *(Applausi)*. Molti di quelli che sono qua dentro e sono stati al Governo se ne sono dimenticati. Allora noi cosa abbiamo fatto? Semplicemente abbiamo rimesso mano, abbiamo fatto le verifiche e cerchiamo di accelerare la spesa. Questo è quanto stiamo facendo: niente di più e niente di meno. Quando diciamo che lo Stato rientra in ASPI, con l'aumento di capitale, sarebbe molto interessante capire le fluttuazioni azionarie di cui parlava il senatore Mallegni - mi avvio alla conclusione, signor Presidente - che sono ovviamente figlie della speculazione finanziaria: quella speculazione finanziaria che uccide le imprese, i mercati e il Paese. E noi forse la dobbiamo contrastare. Abbiamo la forza di contrastare la speculazione finanziaria? I Benetton hanno visto il loro valore azionario scendere da 28 euro ad

noi abbiamo il coraggio di rimettere mano alle cose; pensiamo che lo Stato possa essere forte; pensiamo che lo Stato possa gestire le infrastrutture in maniera neutra, come già avviene per esempio per Terna e per Snam (per fare due esempi importanti di questo Paese. E pensiamo che le infrastrutture fondamentali di questo Paese debbano essere nelle mani pubbliche, e parleremo anche delle infrastrutture in fibra ottica. Questo è l'obiettivo che noi abbiamo: avere una visione in cui lo Stato è forte e il privato, su quella forza, può fare tutto la concorrenza che vuole, ma mai a scapito dei cittadini. finestra"). Si sono così concluse le dichiarazioni di voto. Prima di passare alle votazioni avverto che, in linea con una prassi ormai consolidata, le mozioni saranno poste ai voti... *(Commenti)* Sto leggendo un annuncio.

Signor Presidente, colleghi, la mozione che ci apprestiamo ad esaminare è di grande importanza per la salute degli italiani, invita il Governo ad adottare ulteriori misure di precauzione sul glifosato: una molecola molto conosciuta, un diserbante introdotto sul mercato a partire dal 1974 ad opera della Monsanto, un'azienda multinazionale di biotecnologie agrarie che ne ha scoperto l'azione come erbicida ad ampio spettro. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro nel 2015 ha classificato, però, il glifosato come un probabile cancerogeno per l'uomo e, come tale, lo ha inserito in un gruppo di 66 sostanze a rischio che possono agire anche come interferenti endocrini. Le evidenze scientifiche attestano altri rischi per la salute che consistono nell'alterazione della capacità riproduttiva, della permeabilità intestinale, nonché modificazioni metaboliche e delle funzioni del sistema nervoso. tratta di una sostanza nociva che fa male, specie a neonati e bambini. Il nostro Paese non ha quindi bisogno di alcuna rivisitazione circa l'utilizzo del glifosato, come propone qualcuno. Ieri si è chiaramente pronunciato anche il mondo medico-scientifico attraverso Recenti studi dell'Istituto Ramazzini hanno messo in evidenza che il glifosato e il suo formulato Roundup procurano la formazione di micronuclei, e cioè genotossicità; hanno effetto androgenico e determinano l'aumento del testosterone nel sangue sia dei maschi che delle femmine, causando un'alterazione anche del microbiota intestinale durante le prime fasi della vita. Mi sorprende che alcuni colleghi non siano a conoscenza di questi studi.

ha dovuto patteggiare con oltre 10 miliardi di dollari per chiudere 95.000 cause legali intentate per seri danni alla salute correlati all'uso dell'erbicida. Oltre il 97 per cento dei prodotti alimentari commercializzati nel nostro continente contiene residui di glifosato. Sono state trovate tracce nelle urine di 48 europarlamentari, nel latte materno, nel miele, nella birra e perfino nei vaccini. Il glifosato viene ampiamente usato in pre-raccolta negli Stati Uniti e in Canada nelle coltivazioni di grano duro per favorirne la maturazione artificiale, controllare il momento del raccolto e ottimizzare la trebbiatura, con conseguente presenza di residui nel grano raccolto e nelle semole che ne derivano. Al contrario, tale uso in Europa e in Italia non rientra nelle buone pratiche agricole. Eppure, l'Italia importa grano duro dagli Stati Uniti e dal Canada per la miscelazione e produzione di semola, pasta, pane e altri prodotti da forno contengono residui di glifosato. Gli accordi di libero scambio evidentemente vorrebbero imporre ai consumatori italiani, che sono i maggiori consumatori al mondo di derivati dei cereali, i residui di questi pesticidi in violazione del principio di precauzione. Il sottoscritto, per aver asserito con le analisi che la presenza di questo marcatore fosse un indizio di miscelazione tra grani esteri contaminati e grani nazionali privi di glifosato, ha dovuto subire vari giudizi per diffamazione in sede sia civile che penale, tutti sinora conclusisi - per fortuna - favorevolmente. Diversi *test* effettuati dalle associazioni Granosalus e Salvagente su alcuni marchi di pasta e semola italiana hanno dimostrato la presenza del contaminante, sia pure entro i limiti di legge, anche se nel mercato comunitario e italiano le disposizioni prevedono che dall'agosto 2016 questa sostanza non possa essere somministrata in pre-raccolta nei campi di grano, introducendo così di fatto un divieto al suo uso (e dunque la disapplicazione dei limiti previsti dal regolamento UE 293/2013). Tale divieto paradossalmente non viene esteso alle navi di grano estero, che, pur presentando un livello di residui nei limiti previsti dal predetto regolamento - come conferma anche il monitoraggio predisposto dal Ministero della salute continua ad approdare indisturbato ai porti italiani, generando peraltro una restrizione della concorrenza al prodotto italiano non contaminato, dunque più pregiato e ricercato. Del resto, i controlli effettuati dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (Icqrf) e dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) sulle navi ormeggiate al porto di Bari, ma anche negli altri porti italiani, dimostrano che le analisi sono numericamente ridotte; prevale un controllo documentale rispetto a quello analitico; i laboratori spesso non sono accreditati; le analisi non sono visibili a noi parlamentari, che pure le abbiamo chieste in Commissione agricoltura, e viene campionato solo il 5 o 6 per cento delle navi, mentre durante il periodo Covid non vi sono state attività di controllo. Nonostante sia ormai acclarato che il glifosato sia una sostanza pericolosa, la Commissione ha rinnovato per ulteriori cinque anni l'autorizzazione, che scade tra due; dopodiché, esaurite le scorte, speriamo diventi auspicabile uno *stop* definitivo all'uso di questa molecola. L'ultimo regolamento è stato oggetto anche di un ricorso proposto presso l'Unione europea da parte dell'associazione Granosalus, che svolge per statuto attività di vigilanza tesa a garantire la migliore qualità dei prodotti cerealicoli, anche sotto il profilo sanitario, a tutela dei produttori e dei consumatori. L'associazione ha contestato, da un lato, l'illegittimità del regolamento di esecuzione per violazione del principio di precauzione e per elusione delle disposizioni di procedura circa il rinnovo dell'approvazione della sostanza, che si è attestata su studi scientifici di dubbia provenienza non improntati ai principi di indipendenza, obiettività e trasparenza; e, dall'altro, la mancanza a monte nel regolamento stesso di approfondimenti istruttori circa l'incidenza dell'uso del glifosato sugli animali, sulle acque sotterranee e sui prodotti destinati al consumo umano, come il pane e l'acqua. A livello nazionale, il Ministero della salute non ha introdotto ulteriori misure di natura precauzionale a sospendere gli effetti del comunicato del Ministero della salute del dicembre 2017, con cui si è recepito il rinnovo della sostanza glifosato per cinque anni; a prevedere che i grani esteri, provenienti da aree dove il clima impone l'impiego di glifosato, siano assoggettati al principio di precauzione comunitario previsto dal regolamento (UE) n. 1.313 del 2016, così come recepito dal decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016, ma mai applicato con circolari chiare dai dirigenti nazionali nei confronti degli uffici periferici USMAF; ad emanare una circolare che vieti la presenza di glifosato in tutte le stive di grano importato, anche se viene sdoganato in altri porti europei, e disporre, di conseguenza, l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio attraverso il prelievo di campioni da ciascuna stiva per affidarli a laboratori accreditati e rendendo noti gli esiti delle analisi, con riferimento anche al traffico commerciale e alle connesse operazioni in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della Puglia dove sbarca la maggior parte delle navi contenenti grano duro proveniente dal Canada e dagli Stati Uniti; tutto ciò con lo scopo di garantire sicurezza alimentare, ambientale e sanitaria. il Governo a promuovere, anche mediante lo strumento della decretazione di urgenza, degli interventi normativi finalizzati a vietare l'utilizzo e la presenza della sostanza negli alimenti, oltre che a scoraggiare l'acquisto e l'utilizzo di grani esteri che vengono miscelati con il grano duro nazionale di ottima qualità, falsando le quotazioni del mercato italiano, come ha dimostrato anche una sentenza del TAR Puglia nel 2019. Infine, si intende impegnare il Governo ad adottare tutte le necessarie misure di precauzione sul territorio nazionale volte a proteggere la sanità pubblica, nonché la salubrità dell'ambiente con specifico riferimento alla tutela delle acque, della flora e della fauna.

attenzione dopo aver ringraziato i senatori sottoscrittori che hanno acconsentito al deposito: la Capogruppo, senatrice Unterberger, e i colleghi che hanno aggiunto la loro firma. Il mio auspicio, con la mozione in oggetto, è che in quest'Assemblea e nell'intero Parlamento, nel dialogo con il Governo, si possa instaurare, proprio partendo dall'argomento di oggi, una nuova prassi che promuova la necessità di avvalersi delle evidenze scientifiche come base di partenza delle discussioni politiche, in particolare di quelle molto tecniche che riguardano la salute. il dovere di chiedere semplicemente a voi questo impegno, al di là di ogni schieramento, investendo il Governo di questa nuova modalità e del nuovo metodo, proprio nell'interesse di tutti. Partire dalle evidenze e prove, potendo definire il loro grado di certezza, significa muovere da premesse neutre, sulla base delle quali, poi, ovviamente, deliberare. Mi riserverò magari dopo, nel corso della discussione, di scendere in alcuni dettagli tecnici. L'oggetto in discussione oggi - il glifosato - mi sembra davvero il giusto terreno per chiederci come possiamo discutere razionalmente di un tema che è importante e molto tecnico e complesso, mi viene da dire anche molto affascinante culturalmente, perché contiene molto dei nostri rapporti con il mondo ed è quindi anche molto conflittuale. La domanda è pertanto la seguente: da dove partiamo per discutere razionalmente? L'oggetto di oggi è il glifosato, un analogo della glicina, uno dei 20 amminoacidi di cui siamo composti, caratteristiche interessanti. È un erbicida poco costoso, che ha davvero cambiato lo scenario agricolo negli ultimi viene usato non solo nell'imprenditoria agricola per rimuovere le malerbe; pensiamo anche ai Comuni e agli enti deputati a pulire ferrovie e strade che lo utilizzano proprio per rimuovere le erbe

velocemente, avendo una bassa penetrazione nel suolo - se volete, ci addentriamo nelle questioni tecniche - e soprattutto presenta una bassissima tossicità nei mammiferi, perché agisce su un enzima presente solo nelle piante - noi quell'enzima non lo abbiamo - e non ha alcun bersaglio molecolare nell'uomo. ha una lunga storia: scoperto nel 1950, riscoperto nel 1970, brevettato da Monsanto, utilizzato sulla soia geneticamente modificata, e forse l'avversione a questo erbicida nasce da lì, ma lasciamo questi aspetti tecnici a parte. Il punto cruciale è che dal 2001 il brevetto è scaduto quindi, è di libero impiego e ci sono 350 aziende nel mondo che lo producono. Se questo è l'oggetto, come possiamo essere sicuri che non causi danni all'uomo? Ci sono organi e organismi tecnici in Europa e nel mondo che ci aiutano a capire questo? Come su ogni altro fitofarmaco usato in agricoltura, agricoltura, i fitofarmaci hanno *dossier* enormi, sono tra le molecole più studiate, persino più dei farmaci; quindi, come possiamo decidere? Questi organismi ci danno informazioni, studiano tutti i *dossier*, preparano e raccolgono raccolgono le varie informazioni. Pensate che questi organismi sono tanti, e la stragrande maggioranza valuta

allora, di prestare un attimo di attenzione alla differenza tra pericolo e rischio perché, se non ci capiamo qui, rischiamo di prendere degli abbagli. Non sono sinonimi. Il pericolo è la potenzialità astratta di un prodotto di causare un effetto tossico indesiderato nell'uomo. Questo è il pericolo. Il rischio, invece, è una misura effettiva delle conseguenze che tale sostanza può in funzione delle dosi a cui è somministrata e dei tempi di esposizione. Se prescindiamo da dosi e tempi, abbiamo sbagliato strada, e vorrei farvi un esempio sulla differenza tra pericolo e rischio. Penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che una lama lunga e affilata sia pericolosa - giusto? - ma nessuno di noi si sentirebbe a rischio entrando in un supermercato e andando a comprare coltelli o usando il coltello per pulire la verdura. Allo stesso modo, il fuoco è pericoloso, ma nessuno pensa di accendini e fiammiferi. L'acqua, colleghi, è pericolosissima, a parte il rischio di annegamento: pensate che, bevendone sei litri in poche ore, si può mettere a rischio la propria vita; berne un paio di litri al giorno non solo è sicuro e non rischioso, ma è anche molto consigliabile, soprattutto in questo periodo dell'anno. Quindi, nel valutare divieti o autorizzazioni, il rischio è il parametro a cui guardare, perché dà una misura quantitativa delle conseguenze negative per l'uomo. Quelle 20 agenzie, tra cui lo IARC - ciascuno fa il suo lavoro - come hanno valutato il glifosato? Come ho detto, lo IARC è una branca dell'OMS, fa valutazioni solo di pericolo e, quindi, è il potenziale astratto, e non di rischio; lo dice anche nel preambolo della monografia dedicata proprio al glifosato, la sostanza di cui discutiamo oggi. E poi, come per ogni altra sostanza - una volta che ha concluso la sua disamina del pericolo di una sostanza lo IARC classifica le sostanze in categoria 1 (sicuramente cancerogeno; lo IARC valuta la cancerogenicità). Cosa troviamo in categoria 1? bevande alcoliche, insaccati, carne lavorata e, quindi, i salumi tipici della tradizione gastronomica italiana, che sono sicuramente cancerogeni secondo lo IARC, che valuta il potenziale, a prescindere da dosi

nella categoria 2A ci sono il lavoro notturno, le bevande calde (incluso il mate argentino), i vapori delle tinture per i capelli, i fumi delle fritture, e via dicendo. Faccio notare che, negli anni in cui sono in Senato, non ho mai visto presentare un atto di indirizzo che proibisce il consumo di salumi o il lavoro notturno. C'è questa classificazione dello IARC. Cosa dicono le altre agenzie?

di fronte a una situazione per cui non esiste un'agenzia sanitaria al mondo che abbia stabilito

ma una società impaurita e fragile è preda di tentazioni difensive. Ecco perché chiedo un approccio metodologico. chiede di non assecondare nessun punto di vista, nessuna paura, nessuno dei nostri istinti e nessuna posizione preconcetta, ma semplicemente impegna il Governo ad acquisire i dati, le prove e gli studi più aggiornati affinché ogni decisione possa partire su base scientificamente solida. Poi ci saranno la decisione politica e la supremazia della decisione politica. Una politica basata sull'evidenza sarebbe sempre necessaria, ma davvero credo lo sia ancora di più quando il legislatore è chiamato - come in questo caso - a scelte ad alto grado di tecnicalità. Sono decisioni che hanno un forte impatto su molti settori vitali della nostra economia. Pensiamo al comparto agricolo ed è davvero importante, soprattutto nell'interesse dei cittadini, che decisioni del genere vengano prese su basi scientifiche solide. *(Applausi).*

Presidente, onorevoli colleghi, se chiudiamo gli occhi ci sembra di vedere le spighe ondeggianti illuminate dal sole per la ricchezza del contenuto che custodiscono e nella mitologia sono simbolo di fertilità. Nelle immense distese dei campi il colore è quello dell'oro e sono preziose come l'oro. Sto parlando del grano, germoglio simbolo di rinascita e senso della vita stessa. Il grano italiano è l'emblema della salubrità, fulcro della nostra alimentazione e alla base di quella dieta mediterranea che - non a caso - è patrimonio dell'UNESCO. economic and trade agreement (CETA) tra l'UE e il Canada ha più che quintuplicato l'esportazione in Italia di grano duro e un chicco su tre che arriva dall'estero sulle nostre tavole è canadese. Sui campi gelidi del Canada non risplende il sole come da noi e il grano viene trattato

come un analogo della glicina e può alterare una serie di proteine; ciò può portare all'insorgere di diverse patologie. Le principali, elencate in uno studio condotto da Anthony Samsel e Stephanie Seneff e confermate dal MIT, sono diabete, obesità, asma, morbo di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica morbo di Alzheimer e tante altre che sono già state enunciate da chi mi ha preceduto. Non solo: quel pesticida viene assorbito per via fogliare, successivamente traslocato in ogni altra posizione della pianta, quindi ai frutti; ha una solubilità in acqua di 10,1 grammi per litro a 20 gradi e ciò significa che alle temperature di cottura dei cibi, ben superiore a 20 gradi, passa facilmente nella catena negli animali e quindi nelle persone. Con prodotti invasi dal glifosato mi chiedo che fine potrebbe fare nel tempo l'eccellenza alimentare del *made in Italy* e tutto questo che ricaduta potrebbe avere sul sistema economico Ecco perché chiediamo il divieto di utilizzo di tale diserbante e diciamo convintamente «no» al glifosato. Da tempo se ne denuncia la pericolosità; la cosa ovviamente preoccupa me e tanti altri come me. Provengo da una terra, la Campania, dove i prodotti a base di farina di grano duro sono parte parte del nostro DNA. La nostra storia e cultura gastronomica sono profondamente permeati da questi alimenti, contribuendo a rendere la mia Regione e più in generale la cucina italiana la più apprezzata nel mondo. Chi di voi, onorevoli colleghi, non ha mai goduto delle gioie di un bel piatto di pasta di Gragnano della mia Benevento? Ecco, la tutela di questa eccellenze

come vi illustrerò di seguito. Questa mozione si è resa necessaria affinché si sospendano subito gli effetti del comunicato del Ministero della salute del 19 dicembre 2017, con cui si è recepito il rinnovo della sostanza attiva glifosato per cinque e si è assunta ogni idonea iniziativa in sede europea per promuovere la revisione delle decisioni prese in merito all'utilizzo del glifosato per regolamento di esecuzione (UE) Il Ministero lo ha recepito con il decreto ministeriale 9 agosto 2016, recante misure restrittive precauzionali per gli usi della sostanza diserbante glifosato; in particolare, attraverso tale decreto è stato revocato l'impiego in pre-raccolta sul grano, al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura. Sta di fatto che il precedente regolamento (UE) n. 1305/2013 tollerava la presenza di glifosato,

deve oggi dimostrare con chiarezza se è a favore o contrario al principio di precauzione. Ciò che maggiormente spaventa è proprio l'approvazione dell'accordo di libero scambio tra Europa e il Canada. Come dicevo prima, nessuno nega l'importanza della politica degli accordi internazionali, che tanto beneficio portano alla bilancia commerciale nazionale, ma occorre una maggiore attenzione in sede di trattativa comunitaria per evitare che accadano queste situazioni. Il consumatore alimentare italiano è uno dei più esigenti e preparati nel panorama internazionale; ce lo dice la bibliografia universitaria e non possiamo tradire la sua fiducia introducendo elementi così

difesa della nostra salubrità. Comprendo che alla base ci siano gli interessi di grandi aziende, come per esempio la Monsanto e la Bayer, ma occorrono pene severe. Chiediamo e vogliamo controlli stretti, seri e rigorosi. da tempo stiamo trattando l'argomento e da diverse audizioni è emerso, a mio avviso, qualcosa di molto inquietante a proposito dei controlli: si fanno a campione - ed è giusto che sia così - ma non è accettabile che, se questi risultano essere per tre volte negativi, per il prosieguo si fa solo un controllo documentale sulla mera scorta di ciò dichiarano le aziende. Questo penso che sia assurdo; i controlli devono essere fatti sì a campione, ma tutte le aziende devono sapere che da un momento all'altro possono essere verificati i loro imbarchi di merce. Non possiamo accettare che le navi arrivino liberamente nei nostri porti; le leggi ci sono? Vanno rispettate. Non ci sono? Vanno fatte.

impegna il Governo: 1) a sospendere gli effetti del comunicato del Ministero della salute del 19 dicembre 2017 con cui si è recepito il rinnovo della sostanza attiva glifosato per 5 anni e ad assumere ogni idonea iniziativa in sede europea per promuovere la revisione delle decisioni assunte in merito all'utilizzo del glifosato con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324

normativi finalizzati a vietare l'utilizzo e la presenza della sostanza attiva glifosato negli alimenti; 5)

del 15 dicembre 2017, con il rinnovo del suo utilizzo per 5 anni, per cui la sostanza è oggi in commercio in tutti i Paesi dell'Unione europea; il sistema europeo di autorizzazione e di controllo degli agrofarmaci è il più stringente al mondo, pertanto, se un fitofarmaco è regolarmente in commercio nell'Unione europea, vuol dire che dal sistema di analisi europeo non è emerso alcun elemento concreto che ne giustifichi la messa al bando; i controlli effettuati dall'EFSA a livello comunitario su 48.000 campioni indicano che il 97,2 per cento dei prodotti alimentari analizzati (valore che sale al 98,6 per cento per l'Italia) presenta valori dei residui al di sotto delle soglie di legge e, pertanto, sono da ritenersi sicuri per il consumatore; l'Italia dispone di una legislazione molto restrittiva circa l'autorizzazione e l'impiego dei fitofarmaci, caratterizzata soprattutto da norme che ne impongono l'uso limitato a quanto strettamente necessario per garantire la sicurezza alimentare ed elevati *standard* quantitativi e qualitativi e qualitativi delle produzioni agroalimentari; il decreto 9 agosto 2016 del Ministero della salute, in linea con le decisioni europee (regolamento di esecuzione n. 2016/1313 del 1° agosto 2016), ha modificato le condizioni di impiego della sostanza glifosato; attualmente le limitazioni riguardano: a) l'uso non agricolo su suoli che presentano una percentuale di sabbia superiore all'80 per cento nelle aree vulnerabili e nelle zone di rispetto; b) l'uso nelle aree frequentate dalla popolazione quali parchi, giardini, campi sportivi ed aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie; c) l'uso in pre-raccolta al solo fine di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura; competente al fine dei controlli sull'immissione in commercio e sull'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, è anche il dipartimento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'Ispettorato svolge in particolare i controlli sulle importazioni di prodotti dai Paesi terzi, monitorando l'arrivo delle navi nei porti e svolgendo direttamente le analisi su circa 300 principi attivi. Nel 2019 sono stati svolti circa 2.000 controlli sui cereali, con 1.785 operatori controllati, rilevando un tasso di irregolarità sui prodotti dell'8,7 per cento dovuto in primo luogo ad errate etichettature; l'entrata in vigore delle limitazioni all'uso del glifosato, attuate in Italia con il citato decreto ministeriale del 9 agosto 2016, non ha portato alla disapplicazione dei limiti vigenti, bensì a limitare l'impiego del glifosato nelle coltivazioni nazionali; i dati a disposizione del Ministero della salute evidenziano che dai controlli condotti dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), nell'ambito di un piano di campionamento conoscitivo disposto dal medesimo Ministero per la ricerca del glifosato, tutti i campioni analizzati presentano

gli orientamenti degli Stati europei in merito all'impiego del glifosato nella fase immediatamente successiva alla data del 2022, che coincide con la scadenza del permesso di 5 anni, non sono uniformi; la stessa Commissione europea ha designato 4 Stati membri (Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Svezia) come correlatori della valutazione dell'uso del glifosato, che dovranno presentare entro il mese di giugno 2021 un rapporto di valutazione ai fini del rinnovo all'EFSA, per l'espressione da parte di quest'ultima del parere scientifico; si segue quindi un principio di precauzione; dopo la scelta dell'Austria di non vietare l'uso dell'erbicida, il Lussemburgo ha deciso di bandirlo già dal 2021. In Francia, nonostante un investimento pubblico da 400 milioni di euro, il piano, denominato "Ecophyto", che mira a ridurre del 50 per cento i fitofarmaci in agricoltura entro il 2025, non è ancora partito. Anzi, dal lancio del piano nel 2008, l'uso dei fitofarmaci è aumentato del 12 per cento, secondo i dati presentati dalla Corte dei conti al Governo francese. Dopo una lieve diminuzione nel 2017, le vendite sono salite del 10 per cento per i soli prodotti a base di glifosato; le diverse posizioni assunte dai Paesi membri riflettono la mancanza di un giudizio univoco da parte del mondo scientifico sui rischi per la salute pubblica legati all'impiego del glifosato; le analisi adottate dalle autorità di controllo competenti sulle prove disponibili hanno prodotto una netta spaccatura di pareri in merito all'eventuale nocività dell'erbicida, scatenando un acceso dibattito sulla chiarezza degli stessi metodi di ricerca utilizzati, tanto da spingere la stessa Unione europea a varare un nuovo regolamento per aumentare la trasparenza dei *test* scientifici dell'EFSA; lo scorso gennaio 2020, l'Environmental protection agency statunitense (EPA), nella sua "Interim registration review decision", ovvero nell'ulteriore valutazione del rischio, concluso il suo parere scientifico affermando che non vi sono motivi di preoccupazione quanto a rischi di tipo alimentare per alcun segmento della popolazione, neanche seguendo le ipotesi più prudenziali applicate nelle valutazioni (ad esempio: residui al massimo livello di tollerabilità, applicazione diretta dell'acqua e trattamenti sul 100 per cento delle colture); l'Agenzia ha quindi concluso il rapporto dichiarando che non sussistono rischi né di tipo professionale né per gli astanti non occupazionali; oltre all'EFSA, anche l'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) ha concluso che la molecola è sicura; è opportuno tuttavia considerare che, in generale, molecole e principi attivi vanno sempre utilizzati con metodo e moderazione e l'utilizzo del glifosato è, ad oggi, necessario in agricoltura su svariate colture colture per ottenere buoni risultati, tenendo conto che normalmente per ogni ettaro coltivato si diserba solo il 20 per cento e che la sostanza può essere irrorata solo quando effettivamente indispensabile; inoltre le modalità di utilizzo a livello dell'Unione europea del glifosato sono diverse rispetto a Paesi terzi quali USA, Canada e Turchia, e di gran lunga favoriscono una maggior salvaguardia e tutela dell'ecosistema, degli stessi operatori e dei consumatori; nondimeno è indispensabile, alla luce del clima di assoluta incertezza rispetto ai futuri orientamenti che verranno adottati dall'Unione europea in merito all'uso dei fitofarmaci, che il nostro Paese predisponga fin da subito un quadro di azioni per l'impiego sostenibile della chimica e lo sviluppo di tecniche di agricoltura integrata ed alternative a quelle tradizionali; negli anni più recenti, la disponibilità di nuove molecole ad impatto ambientale sempre più ridotto ed attive a dosi sempre più basse ha creato le condizioni favorevoli al raggiungimento di elevati livelli di sicurezza alimentare e di protezione dell'ambiente, tanto che in Italia, grazie all'impiego di sistemi innovativi di difesa delle colture, l'utilizzo dei fitofarmaci è diminuito ad un ritmo dell'1,8 per cento annuo negli ultimi 10 anni. Oltre il 70 per cento dei prodotti rientra, infatti, tra quelli meno impattanti, e meno del 4 per cento tra quelli classificati come tossici; la riduzione dei quantitativi di fitofarmaci utilizzati in agricoltura evidenzia come già da tempo il comparto agricolo italiano si sia orientato verso un sistema di produzione integrato, in grado di coniugare le esigenze economiche del mondo agricolo con quelle ambientali e sanitarie, per lo sviluppo di un'agricoltura maggiormente sostenibile e competitiva; accanto ai principi attivi di origine chimica ovvero di sintesi, si stanno sviluppando stanno sviluppando studi sulle sostanze di origine naturale aventi effetto erbicida derivate dalle piante officinali, come ad esempio i prodotti a base di acido pelargonico attualmente in commercio scopo, impegna il Governo: 1) a sostenere iniziative volte ad un utilizzo più responsabile dei fitofarmaci in agricoltura permettendo al comparto di continuare a crescere e svilupparsi secondo un approccio fondato sull'uso coordinato e razionale ed ecocompatibile di tutti i fattori produttivi,

utile iniziativa finalizzata alla promozione di programmi di ricerca e a predisporre un piano nazionale sementiero che permetta, da una parte, di investire su colture quali leguminose, frutta in guscio e, soprattutto, frumento duro e tenero, che negli ultimi anni hanno perso superfici coltivate a favore di un forte aumento delle importazioni da Paesi terzi, e, dall'altra, sostenerne il prezzo sui mercati favorendo la coltivazione nelle zone storicamente vocate del Sud Italia. *(Applausi)*.

Signor Presidente, parliamo di glifosato dalla scorsa legislatura. Il glifosato è un erbicida sistemico messo a punto agli inizi degli anni la dichiarazione della sua completa innocuità è stata causa del suo abuso. È stato usato in maniera eccessiva nel corso dei decenni scorsi, nell'ottica di un'agricoltura intensiva

e alle basi scientifiche attorno ad esso, ma bisogna inserirlo in un sistema agricolo che è stato devastante. Il glifosato è stato usato in passato in contesti di grande pericolosità ambientale: pensiamo alla soia transgenica, che non pericolosa perché transgenica, ma perché resistente al Roundup, per cui la modalità di coltivazione della soia transgenica è stata quella delle grandi distese in Sud America, con gli aerei che irroravano glifosato su su centinaia di ettari, andando a caricare quindi il sistema ambientale con quantità di prodotto chimico, che non è mai a rischio zero, perché non esiste la chimica a rischio zero.

forse no. In realtà, quando non si hanno abbastanza conoscenze per arrivare a una certezza, vuol dire che la scienza non ha una risposta definitiva. Nel caso del glifosato è così: se lo IARC ci dice che c'è un pericolo un pericolo di carcinogenicità, vuol dire che esiste un pericolo e noi, come politici, non possiamo dire che quello scienziato ha ragione e quell'altro ha torto, ma dobbiamo prendere atto delle evidenze attuali e dire che esiste una potenzialità di tossicità del glifosato all'interno del grano. Veniamo al grano: per quale motivo noi italiani dobbiamo importare un grano seccato con il glifosato anziché potenziare i nostri grani antichi e la nostra produzione di grano?

la pasta, il pane e così via. Attenzione alle soglie di tossicità, che devono essere calibrate sia sull'età in cui si somministra il prodotto alimentare, sia sulle usanze alimentari del nostro Paese, che sicuramente fa un uso di pasta molto superiore rispetto ad altri Paesi europei. La seconda questione riguarda l'accumulo nella catena alimentare. Non dimentichiamoci che noi diamo grano o comunque prodotti derivati dal grano ai nostri animali; e la scienza sa che, mano a mano che si sale nella catena alimentare, i prodotti tossici vengono metabolizzati e accumulati. Quindi facciamo attenzione quando parliamo di pericolo, perché il pericolo di un coltello al supermercato lo posso affrontare: lo vedo nello scaffale, lo compro e sto attenta. Non posso invece affrontare il pericolo del glifosato nel grano, perché in etichetta non c'è scritto quanto ce n'è; quindi potrei dare al mio bambino chili di glifosato senza saperlo. Attenzione a parlare di scienza, laddove la scienza non c'entra proprio niente. Ben venga una meditazione sul glifosato nel cibo. diversa è dire che dobbiamo diserbare i binari dei treni, altrimenti il treno deraglia. Cerchiamo di distinguere le questioni: una cosa è il glifosato negli alimenti, una cosa diversa è il glifosato dato da mangiare agli animali e una cosa ancora diversa è la questione ambientale

qualche numero per capire di cosa stiamo parlando. Alcune cose sono già state dette, ma vanno sempre precisate per capire esattamente le dimensioni del fenomeno. Il giro d'affari del glifosato nel mondo è di 4,24 miliardi di dollari; questo dato viene dal gruppo di studio sull'impatto e sulle prospettive del glifosato. Sette delle più grandi aziende produttrici mondiali di glifosato sono cinesi; questa è una fortuna, perché la Cina assorbe quasi interamente la produzione di glifosato per uso interno. L'ottava è la Bayer, solo perché si è comprata la Monsanto. è che in Italia si usa mezzo chilo di glifosato per ogni ettaro, non nella sua formulazione base, ma in quella additivata, nota commercialmente per esempio come Roundup, che era il nome commerciale con cui nasceva questo prodotto. Le ferrovie italiane sono grandi utilizzatrici di glifosato; non ho trovato il dato, ma lo mutuo da quello francese della Société nationale des chemins de fer, che ne usa 1,1 chili per chilometro. Supponendo che anche gli italiani facciano lo stesso, per non essere da meno, sono 18 tonnellate solamente per il diserbo, che potrebbe essere fatto in modo termico, per esempio, ma che invece si sceglie di fare in modo chimico, perché sicuramente è meno costoso. Per quanto riguarda invece l'evoluzione della normativa inerente agli studi che sono stati fatti su questa molecola (che, come è stato ben ricordato, è una molecola priva di brevetto e quindi liberamente producibile),

2A. «The Guardian», il quotidiano inglese, ha svelato quindi che parecchie pagine del rapporto con il quale l'EFSA stabiliva solo la probabile cancerogenicità erano copiate pari pari dalla relazione con la quale il produttore che voleva rinnovare l'utilizzo per cinque anni aveva fatto questa proposta alla commissione. Quindi è un rapporto dell'EFSA oppure un rapporto della Monsanto, adesso Bayer? Bella domanda anche questa. Tornando alla classe 2A, probabilmente cancerogeno, secondo la definizione l'inserimento in tale classe vuol dire che provatamente è mutageno su linee cellulari animali, sia in vitro che in vivo. Bene, qualunque prodotto che sia mutageno, in grado cioè di indurre mutazioni del DNA che superino il controllo di qualità cellulare, quindi disattivino o aggirino il meccanismo di autodistruzione, può produrre un accumulo di mutazioni più la vita della progenie cellulare è lunga e più le mutazioni irreversibili si accumulano, fino eventualmente ad originare proliferazioni incontrollate. Già di fronte a questa possibilità, il principio di precauzione che, come ha detto giustamente la collega Fattori, deve arrivare prima per un politico, ti fa dire che no, in presenza di questa situazione io non voglio entrare nella diatriba tra chi dice che è cancerogeno e chi dice che non lo è, chi dice che è mutageno e chi dice che non lo è, perché ci sono studi per tutti, ma stabilire il paletto del principio di precauzione. Arrivando agli studi, è inutile che si tiri fuori il fatto che esiste uno studio che dice che non lo è perché, come ho detto, si possono trovare studi che dicono una cosa e anche il suo contrario non ritrattati, né confutati, sia scritti da una sola persona, sia a più mani. quindi importante a livello politico stabilire chi abbia ragione, perché non siamo noi gli arbitri di questo. isoliamo cioè l'effetto glifosato da tutti gli altri effetti che possono essere distorsivi della sua efficacia. Questo è quello che dovrebbe fare la politica.

come dice uno studio tedesco a campione, su 2.000 persone il 99,6 per cento delle loro urine contenevano glifosato. Quindi, siccome lo 0,4 è un errore statistico, il probabilista dice che

guardano le grandi questioni scientifiche attraverso un velo di ignoranza di chi possiede conoscenze diverse e lontane dal glifosato di cui parliamo oggi. Ho sottoscritto e darò il mio voto alla mozione a prima firma della senatrice Cattaneo, non solo perché mi è sembrato di poterne condividere il contenuto, ma soprattutto per una ragione di fondo che la qualifica anche rispetto ad altre mozioni sullo stesso argomento. La mozione della senatrice Cattaneo contiene sia una forte rivendicazione dell'importanza di quel processo conoscitivo nel quale si sostanzia il metodo scientifico, sia il riconoscimento implicito della grande delicatezza del rapporto tra la scienza e la politica. Una mozione, quella della senatrice Cattaneo, che pur partendo da forti basi scientifiche, non proclama verità, non pretende di dare risposte definitive, ma si appella al Governo perché disponga approfondimenti, ricerchi la soluzione anche nel contraddittorio, esiga le prove di ogni affermazione scientifica, investa le risorse necessarie per arrivare a conclusioni solide e inoppugnabili. La ricerca scientifica e la straordinaria evoluzione tecnologica stanno moltiplicando nel Pianeta le disponibilità di strumenti sempre nuovi che possono aiutarci a battere la fame, ad accrescere le conoscenze, a viaggiare, a cambiare la nostra vita, a vincere le malattie e a vivere molto più a lungo. La libertà di ricerca e la fiducia nel progresso scientifico sono due dei grandi pilastri su cui si fondano la civiltà contemporanea e il pensiero moderno ed è da qui che nasce l'esigenza di mettere bene a fuoco il rapporto tra scienza e politica, perché senza una grande alleanza tra la buona ricerca scientifica e la buona politica sarà molto difficile garantire all'umanità un futuro di pace e di giustizia. Poco fa la senatrice Fattori ha ricordato - io credo molto opportunamente - il rapporto tra scienza e politica nella lotta al Covid-19 e lo ha ricordato opportunamente, solo se pensiamo ai gravissimi danni che negli Stati Uniti, in Sud-America e persino in Gran Bretagna sono stati prodotti da governanti che hanno affrontato la lotta al Covid senza tener conto delle prescrizioni della scienza. La guerra tra il presidente Trump e il dottor Fauci mostra con molta evidenza quali siano le conseguenze di una cattiva politica che si contrappone ad una buona scienza. Nelle ultime legislature parti importanti del Parlamento italiano e dello stesso Senato hanno affrontato grandi temi prescindendo dalle evidenze scientifiche ed anzi imponendo punti di vista ed interessi politici, se non anche economici. Non è così che si risponde alle sfide del futuro. Su un tema delicato come il glifosato, la mozione della senatrice Cattaneo indica non la verità, ma la strada che può aiutarci a raggiungerla. Tempo fa, Papa Francesco ha invitato la scienza e la religione ad un dialogo onesto e trasparente, intenso e produttivo per entrambe. Sarebbe veramente paradossale se la politica non riuscisse a cogliere per sé stessa il senso della sfida che Papa Francesco ha lanciato alla religione. Solo un patto responsabile tra la scienza e la politica può avere la forza necessaria per proteggere l'integrità del corso della natura e dei grandi cambiamenti che vengono proprio dallo studio e dalla ricerca. La scienza può aiutare la politica a valorizzare tutte le possibilità che la natura ci offre, ma può farlo solo se sappiamo riconoscerla come un nostro grande alleato, non come un nemico da da combattere e da temere e nemmeno come un elemento fastidioso di cui possiamo non tener conto a seconda del nostro interesse politico o economico del momento. Poco fa, nel suo intervento in Aula, la senatrice Cattaneo ci ha ben illustrato il pericolo grave che il Parlamento potrebbe far correre al Paese se ci lasciassimo andare a decidere non sulla base di chiare evidenze scientifiche, ma sulla base delle nostre sensazioni. Un importante filosofo, Emanuele Severino, ha detto che molti dei grandi mutamenti del nostro tempo sono dovuti non tanto alla forza delle ideologie, quanto ai progressi della quanto ai progressi della scienza e della tecnologia, che ormai si sono poste al centro delle dinamiche della società, emarginando le grandi tradizioni culturali dell'Occidente. La scienza e la politica hanno quindi bisogno l'una dell'altra, ma devono sapersi rispettare, riconoscendo i rispettivi confini. Dobbiamo temere lo scienziato che vuole farsi re e pretende di dominare il mondo imponendo i suoi saperi con le sue scoperte, ma altrettanto - lo dico a me stesso e a chi tra noi, nel rivendicare il giusto primato della politica, pensa di poter scavalcare le verità scientifiche con disinvoltura - dobbiamo temere quella politica che nulla sapendo e nulla conoscendo pretende di invadere il campo delle scienze facendo diventare buono per legge quel che è cattivo e viceversa. È per queste ragioni di fondo,

rappresentanti del Governo, colleghi, dico subito che io non ho tutte le certezze che ho sentito quest'oggi in Aula ed è per questo che credo sia opportuno inizialmente fare chiarezza con una premessa e soprattutto alla fine porre un quesito. I dati sono evidenti e sotto gli occhi di tutti, ad esempio l'Italia - ricordiamocelo - non ha autosufficienza alimentare: a noi mancano 2,3 milioni di di tonnellate di grano tenero. Ricordo a me stesso, ma anche all'Assemblea o a chi ci ascolta, che durante il periodo del *lockdown* ci siamo trovati in una situazione di emergenza e di crisi perché avevamo scorte alimentari di questo prodotto solamente per circa un mese e sono state immesse sul mercato tutte le farine italiane. In Italia - dobbiamo dirlo - abbiamo un grano straordinario come qualità, dal punto di vista dei controlli, perché passa attraverso dei momenti di valutazione che sono attenti,

Come dicevo, io non ho tutte le certezze che ho sentito invece in quest'Aula, perché è un tema complesso, difficile, è un tema che investe la scienza, ma che deve guardare con grande attenzione anche al primato della politica; io sono un sostenitore del primato della politica e quindi della decisione che ognuno di noi deve saper assumere in momenti delicati e difficili, anche quando si esprime un voto su questioni che possono apparire marginali, ma che tali non sono. Ho apprezzato - e lo voglio dire con grande serenità - l'intervento della senatrice Cattaneo, che mi è sembrato estremamente equilibrato, anche perché ha fatto una distinzione fondamentale, cioè quella tra

tutto sommato, per i controlli che vengono realizzati possiamo essere sostanzialmente tranquilli. Parlavo di dati: sapete tutti che il glifosato è un diserbante

pasta. Quando siamo andati a vedere i dati - visto che poi bisogna guardare e confrontarci anche con i dati reali - ci siamo resi conto che i sei marchi di pasta prodotti in Italia sono in assoluto

di glifosato per ogni chilo del proprio peso e così vedere qual è il minimo accettabile. Allora, facendo questa valutazione, che è una semplice operazione matematica, vediamo che la presenza

Credo quindi che possiamo essere sostanzialmente tranquilli anche perché, facendo un calcolo molto semplice, una moltiplicazione del peso di un uomo medio - ripeto di non guardare chi vi parla -, per arrivare alla dose velenosa, pericolosa, dovremmo ingerire giornalmente dai 100 ai 600 chilogrammi di pasta. Questo è il dato vero. Abbiamo un'eccellenza alimentare: io non capisco come mai ci si metta a fare i monaci stiliti, appollaiati sulla colonna di ideologie che secondo me dovrebbero essere superate. Certamente noi non abbiamo - lo ripeto - tutte le certezze, ma credo di poter dire che siamo comunque ampiamente al sicuro. C'è qualcuno che, invece, ha riferito che c'è una situazione genotossica, ma non ne abbiamo alcuna evidenza scientifica. Vi è un altro dato estremamente importante, che riguarda la produzione del grano.

Sapete quanto produce la Francia? La Francia produce quasi dieci volte quello che produciamo noi: 37 milioni di tonnellate.

tonnellate. Ci troviamo quindi in una situazione di estrema difficoltà. L'Italia, se vuole risolvere anche il problema del glifosato, qualora avesse qualche dubbio, dovrebbe avviare una nuova battaglia del grano: dovremmo riappoderare i nostri terreni e coltivarli in quella prospettiva e in quella direzione. Lo vogliamo fare? Abbiamo preso altre direzioni, al contrario: abbiamo inseguito l'energia pulita, quella verde. Mi riferisco al fotovoltaico, che ha sostituito nei campi molte coltivazioni; abbiamo preferito mettere il fotovoltaico, che ha prodotto poco, rispetto all'appoderamento e alla coltivazione di alimenti estremamente importanti, dimenticandoci che in fondo l'agricoltura è realmente il settore primario ed è quello che noi dovremmo difendere. lo ripeto - non ho tutte queste certezze, valuterò con attenzione ogni mozione che è stata presentata. Con molta serenità vi dico che il nostro grano è caratterizzato da una sicurezza alimentare davvero straordinaria. Quando il grano proveniente dagli Stati Uniti o dal Canada

oggi parliamo di un argomento molto importante, anche se penso che non sia molto conosciuto da tutti i cittadini. È un argomento venuto alla ribalta in quest'ultimo periodo per i ragionamenti fatti

in quest'Aula emergerà se sia pericoloso o no: almeno io, personalmente, non ho quella conoscenza tecnico-scientifica analitica per permettermi di dare un giudizio così preciso.

alla IARC, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, o all'AIRC, l'Agenzia italiana per la ricerca sul cancro, che hanno detto che il glifosato molto probabilmente è potenzialmente pericoloso.

Non credo assolutamente che l'agricoltura italiana abbia bisogno di questo, però gli agricoltori italiani devono poter competere alle stesse identiche condizioni con gli agricoltori degli altri Paesi dove invece è consentito

Se vogliamo analizzare, dal punto di vista tecnico, il metodo di coltivazione per cui il glifosato viene usato in agricoltura, vediamo che si risparmia molto adoperandolo soprattutto - e questo è un un argomento prettamente tecnico - sulla semina, sul sodo: si dà una bella irrorazione di glifosato, poi si semina sul sodo e il lavoro è bello e finito: il prodotto cresce rigoglioso senza spendere soldi di aratura, di erpicatura, di fresatura del terreno.

fa fatica a non usare prodotti di questo tipo pur di avere un minimo di reddito. È quel minimo di reddito che la politica, invece, gli deve garantire. Noi abbiamo una grandissima estensione di territorio del nostro Paese, soprattutto nel Sud Italia, che sarebbe votato alla coltivazione del grano, ma se non diamo a queste persone la possibilità di sopravvivere incentivando la filiera del grano, in particolare del grano duro, è difficile che i nostri agricoltori vadano vadano a impegnare le proprie risorse su tale coltivazione. Quindi, alla fine siamo costretti a importarlo. Sentivamo prima diversi colleghi

in Commissione agricoltura, il quale ci ha raccontato come avvengono i controlli sulle navi da parte dei tecnici dell'Istituto - vedo il senatore De Bonis che annuisce, essendo stato il promotore di questa audizione

però la campionatura fisico-tecnico-scientifica sul grano avviene a campione: due navi su dieci, cinque navi su dieci, una nave su dieci, a seconda di una determinata casualità che loro vanno a decidere. Mi rivolgo al sottosegretario Sileri: la prego, faccia

nei nostri porti, non solo in Puglia ma anche negli altri porti dove arriva il grano duro dai Paesi esteri, siano controllate una per una perché ne va della salute dei nostri cittadini.

Presidente, gentili colleghi, vi chiedo ancora un po' di pazienza perché vorrei provare ad utilizzare questi minuti per inquadrare meglio alcuni aspetti tecnici, forse per arrivare alla conclusione che è quella promossa dalla mozione - che di fatto serve una disamina, serve a mio avviso un impegno conferito al Governo affinché i suoi organismi si facciano carico di raccogliere la letteratura e le informazioni tecnico-scientifiche sul glifosato che riguardano l'ambiente, la salute, gli scambi, le importazioni e i costi economici dell'usare o del non usare questo prodotto. Quindi, questo è esattamente l'obiettivo della mozione. Ci tenevo anch'io a intervenire tornando all'esempio del grano perché è chiaro che è qualcosa che ci colpisce; è stato già citato dai senatori Aimi e Vallardi,

ci tocca molto, anch'io volevo tornare sui numeri perché anch'io ho fatto dei calcoli. Noi siamo terrorizzati dal glifosato, diciamolo. È il nemico perfetto: erbicida, costa poco, c'è dietro la Monsanto, ci sono gli studi sulla probabile cancerogenicità e lo dice una sola associazione (IARC) (le altre 19 che che valutano il rischio dicono di no). Lasciamo, però, tutto questo alla disamina che spero venga fatta a valle della mozione. Facciamo finta di essere veramente terrorizzati dal glifosato perché è il nemico perfetto. Andiamo allora a vedere quanto glifosato c'è

di nanogrammi per chilo o per litro, pari a una goccia o meno in una piscina olimpionica o una capocchia di spillo in un tir di pasta. pasta. Ce n'è pochissimo e teniamo presente, come ha detto il senatore Aimi, che il limite di glifosato per legge previsto per il grano è di 10 milligrammi per chilo e, se andiamo a misurare, ne troviamo da 54 a 526 volte meno.

come ha detto il senatore Aimi, dovremmo assumere tra i 100 e i 600 chili di pasta al giorno tutti i giorni della nostra vita, fino all'ultimo giorno, e non arriveremmo ancora ai livelli di

come nel periodo Covid, perché si sta facendo un dibattito pubblico. È il momento in cui si sta scoprendo e si stanno studiando diverse tematiche e diversi ambiti. C'è divisione perché non c'è ancora

Sulla storia della scienza divisa e mi viene in mente quando all'epoca Stamina si sentiva dire «la scienza è divisa», e la divisione era uno di qua e centomila di là.

come se fosse una prova di colpevolezza, guardate che questo fa parte del fascino e anche della complessità dell'argomento: com'è che la Bayer - che ha acquisito Monsanto

120.000 cause di agricoltori che hanno fatto causa alla Monsanto? Vi sarà capitato di girare negli Stati Uniti; più volte mi sono trovata di fronte a cartelli pubblicitari che dicevano: «Hai un tumore? Hai lavorato o sei passato vicino a un terreno in cui è stato sparso del glifosato? Vieni da noi». Sono questi studi di avvocati (è una tecnica

come la scienza non si può sostituire alla politica, neanche un tribunale si può sostituire alla scienza; la scienza non si fa in tribunale. Se andate a leggere che cosa è stato detto durante il dibattito in tribunale di questa causa, potrete verificare che non c'è un'ammissione di colpevolezza. La Bayer continua a sostenere l'assenza di prove di cancerogenicità di questo prodotto e la dimostrazione è che - potete verificarlo sul sito *web* della Bayer - continua a produrre

tra la decisione di chiudere quelle migliaia di cause e una presunta colpevolezza. Ci sarebbero molti altri argomenti da trattare, ma forse l'aspetto più importante da ricordare è quali possono essere le conseguenze di un divieto e quale sarebbe la conseguenza per i nostri imprenditori agricoli e per la nostra agricoltura, già altamente sofferente. Mi chiedo anche come facciamo a diserbare strade, autostrade, ferrovie e aree verdi pubbliche per la sicurezza di tutti noi. Non c'è alternativa. Continuiamo a studiare; non è vero che guardando dentro la scienza ci trovi di tutto, perché le pubblicazioni possono essere pesate. Ci sono pubblicazioni che non valgono niente e ci sono pubblicazioni che dimostrano che su 50.000 agricoltori non c'è alcuna correlazione con lo sviluppo di tumori. C'è uno studio bellissimo

del dispositivo sia riformulato come segue: «assumere ogni idonea iniziativa in sede europea per promuovere la revisione delle decisioni assunte in merito all'utilizzo del glifosato con regolamento di esecuzione UE 2017/2324 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, e a valutare la possibilità di sospendere nelle more gli effetti del comunicato del Ministero della salute del 19 dicembre 2017 con cui si è recepito il rinnovo della sostanza attiva glifosato per cinque

Chiedo ai presentatori delle mozioni di dirci se accettano le condizioni poste dal Governo.

in questi anni troppo spesso la politica ha compiuto delle scelte prescindendo dalle indicazioni della scienza. Questo è paradossale in un'epoca nella quale si fa un gran parlare dell'importanza delle competenze, che poi però vengono sistematicamente disattese per farsi guidare dalla paura o da altri sentimenti che attraversano l'opinione pubblica. Gli esempi sono davvero tantissimi: dalla paura per i vaccini che in certi ambienti continua a permanere, nonostante l'esperienza drammatica del Covid-19, quella per il 5G, nonostante ad oggi non esista alcuna evidenza scientifica sui danni alla salute. Ricordo anche il metodo Stamina che, cosa gravissima, entrò come sperimentazione in alcuni ospedali nonostante la netta opposizione della comunità medica. Il decisore politico deve essere sempre guidato dai principi della prudenza, ma deve basare le sue decisioni sull'evidenza e sul metodo scientifico, che rappresenta il discrimine tra una società moderna e una premoderna in cui le decisioni si prendevano sulla base del pensiero magico e delle superstizioni. Per queste ragioni, nel dibattito sul glifosato reputiamo di grande pertinenza la mozione presentata dalla senatrice Elena Cattaneo. Il merito di questa mozione è quello di ripristinare un metodo senza schierarsi a favore o contro, perché non conta l'approdo ma il rigore con cui vi si giunge, e conta il fatto che il legislatore abbia dalla sua tutte le informazioni scientifiche prima di potersi esprimere su un tema così importante. La verità è che le scelte non sono sempre il risultato di una meditata riflessione sulla base di dati oggettivi ed esaustivi e questo la dice lunga proprio sul processo decisionale relativo a materie dove si presta meno attenzione a quante cattive misure misure a volte si introducono per via di un processo di valutazione che si basa su informazioni inesatte o incomplete. Questa mozione è anche un invito ad avviare una riflessione sull'intero meccanismo della decisione pubblica, soprattutto in un'epoca in cui le materie sono sempre più complesse, ricche di sfumature e di implicazioni e inquinate dalle *fake news* che circolano sulla Rete e che sanno aizzare sentimenti di paura e di sfiducia. L'impegno da chiedere al Governo non è quello di schierarsi ma di dotarsi di un metodo, acquisendo e, laddove necessario, producendo tutte le informazioni utili per poi coinvolgere il Parlamento, che deve restare il luogo del confronto su temi così importanti e sentiti dalla cittadinanza. Per questo il nostro Gruppo esprimerà un voto favorevole alla mozione Cattaneo.

della mozione, dagli interventi che sono stati fatti e anche dalla senatrice Cattaneo nel proprio intervento, possa essere davvero l'occasione per poterci interrogare su quanto le nostre scelte politiche debbano basarsi su fatti di evidenza scientifica e quanto debbano invece essere influenzate dalle percezioni,

le verità che la scienza ci può offrire attraverso le proprie ricerche, attraverso i propri approfondimenti, attraverso la condivisione e il confronto di diversi studi, ci possano davvero aiutare a fare scelte appropriate.

che non hanno trovato riscontri nella realtà. Un passaggio della mozione che mi pare davvero importante, ed è stato sottolineato sempre della senatrice Cattaneo nel suo intervento, è quello relativo alla differenza tra il pericolo e il rischio. Appare di tutta evidenza - avete letto le mozioni e se avete letto l'articolato della mozione a prima firma Cattaneo - che c'è davvero una differenza di approccio nella modalità con la quale le diverse autorità scientifiche hanno condotto i propri studi, i propri percorsi e anche come hanno definito le proprie posizioni. nel 2015, classificando il glifosato tra le sostanze probabilmente cancerogene, inserendo questo elemento nel gruppo 2A, non ha definito quale sia il rischio

umano di tipo 68, nonché i composti del piombo. C'è addirittura la malaria causata da infezioni da Plasmodium falciparum nelle aree endemiche, cui si aggiungono anche le esposizioni professionali in spruzzatura e applicazione di insetticidi non arsenicali

elementi che risultano pericolosi, senza definire quello che è il rischio. Se avete letto l'articolato della mozione, si evince in maniera chiarissima come

dall'utilizzo di glifosato, quindi una condizione assolutamente impossibile da verificarsi. Al netto di queste considerazioni molto specifiche, il principio che sta alla base di questa mozione e che ci spinge quindi a sostenerla, a votare a favore e a chiedere a tutta l'Assemblea di sostenerla, è proprio

le ricerche alle quali oggi si può accedere per permettere all'Assemblea e alle Commissioni di avere un'evidenza chiara, precisa e scientifica di quella che è la realtà, di quelli che sono i reali rischi e non solo dei rischi e non solo dei pericoli che, lo ribadisco, sono diffusi per molte altre sostanze. Se procederemo in questa direzione e avremo quindi elementi molto chiari che ci dicano

assunto e legato alle evidenze che la scienza ci può fornire, non soltanto con ricerche che mettono in luce i possibili pericoli, ma, soprattutto, con la misurazione dei reali rischi in questo caso legati ad una sostanza specifica come il glifosato.

dibattuto e di cui se ne sono occupati moltissimi organismi scientifici. Potrei qui ampiamente citare altrettanti esponenti del mondo scientifico e del mondo medico,

in modo efficace e molto pesante a tutela dei consumatori, vi sono state recenti sentenze che hanno condannato la Monsanto a risarcimenti miliardari.

da ogni punto di vista e soprattutto dal punto di vista scientifico; poi possiamo fare tutti gli approfondimenti che vogliamo, ma abbiamo già delle evidenze scientifiche e, torno a ripetere, potremmo portare in Aula trattati su trattati. Ebbene, noi chiediamo

dei Paesi europei e soprattutto del nostro Paese. Ho sentito affermazioni in cui si dice che il nostro grano è di scarsa

Paese è stato un grande produttore, abbiamo fatto negli ultimi tempi dei progressi incredibili dal punto di vista della qualità,

A noi invece garba, riteniamo che puntare sulla qualità, sulla sicurezza alimentare, sulla filiera corta, sulla produzione biologica sia

per la competizione dei nostri prodotti e per il rispetto della qualità della nostra agricoltura, che assumessimo qui delle decisioni importanti. Questo Parlamento può sostenere il nostro Paese per fare in modo che in Europa si riveda l'autorizzazione, che vengano messi in atto una serie di controlli sulle importazioni sulle importazioni - perché sulla questione dei residui credo che dovremo lavorare ancora di più - prevedendo quindi una serie di possibilità, che indichiamo nella nostra mozione, per

come ha dimostrato anche la replica del sottosegretario Sileri, per fare in modo che il nostro Ministero della salute sia pronto a intervenire e faccia tutti i passi per fare in modo che non sia prorogata l'autorizzazione, ma che anzi sia revocata, che nel nostro Paese ci sia la sicurezza di avere prodotti assolutamente

e contraddice gli elementi scientifici che noi abbiamo portato nella discussione odierna e soprattutto non fa il bene del nostro Paese, della salute dei cittadini e degli interessi italiani in campo agricolo.

TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia nella consapevolezza di tutti quanto nell'ultimo secolo, ma soprattutto nei decenni del Dopoguerra, la ricerca scientifica e l'innovazione a questa connessa abbiano messo a disposizione dei cittadini e delle comunità, quantomeno in larga parte del mondo, strumenti e opportunità che hanno come mai nella storia permesso di aiutare l'uomo a soddisfare i propri bisogni e a liberarlo da tante limitazioni e vincoli che ne avevano caratterizzato l'esistenza nei decenni passati. Non è un caso che le aspettative di vita si siano ampliate e che la nostra percezione di normalità o di legittima aspettativa si siano innalzate in merito alla qualità della vita, quantomeno rispetto a tanti aspetti pratici della stessa, abbiamo scoperto anche, con sempre maggiore evidenza ed è cresciuta in questi anni in noi la consapevolezza che tutte le nostre azioni hanno, proprio per questa pressione tecnologica che abbiamo messo in campo, molto più che in passato, riverberato sul contesto ambientale nel quale viviamo e sull'ambiente in generale, sulla nostra stessa salute e su quella del Pianeta, conseguenze ed impatti non sempre solo positivi. In molti casi, siamo stati costretti a rettificare i comportamenti, a darci delle regole più stringenti, a fare marcia indietro, a rivedere convinzioni e decisioni che pensavamo sagge e fondate. a mo' di esempio, la storia dell'amianto, dell'utilizzo industriale della fibra di amianto. Messa in campo a fine Ottocento, sembrava aver risolto tecnologicamente molti sistemi produttivi; all'inizio del Novecento ci furono le prime sensazioni di pericolosità connessa all'utilizzo di questi materiali; negli anni Trenta studi e denunce hanno evidenziato le conseguenze che questo utilizzo portava. Questo è durato fino alla fine degli anni Settanta. Negli anni Ottanta la consapevolezza acclarata dell'asbestosi e del mesotelioma ha portato poi, all'inizio degli anni Novanta, al divieto di utilizzo, nel Piemonte, con epicentro a Casale, si sono avuti migliaia di morti e decine di migliaia di famiglie rovinate dalla presenza di questi materiali. La storia di tante grandi scoperte e di tanti salti avanti dell'umanità ha comportato rischi e a volte la necessità di fare passi indietro per creare le premesse per poter nuovamente andare avanti, ma in modo più giusto ed equilibrato. In fondo, questa è la storia della chimica e dell'innovazione tecnologica in agricoltura, che ha permesso - sia ben chiaro - di fare enormi passi avanti. Quando negli anni Sessanta fu varata la Politica agricola comunitaria (PAC), l'obiettivo che fu affidato a questa politica era di dar da mangiare agli europei e di evitare il rischio di una mancanza pesante di autosufficienza alimentare. Questa è anche la consapevolezza che ha riguardato i percorsi di moltissime attività umane e che ha portato a mettere in campo iniziative, tecnologie e prodotti che poi hanno dovuto essere ritirati. Io vivo in un'area a fortissima vocazione agricola specializzata, soprattutto per quel che riguarda la frutticoltura e la vitivinicoltura e credo di non svelare un segreto se dico che la qualità e la sicurezza delle nostre vite, della nostra salute e dell'impatto ambientale oggi è nettamente superiore a quella che abbiamo vissuto negli anni Ottanta. Ricordo ancora quando, da ragazzino, allestivo un frutteto familiare e mi recai da un rivenditore di prodotti per l'agricoltura fitoiatrici e questo rivenditore mi consigliò alcuni insetticidi ad ampio spettro d'azione di straordinaria efficacia, che in quel momento erano legittimamente autorizzati all'uso, che qualche anno dopo furono ritirati dal mercato perché avevano un impatto devastante sulla salute e sull'ambiente in cui erano chiamati ad operare. Moltissimi prodotti ritenuti sicuri e che avevano avuto autorizzazioni, dopo anni sono stati oggetto di un ripensamento. La storia dell'attività umana è la storia di una materia in divenire, in termini di conoscenza scientifica, di consapevolezza tecnica, comunitaria, politica e di tangibili percezioni e riscontri esperienziali. Proprio questa consapevolezza, illuminata dal principio di precauzione, su queste tematiche ha portato l'Unione europea ad una revisione delle proprie convinzioni e delle proprie linee normative. La classificazione tossicologica dei fitofarmaci e l'etichettatura, che è l'esito di un processo iniziato trent'anni fa, con la direttiva n. 414 del è stata oggetto di una profonda revisione per tutelare la salute umana, per tutelare l'ambiente e al tempo stesso mettere a disposizione dei produttori i mezzi idonei a proteggere le colture.

128 del 2009 sull'uso sostenibile, con procedure più rigide per l'approvazione dei prodotti fitosanitari; quest'ultima è stata poi recepita a livello nazionale dal decreto legislativo n. 150 del 2012 che ha portato al Piano e ha fatto emergere una serie di criticità che sono oggetto di osservazione nel quinquennio 2019-2024 e che saranno poi valutate all'esito da un comitato scientifico.

la peculiarità di essere facilmente degradabile negli strati superficiali del terreno, quindi da un punto di vista tecnico-agronomico è sicuramente un prodotto molto efficace e molto utile. è anche un prodotto che, come è stato detto nelle discussioni che abbiamo sentito, ha sollevato paure e perplessità molto importanti. Molte di queste paure sono legate a perplessità emerse nell'utilizzo nel corso degli anni. Sicuramente, chi come me lo ha utilizzato sa che non è una passeggiata farlo, perché anche da un punto di vista olfattivo e dell'impatto che rilascia è molto pesante. suscitato molte perplessità soprattutto alcuni utilizzi che ne sono stati fatti: è già stato detto prima che immaginare l'utilizzo di questo prodotto come disseccante laddove produzioni di grano duro non riescono ad andare a maturazione sicuramente suscita in noi sensazioni molto pesantemente negative.

di oltre 10 miliardi di dollari per tacitare gran parte dei ricorsi che erano in campo, solleva qualche dubbio e perplessità al di là di ogni ragionevole incertezza.

dell'indipendenza delle valutazioni scientifiche che verranno utilizzate in vista della revisione dell'autorizzazione all'utilizzo, che sarà fatta tra pochi anni, come anche l'aver richiesto al Governo un investimento importante sui controlli per rafforzare soprattutto le produzioni che arrivano dagli ambiti produttivi nei quali c'è un uso, dal nostro punto di vista, molto distorto di questo prodotto e l'impegno a rendicontare a questo Parlamento

nel percorso che ci porterà alla revisione delle autorizzazioni. A nostro avviso, inoltre, è importante che il Parlamento su queste tematiche, alla luce di tutte le evidenze scientifiche che dovranno essere messe in campo, possa esprimersi perché è un aspetto importante della nostra vita che crediamo non possa essere relegato dalla politica

Signor Presidente, gentili colleghi, l'emergenza da coronavirus ha creato nei cittadini italiani una nuova consapevolezza del valore strategico della filiera agroalimentare e della difficoltà che purtroppo ogni giorno i nostri agricoltori incontrano e superano, per garantire quegli alimenti di alta qualità che rendono grandi i nostri prodotti enogastronomici nel mondo. La materia che stiamo trattando oggi, pertanto, assume sotto questa nuova luce un'importanza maggiore, in quanto è nostro dovere garantire la salubrità di questi alimenti. In questo senso, l'uso del glifosato divide da anni il mondo scientifico (nuoce, non nuoce), oltre che produttori e consumatori, in particolare questi ultimi mondi, contrapponendoli un po': da una parte i consumatori, che giustamente hanno il diritto di essere tutelati mangiando cibi sani, salubri e corretti, e dall'altra i nostri produttori agricoli, che vengono quasi tacciati di utilizzare prodotti che fanno male e nuocciono alla salute. Forse si cerca l'idea facile del nemico pubblico. Negli Stati Uniti assistiamo a numerose cause di risarcimento intentate da cittadini che lamentano danni alla loro salute, dovuti all'utilizzo eccessivo di questa sostanza nella filiera agroalimentare. Vero, queste situazioni ci allarmano sicuramente, pur nella consapevolezza che gli eccessi tipici delle colture intensive nordamericane non appartengono al nostro *modus operandi*. Vorrei tuttavia porre l'accento del dibattito su un altro tema, oltre a quello già ampiamente discusso dai colleghi sulla tutela della salute. Mi riferisco alla necessità di armonizzare la normativa a livello nazionale (ma in realtà si auspica anche a livello comunitario, europeo e anche oltre). Come è noto, infatti, le direttive regionali sull'utilizzo del glifosato differiscono profondamente, ad oggi. Ho denunciato con forza, prima di tutto da imprenditrice agricola, come gli agricoltori della mia Regione, la Calabria, abbiano subito nel 2016 un danno concorrenziale importante a a causa della scelta della Giunta regionale dell'epoca di impedire l'uso del glifosato e dei pesticidi, da un giorno all'altro, per le produzioni integrate. Vedete, colleghi, non usare questo prodotto costringe i nostri imprenditori agricoli ad utilizzarne altri meno performanti e più costosi. Tutto ciò provoca un aumento esorbitante dei costi, che però, per non gravare sui consumatori, non viene compensato da un uguale aumento dei prezzi di vendita, cagionando dunque un'erosione importante dei ricavi. Sappiamo, colleghi, che i profitti sono già seriamente compromessi da fattori climatici, di mercato, oltre che da danni e problematiche causati dagli agenti patogeni e da animali esogeni al nostro ambiente e, da ultimo, ma non in ordine di importanza, dalla concorrenza sleale provocata appunto da disparità nelle regole produttive. Dunque, approvare questa mozione serve anche per permettere a tutti di giocare ad armi pari, riequilibrando il mercato almeno a livello nazionale. naturalmente, tuteliamo la salute dei nostri concittadini. In tal senso, però, auspichiamo che si continui nella ricerca sul tema, visto che gli organismi comunitari alla valutazione dei principi attivi non sono ancora giunti ad una decisione unanime e certa. Ad esempio, si dimostra che, se utilizzato nelle giuste quantità, come è stato già detto, non ci sono motivi di preoccupazione particolari. Semmai i problemi sussistono sugli alimenti di importazione, come è stato già ampiamente ricordato. È importante quindi che ci si continui ad affidare alle comunità scientifiche, così come è stato fatto nel recente periodo con riferimento al Covid-19, quando la maggior parte delle decisioni sono state affidate proprio alle comunità scientifiche. Perché in questo caso non bisogna continuare a farlo? Come dicevo poco fa, i consumatori italiani durante questa emergenza hanno compreso l'importanza di comprare i prodotti nazionali per sostenere l'occupazione e l'economia italiana. In particolare, è notevolmente aumentato il consumo della pasta italiana, che utilizza solo grano nazionale, e dei legumi.

dei banconi alimentari dei nostri supermercati. La seconda ragione è perché, così facendo, si difende il *made in Italy* dalla concorrenza sleale di prodotti esteri che, non rispettando le stesse regole in tema di sicurezza alimentare

di assumere ogni idonea iniziativa in sede europea per promuovere la revisione delle decisioni assunte, in merito all'utilizzo del glifosato, con regolamento di esecuzione (UE) n. 2324 del 2017 e ad adottare le necessarie di precauzione su tutto il territorio nazionale volte a proteggere la sanità pubblica, nonché la salubrità dell'ambiente con specifico riferimento alla tutela delle acque, della flora promuovere, anche mediante lo strumento della decretazione d'urgenza, tanto utilizzato, degli interventi normativi finalizzati a vietare l'utilizzo e la presenza della sostanza attiva glifosato negli alimenti.

Noi riteniamo che la salute dei cittadini, delle nostre imprese e dei nostri agricoltori vada tutelata e che vadano garantiti i diritti dei consumatori.

bisogna capire se sia effettivamente vantaggioso per il nostro Paese, perché le nostre tavole non hanno bisogno di prodotti potenzialmente nocivi.

scientifico, sanitario e - soprattutto - di genuinità del prodotto, sta toccando profondamente il consumatore. Secondo gli ultimi dati forniti dall'Istat, nell'anno appena trascorso le quantità dei principali cereali, semi oleosi e farine proteiche prodotte evidenziano un tasso di autoapprovvigionamento in complesso di appena il 41 per cento del nostro fabbisogno interno. Ciò significa che noi importiamo il 59 per cento di questa tipologia di materie prime. Il tutto provoca una perdita, per la nostra agricoltura, pari a 4,5 miliardi di euro in termini di mancata produzione, con uno speculare aggravio di spesa sulla nostra bilancia commerciale. Le criticità maggiori riguardano oltretutto quelle produzioni strategiche e non rinunciabili per l'agroalimentare italiano, come il mais, il grano e le farine di soia.

La ricerca di grano 100 per cento *made in Italy* si scontra però con anni di disattenzione e abbandono, che nell'ultimo decennio hanno portato alla scomparsa di 1 campo su 5 a livello nazionale, con la perdita di quasi mezzo milione di ettari coltivati ed effetti dirompenti sull'economia agricola, sull'occupazione, sull'ambiente e sull'agroalimentare in generale. Una situazione aggravata dalla concorrenza sleale delle importazioni, soprattutto da aree del Pianeta che non rispettano le stesse regole di sicurezza alimentare in vigore nel nostro Paese, come il Canada, appunto, dove il grano duro per la pasta viene trattato con l'erbicida glifosato prima del raccolto, in modalità vietate sul territorio italiano, dove invece la maturazione avviene grazie alla natura, grazie al sole. Se vogliamo puntare a prodotti di altissima qualità e quindi alla garanzia che tali prodotti siano diversificati a livello mondiale, bisogna incrementare la ricerca; ma per farlo è necessario intraprendere un percorso di innovazioni per rintracciare alternative sostenibili all'utilizzo del glifosato. È chiaro che questo processo richiede tempo, e siccome di tempo ne abbiamo già perso abbastanza, invitiamo il Governo a darsi una sveglia dal letargo su questo argomento: si assuma le sue responsabilità, soprattutto il Ministro dell'agricoltura, altrimenti può sempre cambiare mestiere rispetto al lavoro che sta facendo adesso. *(Applausi)*. Ma se non sa che pesci prendere, suggeriamo volentieri noi cosa c'è da fare, ad esempio, puntare sulla ricerca che valorizzi la qualità dei prodotti. Oggi, infatti, il consumatore compra prodotti sani, come emerge dai dati relativi alle ricerche di mercato: il consumo del biologico aumenta dal 14-15 al 20 per cento annuo, quindi, il consumatore sta già dando indicazioni al Governo, al Ministro, alle organizzazioni di categoria, sulla strada da percorrere. chiaro - è l'adozione di un piano sementiero nazionale serio, che punti a far crescere il settore e ad assicurare al sistema agroalimentare sementi tracciate italiane e di qualità. È necessario individuare gli ambiti di azione e gli strumenti idonei a realizzare il potenziamento del comparto sementiero. Gli obiettivi che un piano sementiero si deve porre sono, intanto, accrescere la produzione sementiera per essere competitivi come settore a livello Italia, ma anche a livello mondiale, garantire ai produttori agricoli gli approvvigionamenti di sementi e semplificare le procedure burocratiche legate all'attività sementiera. Oggi è più che mai importante investire sull'agricoltura italiana per poter offrire produzioni di qualità realizzando rapporti di filiera virtuosi, con accordi che valorizzino, sì, il *made in Italy*, ma anche la sostenibilità della produzione in Italia. Un impegno importante per garantire la sovranità alimentare del nostro Paese e ridurre la dipendenza dall'estero, in un momento in cui l'emergenza della pandemia ha evidenziato tutte le criticità del commercio internazionale. Per tali ragioni si ritiene di assoluta necessità per l'Italia sviluppare le azioni già messe nero su bianco dalle associazioni dei produttori e consegnate al Presidente del Consiglio e ai Ministri competenti. Il Governo deve essere il regista di queste situazioni, non può fare l'ultimo degli spettatori. Intanto, deve incentivare quanto più possibile le produzioni nazionali nel comparto agroalimentare attraverso un sistema di incentivi comunitari e nazionali diretti agli agricoltori, che sono l'anello debole della filiera, in questa prima fase di emergenza anche utilizzando al massimo consentito quanto indicato nella recente comunicazione della Commissione europea, il *temporary framework*. Poi, occorre mantenere alta l'attenzione sul negoziato europeo per la Politica agricola comune, chiedendo a gran voce di mantenere inalterato il *budget* della PAC - è fondamentale - e in parallelo stimolare la politica di sviluppo sostenibile attraverso le altre linee di spesa dedicate al *green deal* europeo. ancora promuovere i sistemi di premialità, soprattutto a chi produce queste materie prime, essere consapevoli di farlo, ma in tempi brevi; rafforzare e favorire una maggiore attività di ricerca e consentire la libertà di utilizzo e accesso all'innovazione, compresa l'agricoltura di precisione, fondamentale per combattere tutti quelli che sono i parassiti a livello di agricoltura, gli infestanti, favorendo anche le semine in quei terreni che negli ultimi anni sono stati messi a riposo, in applicazione delle misure agroambientali oppure che sono stati del tutto abbandonati dalla produzione agricola. Queste sono una serie di misure che servono per implementare la produzione di qualità italiana sostenendola in modo reale e non soltanto a parole. Per tutte queste ragioni, oltre a quelle dette in precedenza dai colleghi, votiamo favorevolmente alla nostra mozione. Ringraziamo anche il Governo per non averla modificata. È una mozione equilibrata tra ciò che sta vivendo il Paese Italia in questo momento, le mille difficoltà per le importazioni di prodotti dall'estero che non sono coerenti con la nostra qualità e genuinità

altrimenti rischiamo di fare un mucchio di parole senza arrivare a risultati concreti per la produzione dell'agricoltura italiana. Questo è il tempo delle scelte, soprattutto per quanto riguarda la prima parte della filiera. Non ci vogliono più tentennamenti. Lo chiediamo al Governo e al Ministro delle politiche agricole, che è sempre presa da mille aspetti di politica generale, mentre abbiamo bisogno di concretezza per questa parte produttiva del nostro Paese: prima la salute degli italiani e la qualità dei nostri prodotti. *(Applausi).*

il glifosato, il diserbante ed erbicida ad ampio spettro più venduto nel mondo, è una sostanza chimica che mostra effetti sul sistema endocrino e la produzione ormonale sia negli animali che nell'uomo. Soprattutto è una sostanza potenzialmente capace di provocare tumori. Nelle zone di produzione soprattutto di cereali, dove viene ancora utilizzato in maniera intensiva e massiccia, si evidenziano problematiche cliniche sia a livello ormonale che renale collegate direttamente all'assunzione continuativa e protratta di glifosato. Tale sostanza ha dimostrato, infatti, di abbassare i livelli degli ormoni sessuali, in particolare di testosterone, estrogeni e progesterone, di favorire la prevalenza estrogenica sia nell'uomo che nella donna. In particolare, nell'uomo fa abbassare i livelli plasmatici di testosterone, con conseguente riduzione della libido e della potenza *coeundi*, mentre nella donna aumenta il rischio di sviluppare il cancro degli organi sessuali (ovaie e utero). Il Centro internazionale di ricerca sul cancro (CIRC) considera il glifosato come una sostanza dal potenziale cancerogeno per l'essere umano. Anche l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) nel 2015 ha inserito il glifosato in un gruppo di 66 sostanze a rischio e lo ha classificato come probabile cancerogeno. L'Unione europea ha inserito il diserbante tra le sostanze che possono agire come interferenti endocrini. Importante è il ritrovamento di tale erbicida nelle urine umane, a volte in concentrazioni superiori alla norma, e nelle secrezioni esogene come il latte materno. Quest'ultima circostanza è da valutare con particolare attenzione per i rischi connessi al conseguente passaggio al lattante attraverso tale modalità. modalità. Il glifosato viene ritrovato ovviamente nelle farine di frumento e del pane, con tutte le conseguenze legate al consumo di tali sostanze.

ridurre i tempi di produzione, aumentare la resa quantitativa di tali prodotti, riducendo le difficoltà legate al clima e ottenere produzioni più tempestive e più competitive sui mercati internazionali, che risultano monopolizzati in tal senso. Infatti, negli Stati Uniti e in Canada il glifosato viene ampiamente utilizzato nelle coltivazioni di grano duro per favorirne una maturazione artefatta, ma più rapida. La conseguenza di ciò è la sua presenza in quantità non trascurabili nei grani raccolti e nelle semole da essi derivanti. L'Italia è importatrice da questi Paesi di grano duro per la produzione di pasta, pane e altri prodotti da forno di largo utilizzo presso i consumatori. Il risultato finale di tutto ciò è sotto gli occhi di tutti: la stragrande maggioranza delle nostre paste, salvo qualche marchio, contiene concentrazioni di tale erbicida estremamente significative, pur non superando i limiti imposti dalle norme di legge attuali. Un passaggio che volevo sottolineare è che, nonostante sia oramai riconosciuta la nocività di tale sostanza e la sua potenziale cancerogenicità, la Commissione europea nel dicembre del 2017 ha ritenuto di rinnovare per ulteriori cinque anni l'autorizzazione all'immissione e all'utilizzo del glifosato nell'ambito dei territori della UE. Credo che il principio di precauzione invocato quando un prodotto può avere effetti scientificamente dimostrati come potenzialmente pericolosi e lesivi per la salute umana, pur non riuscendo a quantificare e determinare con sufficiente certezza tale rischio, si possa e si debba applicare. Questo principio è perfettamente in linea con le caratteristiche del glifosato, proprio in ottemperanza alla necessità non demandabile, ma inviolabile di tutelare la salute pubblica. Logica conseguenza dovrebbe essere il divieto definitivo della produzione, della commercializzazione e dell'utilizzo in agricoltura dei prodotti fitosanitari contenenti tale erbicida. La prevenzione di cui tanto spesso si parla e che costituisce un cardine importante e fondamentale della nostra organizzazione sanitaria, insieme alla fase assistenziale, territoriale e ospedaliera e alla fase riabilitativa,

lesive dell'integrità psicofisica dei cittadini o a sostanze potenzialmente nocive per la salute di tutti noi. Essa può e deve trovare in questo caso la sua giusta applicazione e la sua efficace dimostrazione. Credo che rimuovere ed eliminare qualcosa che sia anche solo potenzialmente patogeno, senza se e senza ma, rappresenti un obbligo morale nei confronti dei cittadini e un rispetto per le conoscenze di tutti. *(Applausi)*. Solo così si possono dare risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini. Occorre promuovere interventi normativi finalizzati a vietare concretamente l'utilizzo del glifosato e la sua conseguente presenza negli alimenti. Concludo invitando tutti ad una maggiore attenzione verso il consumo dei prodotti nostrani, sempre più biologici e liberi dall'uso e abuso di diserbanti e pesticidi. Non occorre fermarsi all'apparenza; è necessario quindi scegliere un prodotto meno perfetto e meno appariscente, ma che sicuramente ha meno possibilità di essere trattato rispetto a prodotti esteticamente più attraenti o più belli a vedersi, ma magari intensamente trattati e contenenti un'alta concentrazione di sostanze potenzialmente tossiche. La perfezione non è nella natura e spesso si paga in modo salato. Occorrono campagne di sensibilizzazione e di informazione dei cittadini e delle stesse organizzazioni di categoria: un'intensa promozione della dieta mediterranea e dei principi nutrizionali che la compongono; l'attenzione su un uso corretto, ponderato e controllato di prodotti che dimostrino un impatto sullo stato di salute di tutti noi; intensificare la promozione e l'insegnamento della corretta alimentazione nelle scuole e il suo diretto rapporto con una corretta gestione dei territori e dell'ambiente circostante. Rispettare l'ambiente e utilizzare i prodotti delle nostre terre è un obbligo e un dovere nei confronti di tutti noi e delle generazioni future. Per quanto sopra esposto, il Gruppo MoVimento 5 Stelle voterà a favore della mozione n. 93 (testo

nuova finestra"). Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

grazie.

è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali; le scuole paritarie, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e della citata legge, sono abilitate, dunque, a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nel rispetto dei requisiti di qualità ed efficacia;

del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap*, l'organica costituzione di corsi completi; personale docente fornito del titolo di abilitazione, contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante. Le procedure per il riconoscimento, il mantenimento e la revoca della parità scolastica sono disciplinate nel dettaglio da un regolamento ministeriale. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del suddetto regolamento, con l'istanza di riconoscimento il gestore o il rappresentante legale deve dichiarare una serie di dettagliate disposizioni

la permanenza del possesso dei requisiti richiesti all'ufficio scolastico regionale competente; in caso di mancata osservanza delle prescrizioni richieste o di gravi irregolarità nella gestione l'ufficio scolastico regionale può revocare l'atto di riconoscimento della parità;

trasparenza e diffusione di informazioni, ai fini di garantire maggiore conoscibilità e trasparenza nella gestione di tali istituti (fermi restando le verifiche amministrative già previste dalla normativa vigente esposta); difatti, come già avviene per le scuole statali ai sensi della disciplina introdotta a partire dal 2013 dal cosiddetto "decreto Trasparenza", assolvendo le scuole paritarie private e degli enti locali ad una funzione di natura pubblicistica, pare opportuno assoggettare anch'esse al rispetto di taluni obblighi di pubblicità e trasparenza, con lo scopo prioritario di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"; durante l'*iter* di conversione in legge del cosiddetto "decreto Rilancio" (decreto-legge n. 34 del 2020) sono state aumentate di 150 milioni di euro, rispetto allo stanziamento originario disposto dal provvedimento, le misure di sostegno economico previste per l'istruzione paritaria (65 milioni) e il sistema integrato da zero a sei nel particolare, alle scuole "primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, viene erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nel 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19" Con questa mozione si intende impegnare il Governo a porre in essere le iniziative necessarie volte a tutelare i soggetti che assicurano questo importante servizio scolastico, ma sempre contemperando il primario interesse collettivo e pubblico. è necessario adoperarsi per l'estensione alle scuole paritarie, ai soggetti che gestiscono in via continuativa servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del del 2017, delle norme inerenti agli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni contenute nel decreto legislativo n. 33 del 2013, compatibili con le funzioni svolte da tali istituti, in particolare per quanto concerne l'organizzazione interna, la titolarità di incarichi di collaborazione e consulenza, il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute - con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio al relativo costo -, i dati relativi al personale non a tempo indeterminato, i dati sulla contrattazione collettiva integrativa, i documenti allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo, i beni immobili e la gestione dei patrimoni.

del contributo straordinario statale. Con questa mozione si intende sollecitare quindi il Governo ad impegnarsi fattivamente per permettere la realizzazione di un servizio scolastico efficace e qualitativo a coloro che possiedono e assicurano il rispetto di tutti i requisiti e le disposizioni di legge a tal fine previste.

le scuole paritarie e degli enti locali, come stabilito dalla legge 10 marzo 2000 n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», rappresentano, insieme e accanto alle scuole statali, una fondamentale componente costitutiva del «sistema nazionale il principio della «libertà di educazione» promanante dall'articolo 33 della Costituzione, che ha posto in capo a enti e privati il diritto di istituire, sul territorio nazionale, scuole e istituti di di educazione, in combinato disposto con i principi di sussidiarietà orizzontale e pluralismo istituzionale, nonché al parametro della virtuosa collaborazione tra iniziativa statale e privata, ha infatti determinato la configurazione di un «sistema scolastico integrato» caratterizzato da un giusto contemperamento tra l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati e lo svolgimento di attività di interesse generale; a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, e con particolare riguardo all'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, la legge qualifica e definisce le scuole paritarie come quelle istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, a partire dalla scuola dell'infanzia, cui è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico e che presentano, quali requisiti caratteristici, la corrispondenza agli ordinamenti generali dell'istruzione, la coerenza con la domanda formativa delle famiglie e la sussistenza di requisiti qualitativi e di efficacia, valutabile, quest'ultima, secondo parametri espressamente previsti dalla medesima legge che disciplina questo essenziale comparto complementare e sussidiario dell'erogazione di servizi di educazione e formazione nel nostro Paese; secondo un recente *report* elaborato dall'Ufficio Gestione patrimonio informativo e statistica del Ministero nell'anno scolastico 2018/2019 le scuole paritarie erano 12.564 e gli studenti frequentanti 866.805; in questo contesto, in particolare, la scuola dell'infanzia rappresenta il settore educativo in cui si concentra il maggior numero di studenti delle scuole paritarie: 524.031 bambini, distribuiti in 8.957 scuole, mentre 1.385 sono le scuole primarie, 622 le scuole di primo grado e 1.600 le scuole paritarie di secondo grado; oltre alla funzione sociale che questo segmento del sistema nazionale d'istruzione rappresenta, in termini di articolazione, orientamento e possibilità di scelta, da parte di famiglie e cittadini, tra opzioni didattiche e formative, alternative e diversificate, sia pur nella loro armonia e compatibilità con i principi costituzionali e nel quadro della normativa nazionale, assumono particolare rilevanza, specie nel contesto attuale di grave crisi economica, i volumi di attività registrati sul piano occupazionale: il sistema delle scuole paritarie occupa infatti 90.000 docenti e 70.000 dipendenti tecnici amministrativi, assicurando l'allocazione attiva di un considerevole bacino di professionalità riconducibile al settore dell'educazione e formazione; il settore scolastico è stato tra i primi ad essere pesantemente investiti dalla crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19: a decorrere dallo scorso 23 febbraio tutte le scuole e università di Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna venivano chiuse; dall'8 marzo in poi, con diversi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, la sospensione delle attività didattiche veniva gradualmente e progressivamente estesa a vaste aree del territorio nazionale, partendo da ulteriori 14 Province del Nord, sino a disporre, con il decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020, la sospensione delle attività didattiche in tutto il territorio nazionale. L'impatto di tale sospensione per le scuole paritarie, in particolare per la tenuta del sistema e la continuità delle attività del comparto, è stato dirompente. La riduzione di disponibilità finanziaria determinata dalla sospensione del versamento da parte dei fruitori delle rette scolastiche e delle compartecipazioni previste, in ragione dell'interruzione dei servizi venutasi a creare in seguito alle misure adottate, ha determinato l'emersione di fortissime difficoltà, specie in termini di equilibrio nella gestione finanziaria e di possibilità, in molti casi, di far fronte alle spese vive di gestori, quali ad esempio i canoni di locazione e tutto il mantenimento delle strutture e dei costi amministrativi. La persistenza della grave situazione ha portato, negli scorsi mesi, numerose associazioni rappresentative di queste strutture scolastiche, oltre a gestori e ad analisti delle politiche scolastiche, a lanciare un preoccupato grido d'allarme, evidenziando le stime e le proiezioni dell'anno scolastico venturo, nelle quali emergeva con chiarezza come il 30 per cento delle scuole paritarie, in assenza di interventi e chiari segnali di supporto, risultasse esposto al rischio concreto e attuale di chiusura. Tali istanze del mondo associativo e scolastico hanno faticosamente e comunque solo tardivamente trovato spazio nei diversi provvedimenti normativi adottati dal Governo nelle more della gestione dell'emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica, specie nella prima fase, nella quale pur risultava evidente - ed era già chiaramente delineato - il perimetro e l'entità del rischio concreto per tali strutture. Specularmente, nell'ottica della massima e più leale collaborazione che sin dall'inizio dell'emergenza ha caratterizzato l'atteggiamento del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia rispetto all'interesse nazionale a una gestione adeguata della crisi, erano stati già identificati, identificati, mediante numerose proposte emendative sistematicamente bocciate, i possibili percorsi risolutivi e le vie percorribili per assicurare un sostegno adeguato anche a questo comparto fondamentale per l'erogazione di servizi essenziali per i cittadini. Al riguardo giova ad esempio ricordare come del tutto carenti in tal senso risultassero le misure che il cosiddetto cura Italia prevedeva rispetto a tali istanze, nonostante fosse già noto l'impatto dirompente della crisi per le scuole paritarie e nonostante sin da allora, sia formalmente nelle Commissioni parlamentari, sia nel dibattito politico pubblico, il Gruppo Fratelli d'Italia ad ogni occasione utile avesse avanzato proposte concrete e puntuali quali l'istituzione di un fondo delle scuole paritarie o la previsione di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione per il periodo di sospensione dell'attività; nonostante ciò la previsione di misure di sostengo economico all'istruzione paritaria è confluita negli atti di Governo solamente con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; l'articolo 233 del testo del decreto varato dal Governo prevedeva uno stanziamento pari a 150 milioni di euro, per le scuole primarie e secondarie paritarie, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza

maggioranza di Governo, l'incremento è stato portato ad euro 300 milioni. Ciò a testimonianza della della fortissima sofferenza che questo importante segmento del sistema dell'istruzione italiana stava vivendo e vive. Noi chiediamo però al Governo impegni concreti sui tempi e sulle misure, visto il sopraggiungere dell'inizio del nuovo anno scolastico. al Governo di adottare tutte le iniziative necessarie ad assicurare anche nelle scuole paritarie un'ordinata e sicura ripresa dell'anno scolastico; ad assicurare, rispetto alle difficoltà di carattere finanziario ed economico, connesse alla sospensione delle attività didattiche, la continuità amministrativa e didattica delle scuole paritarie, anche mediante verifiche periodiche sui fabbisogni finanziari in relazione all'andamento futuro dell'emergenza epidemiologica; epidemiologica; a tutelare il bacino di professionisti occupati nel comparto delle scuole paritarie mediante ogni atto finalizzato a preservare i volumi e i livelli quantitativi e qualitativi di attività educativa, didattica e amministrativa prestata all'interno degli istituti; ad assicurare, in ultimo, un'adeguata tempistica dell'erogazione delle risorse stanziate, garantendo a famiglie e studenti, in modo omogeneo sul territorio nazionale, uniformità e parità di accesso e consentendo alle scuole paritarie all'inizio dell'anno scolastico, a settembre, di essere nelle condizioni di garantire una regolare ripresa delle attività didattiche e dei servizi educativi di competenza.

Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, siamo qua a difendere ancora una volta le scuole paritarie e l'indiscussa importanza nel sistema scolastico nazionale e nel nostro tessuto sociale. Sì, a difendere perché è un dato di fatto che nei numerosi provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare e contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19 non erano state inserite particolari misure di sostegno sia per le scuole paritarie che per le famiglie degli stessi studenti che le frequentano. Senza un intervento per tamponare la pesante perdita economica per le suddette scuole, causata dalla mancata corresponsione delle rette da parte delle famiglie, si sarebbe verificata la chiusura certa di moltissimi istituti scolastici paritari. Questo avrebbe comportato, oltre alla perdita del diritto di scelta educativa e di posti di lavoro, un notevole aggravio per i conti pubblici, per l'inevitabile passaggio degli studenti dagli istituti paritari a quelli statali, rendendo ancora più gravoso oltretutto il problema del reperimento degli spazi necessari per applicare le misure di distanziamento sociale. Solo negli ultimi giorni la maggioranza trasversale che si è concretizzata nella Commissione bilancio della Camera dei deputati sul cosiddetto decreto-legge rilancio ha portato ad aumentare i fondi destinati alle paritarie. Si parla ora di 300 milioni di euro contro i 65 milioni iniziali; 300 milioni che permetteranno di aiutare 12.000 istituti, 900.000 famiglie e 180.000 dipendenti tra docenti e operatori vari. Un risultato portato a termine grazie all'impegno delle forze di opposizione e dei cittadini che si sono spesi in prima persona nel richiedere questo intervento finanziario allo Stato. È così che il connubio tra opposizione e società civile ha trainato parte della maggioranza ad approvare questa modifica al decreto rilancio ed è stato così che quasi tutti i partiti - non tutti - hanno sostenuto la libertà di scelta educativa delle famiglie, ribadendo una volta per tutte che la scuola paritaria è pubblica al pari della scuola statale e che sono fondamentali entrambe nel sistema scolastico italiano. Avere il 30 per cento delle paritarie a rischio chiusura avrebbe significato lasciare scoperti 300.000

di quel 33 per cento di studenti delle scuole paritarie che avrebbero chiuso. Scongiurare la chiusura di molte scuole paritarie, quindi, con lo stanziamento di fondi aggiuntivi rispetto a quelli iniziali è stato assolutamente positivo, come è assolutamente importante ripartire con la scuola in presenza a settembre, perché se ciò non avvenisse si correrebbe il forte rischio di consegnare i ragazzi svantaggiati alla criminalità, specialmente nelle aree del Sud e ancora, di non riattivare il comparto 0-6 anni, così importante per le donne, altrimenti costrette a rinunciare al lavoro, specialmente nelle aree economicamente più fragili del Paese. A tutto questo dobbiamo aggiungere che, se è vero che una sana concorrenza tra le scuole alza il livello di qualità di tutto il sistema dell'istruzione, non dobbiamo però chiudere gli occhi davanti al *gap* tra i quasi 8.000 euro stanziati ogni anno per ciascuno studente delle scuole statali contro gli 800 euro che lo Stato stanzia per gli studenti delle paritarie. gli 8.466.064 studenti delle scuole statali e paritarie fosse applicato un costo *standard* di 5.500 euro, oltre a superare questo *gap*, facendo i conti lo Stato arriverebbe a risparmiare notevolmente. Pensiamo poi allo stanziamento del Governo di 29 milioni di risorse europee per istituire la *smart class* alle superiori, ovvero la fornitura di dispositivi elettronici per l'apprendimento *online.* A nostro avviso, questi stanziamenti dovevano essere destinati anche alle paritarie, visto che l'avviso pubblicato sul sito ministeriale recita di voler garantire pari opportunità e il diritto allo studio. Sotto un altro aspetto, va segnalata inoltre la grave discriminazione che investe gli alunni disabili: a fronte di un costo che lo Stato sostiene per loro, pari a 20.000 euro nelle scuole pubbliche statali, per i disabili che frequentano la scuola paritaria lo Stato destina 1.700 euro, lasciando l'onere a carico della famiglia o della scuola, con conseguenze ancora più pesanti per i meno agiati. In merito al distanziamento necessario per riprendere le lezioni a settembre, sarebbe un gravissimo errore ignorare la generosa offerta pervenuta dalle scuole paritarie, che hanno dato la disponibilità per l'utilizzo dei propri spazi in eccedenza per accogliere oltre un milione di alunni che non potranno rimanere negli istituti pubblici. Ma il tempo ormai è alla fine e anziché ricorrere a soluzioni di difficile attuazione, forse questa sarebbe la scelta migliore. Non so se quella parte di maggioranza tanto ostile alle paritarie, fino a definirle incostituzionali e addirittura meri diplomifici, si rende conto del fatto che le paritarie, in questo momento così delicato, possono fare la differenza. A noi non piace il modo di ragionare distruttivo e demonizzante che spesso viene assunto nei confronti delle scuole paritarie da una certa parte politica. Noi nelle scuole paritarie vediamo tutto il buono che possono portare soprattutto in questo momento di emergenza. Se sosteniamo le scuole paritarie, evitiamo di convogliare verso le scuole statali 300.000 studenti, ma anzi queste potrebbero addirittura accogliere quel 15 per cento di studenti delle scuole statali che, per garantire il distanziamento sociale, dovranno essere collocati altrove. In sintesi, a causa della compressione eccessiva dei tempi di esame del decreto-legge rilancio nel passaggio al Senato, non c'è stato modo di agire con ulteriori interventi a favore delle scuole paritarie. Per questo oggi invitiamo il Governo a proseguire con le azioni positive messe in campo a favore delle scuole paritarie, in linea con quanto segnalato dalle opposizioni, prevedendo la detraibilità integrale del costo delle rette versate dalle famiglie alle scuole paritarie nei mesi di sospensione della didattica, con tetto massimo di 5.500 euro, che è il costo standard di sostenibilità per allievo; prevedendo l'attribuzione alle famiglie di una quota pari al costo standard di sostenibilità per allievo, con una media di 5.500 euro, consentendo così la libera scelta educativa delle famiglie; prevedendo una concertazione tra Stato e Regioni per trovare la piena copertura dei docenti di sostegno, sull'esempio di quanto fatto dalla Regione Lombardia, che destina 3.000 euro per ogni allievo disabile che frequenta la scuola paritaria; inoltre, l'attivazione rapida di intese con le 12.564 scuole paritarie, visto che dispongono degli spazi necessari per raccogliere in sicurezza quel 15 per cento di studenti che, a causa del distanziamento, non troveranno posto nelle 40.749 sedi scolastiche statali. Con questa mozione vogliamo sollecitare il Governo. Abbiamo ancora poco tempo per decidere: settembre è dietro l'angolo, stiamo attenti a non riversare sui nostri studenti scelte sbagliate,

abbiamo investito risorse molto importanti, che hanno portato, perlomeno a livello dell'opinione pubblica, come mai forse era accaduto, a comprendere fino a che punto la scuola paritaria è parte integrante della scuola pubblica, insieme alla scuola statale. È un primo punto per cui perfino i nostri colleghi 5 Stelle, che forse all'inizio di questo dibattito sollevavano qualche eccezione sul fatto che la scuola paritaria potesse essere considerata tra le scuole pubbliche, riconoscono nella loro mozione esattamente il fatto che la scuola paritaria è parte integrante della scuola pubblica e in qualche modo fa sue

con la stessa passione da parte dei docenti, se non si fossero sentiti parte integrante di un unico sistema educativo nazionale. Detto questo, bisogna anche sottolineare un altro punto di questa mia mozione che, evidentemente, non essendo stata illustrata, potrebbe rimanere sotto silenzio. L'articolo 33 della Costituzione afferma che possono essere istituite scuole di tutti i tipi, generi e specie (fa riferimento agli istituti di educazione), senza oneri per lo Stato.

al sistema scolastico arrivano risorse concrete e positive. Non si tratta solo di risorse economiche; dalla scuola paritaria arriva soprattutto una cosa, che a mio avviso è la più importante di tutte ed è quella che giustifica, in premessa, il motivo per cui difendiamo questo tipo di scelta: di scelta: la libertà di educazione dei genitori, ma anche la libertà di insegnamento dei docenti. Nessuno di noi ignora come alla scuola statale siano arrivate molte volte suggestioni, stimoli, proposte, sperimentazioni che erano nate nell'ambito delle scuole paritarie. Questo mi sembra un fatto particolarmente interessante, se penso - ad esempio - al sistema tutoriale, ai licei linguistici, alle esperienze che poi sono confluite nel liceo coreutico e nel liceo musicale. La La scuola paritaria è stata sempre un laboratorio creativo di iniziative educative, che in ogni caso hanno fatto anche da punto di riferimento per la scuola statale.

del Ministero della pubblica istruzione, e considero pubbliche sia la scuola statale che la scuola paritaria, non vedo perché lo studente, portatore di un suo *budget*, riconosciuto corrispondente a un determinato costo *standard*, non possa scegliere dove andare a completare la propria formazione. Il sistema italiano rasenta una serie di piccole discriminazioni. Eppure già nell'anno 2000, quando era ministro Berlinguer, la legge n. 62 stabilì con estrema chiarezza quello che era già presente e accennato abbastanza chiaramente all'interno della Costituzione; e lo stabilì riconoscendo, da questo punto di vista, la parità di dignità ai titoli che venivano che venivano distribuiti attraverso la scuola paritaria. Tuttavia, mentre si riconosce allo studente una sua dignità, attualmente non se ne riconosce il costo; mentre si riconosce al titolo che viene fornito la parità di dignità (qualunque titolo: di scuola media superiore o di liceo, che io l'abbia preso all'Istituto Marcelline a Milano, al San Raffaele

un professore universitario di un'università statale può spostarsi tranquillamente e insegnare in una delle varie università (penso alla Cattolica, al Campus, al San Raffaele) e invece un professore di una scuola paritaria non può usufruire della medesima mobilità interna.

di studenti e di 12.000 scuole, ossia di una realtà complessa e composita molto ampia. Non capisco perché non debba essere questo il momento più opportuno affinché il Governo faccia sua un'istanza di equità, un'istanza contro la discriminazione. Noi chiediamo questo: chiediamo esattamente che i genitori abbiano il rimborso della loro quota, posto che pagano già le tasse, esattamente come le pagano i genitori delle scuole statali. Chiediamo che lo studente abbia autenticamente una libertà di scelta, spostandosi da una scuola all'altra, sulla misura di una scelta che riguarda il patto educativo. E lo chiediamo per dire basta, una volta di più, a a tutte quelle ingiustizie che vengono da lontano, perché - insisto - vengono dalla cattiva interpretazione di un articolo della Costituzione e dalla mancata corretta interpretazione della legge 10

offrendo modelli e servizi. Mentre il nostro commissario si dedica alla ricerca del banco ideale a costi veramente enormi (450 euro per ogni bambino per cui andrà ordinato un banco),

non voglio dire perfetto, ma sicuramente soddisfacente, sereno e capace di venire incontro ai bisogni delle madri, dei figli e anche degli stessi docenti.

in Italia sono 880.000 gli studenti che frequentano le oltre 12.000 scuole paritarie che svolgono servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale d'istruzione. Stando alle stime, circa il 30 per cento di queste realtà sarà in seria difficoltà e non potrà ripartire a settembre dopo la gestione dei mesi intensi di emergenza sanitaria. Le scuole paritarie non sono un accessorio. L'importanza degli istituti non statali in un sistema educativo integrato è stata sottolineata è stata sottolineata anche alla Camera dei deputati da Patrizio Bianchi, coordinatore del comitato di esperti voluto dal Ministro dell'istruzione per preparare la ripresa di settembre, che però potrebbe non vedere ai blocchi di partenza tante scuole paritarie, tra le principali vittime del *lockdown* imposto dall'emergenza coronavirus. Il diritto dei genitori nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli è un valore inestimabile che rende grande il nostro Paese ed è oltretutto riconosciuto nella Dichiarazione universale dei diritti umani. A vent'anni di distanza dall'approvazione della legge 62, che ha sancito l'appartenenza delle scuole paritarie al sistema nazionale di istruzione e ne ha riconosciuto il ruolo all'interno del servizio pubblico, la scuola paritaria paga oggi le difficoltà connesse alla gestione dell'emergenza Covid-19. Le scuole paritarie (vale a dire scuole senza fini di lucro) a oggi possono utilizzare soltanto la cassa integrazione in deroga per i dipendenti. È evidente che, venendo meno l'obbligo del pagamento delle rette da parte dei genitori a seguito della chiusura delle scuole, al netto delle spese per il personale sostenuto in parte dalla cassa integrazione in deroga prevista dal cosiddetto decreto cura Italia almeno fino al 31 luglio 2020, le altre risorse necessarie al mantenimento in vita delle scuole paritarie mancano del tutto. Senza un intervento propositivo dello Stato, circa un terzo delle scuole pubbliche paritarie sarà destinato a chiudere entro settembre ed è un vero peccato. peccato. Meno scuole paritarie, infatti, non vuol dire solo e semplicemente studenti che si trasferiscono nelle scuole pubbliche, ma significa più problemi per quanto riguarda l'ordine sanitario, più problemi per quanto concerne il discorso economico, e quindi più soldi più soldi che lo Stato dovrà versare. Secondo l'OCSE uno studente della scuola paritaria costa allo Stato 500 euro all'anno, mentre nel nostro Paese ogni alunno iscritto negli istituti pubblici costa 8.200 euro l'anno. Dunque, i 3.000 studenti in più che si iscriverebbero alla scuola statale, qualora dovesse fallire il sistema delle scuole paritarie - ci auguriamo che questo non avvenga mai - costerebbero alle casse pubbliche circa 2,3 2,3 miliardi di euro aggiuntivi. È da numeri inconfutabili che, ragionevolmente, il Governo, con buonsenso e lungimiranza, in un'ottica anche di risparmio economico, dovrebbe sostenere con forza il diritto alla libertà di scelta educativa, e piuttosto rinvigorire la presenza delle scuole paritarie nel nostro Paese. Non dimentichiamoci che molte scuole paritarie sono gestite da ordini religiosi, che si prodigano per consolidare una formazione improntata sul rispetto dell'educazione, sul rafforzamento dei valori umani e culturali. Chi di noi non ha avuto esperienze dirette o di familiari che hanno studiato in istituti religiosi? Non fanno parte di un passato dimenticato, ma restano tutt'oggi un'istituzione fondamentale per lo sviluppo sociale di tante famiglie. Mantengono viva una tradizione tuttora esistente del nostro Paese e, perciò, obliarle porterebbe porterebbe ad un pericoloso passo indietro. Le prime scuole cattoliche risalenti al 1500 sono nate, infatti, con lo scopo, oltre a quello di proporre un'educazione etica e religiosa, di riscattare il ceto medio-basso dall'ignoranza. Si tratta di un incontestabile merito che è bene ricordare ogni qualvolta si parli dei sistemi formativi, di libertà di scelta educativa delle famiglie, di finanziamento pubblico della scuola paritaria. Non da ultimo, le scuole paritarie di impronta cattolica fin dalle origini hanno promosso un'inclusione di giovani diversamente abili, sordi, muti, neuro diversi, ma anche di orfani, carcerati e poveri. Oggi più di allora il problema inclusione non può e non deve gravare solo sulla scuola pubblica, ma usufruire dell'aiuto concreto e lodevole delle scuole paritarie per promuovere modalità educative dignitose nel rispetto delle scelte. queste ultime settimane, al Senato e alla Camera si è sviluppato un importante dialogo con tutte le forze politiche, basato su un confronto scientifico e documentato, che ha consentito di chiarire le ragioni sulle quali si regge il sistema scolastico italiano; un sistema integrato perché composto da scuole pubbliche statali e scuole pubbliche paritarie. Presidente, penso che il rilancio della scuola italiana, e quindi la formazione di studenti critici e preparati, debba partire dalla centralità della formazione scolastica nell'agenda di Governo, attraverso un confronto puntuale delle misure di emergenza, abbattendo gli steccati ideologici e creando le condizioni perché la scuola sia davvero per tutti. Costruendo un dialogo propositivo tra tutte le parti potremmo portare il sistema scolastico italiano a un livello qualitativo più oggettivo e sicuramente migliore.

che leggo: «Impegna il Governo: a dare piena attuazione alla libertà di scelta educativa attraverso un sostegno delle scuole paritarie nell'ambito dei vincoli costituzionali e delle conseguenze normative

ad adoperarsi, attraverso provvedimenti di propria competenza, al fine dell'estensione alle scuole paritarie e ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017, delle norme inerenti agli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni contenute

delle risorse di cui all'articolo 233 del decreto-legge n. 34 del 2020, autocertificazione resa ai sensi del decreto del

la scuola pubblica paritaria, impegna il Governo a dare piena attuazione alla libertà di scelta educativa attraverso un sostegno adeguato delle scuole paritarie, nei limiti delle disposizioni costituzionali e delle normative vigenti

Signor Presidente, fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria Fratelli d'Italia sta esprimendo la sua preoccupazione per l'intero mondo della scuola italiana purtroppo, dobbiamo registrare, anche in questa occasione, con la contrarietà secca del Governo alla nostra mozione, un atteggiamento di chiusura totale. totale. Si approssima l'inizio del nuovo anno scolastico, ma il Governo sembra non guadagnare consapevolezza rispetto agli effetti agli effetti delle scelte sbagliate e tardive che vengono intraprese. Fin dai primi giorni ci ci siamo concentrati anche sull'aspetto che riguardava le scuole paritarie perché riteniamo che sia un mondo che vada assolutamente rispettato. Le scuole paritarie non sono figlie di un Dio minore: rappresentano uno spaccato dell'istruzione italiana assolutamente imprescindibile, come già detto anche anche dai colleghi dei partiti alleati del centrodestra. Sul cura Italia ci siamo però, visti rinviare alle misure del decreto rilancio.

economici non hanno dispiegato alcun nessun effetto. Nessuno le ha viste. Quindi il nostro intento, anche attraverso la mozione, era quello di rappresentare un ulteriore pungolo, facendo comprendere che gli imprenditori di questo settore non hanno la possibilità di occuparsi delle misure misure per garantire la sicurezza. Quindi, quella mortalità che veniva riferita da tutte le mozioni dei Gruppi di opposizione è destinata a concretizzarsi e ad aumentare. E cosa ne sarà degli alunni, delle famiglie,

Vorrei ancora sperare in un guizzo di consapevolezza, ma mi rendo conto che da una parte c'è una furia ideologica contro le scuole paritarie e, dall'altra, c'è l'imbarazzo per un accordo politico di maggioranza per fare in modo che intervenga la ragione. Per questo non possiamo fare altro che esprimere, oltre al voto favorevole alla nostra mozione, il voto favorevole di Fratelli d'Italia alle mozioni di Lega e di Forza Italia. Allo stesso modo avremmo condiviso anche l'impegno della mozione di Italia Viva, ma è evidente che la riformulazione che è stata proposta dal Governo

Presidente, perché sono importanti le scuole paritarie? perché, con la loro presenza e la loro attività, assicurano un diritto semplicemente fondamentale in democrazia, che è quello della libertà educativa e, cioè la facoltà per le famiglie di poter garantire ai loro figli la formazione che meglio credono: è questo il senso e la ragione per la quale da diversi anni si conducono battaglie tese a sostenere le scuole paritarie nel nostro Paese, anche dopo che una legge dello Stato ha parificato, appunto, le scuole paritarie con quelle statali, definendo in maniera davvero lungimirante entrambe queste due tipologie «servizio pubblico». Non è bastata però una legge per parificare tutto questo e per garantire pari dignità, pari trattamento e pari attenzioni da parte dello Stato. Credo e crediamo che la strada sia ancora lunga. Oggi però ci troviamo di fronte ad una condizione molto particolare, che è quella determinata dalla pandemia, che ha scatenato i problemi che ben conosciamo;

buchi nei bilanci delle scuole paritarie, dovute al fatto che numerose famiglie non hanno più potuto pagare le rette per mancanza delle risorse, perché i genitori sono andati in cassa integrazione e in alcuni casi hanno addirittura perso il posto di lavoro. Ebbene, con il decreto rilancio abbiamo fatto sicuramente

Viva. La situazione resta tuttavia critica e non è certo che le risorse messe in pista possano bastare ad assicurare alle scuole paritarie la sopravvivenza a settembre. Guardate che non è una questione che riguarda soltanto queste scuole perché, nel momento in cui quelle scuole dovessero chiudere, i ragazzi che le frequentano dove pensate che vadano?

ma restiamo profondamente convinti che il percorso debba prevedere altri interventi da parte dello Stato e altri riconoscimenti, proprio perché proprio perché crediamo fermamente che la democrazia veda il proprio fondamento nella libertà data alle persone di poter compiere delle scelte. La libertà di scelta delle famiglie è una questione che va difesa nel miglior modo possibile. Permettetemi di ricordare che proprio oggi, alla Camera dei deputati, è stato approvato in maniera unanime il primo tassello del *family act*, il riconoscimento di un *bonus* dedicato ai figli: una scelta importante che mi auguro venga presto anche qui in Senato per poter essere discussa e valorizzata, che consente alle famiglie di poter avere un reale supporto e un reale sostegno per poter crescere i loro figli. Anche poter supportare meglio le famiglie nella scelta che riguarda la scuola con una maggiore detraibilità delle risorse delle risorse spese per l'iscrizione dei figli alla scuola paritaria andrebbe in questa direzione. Avremo certamente modo di riparlarne, anche con il decreto-legge rilancio *bis*, che sarà proposto dal Governo dopo che avremo votato il prossimo scostamento di bilancio. Avremo modo di tornare su tali questioni, ma per Italia Viva - e sono certo non solo per noi di Italia Viva - il tema delle paritarie resta importante; il tema delle famiglie è fondamentale. Il ministro Bonetti oggi oggi porterà a casa un risultato importante per il Paese e non per un partito. Noi continueremo a lavorare su questa strada e in questa direzione, ritenendo che le scuole paritarie svolgono una funzione importante non solo nel sistema educativo della nostra Nazione, ma anche nel quadro della nostra democrazia, consentendo alle famiglie di poter esercitare una libertà di scelta in ambito educativo. [DE

Signor Presidente, colleghi, vorrei ricordare innanzitutto a me stessa, sentendo il dibattito di oggi e la discussione svolta anche nel merito di ogni singola mozione, la parità scolastica compie adesso vent'anni: fu approvata il 10 marzo del 2000. prodotto? Ha prodotto il fatto che le scuole paritarie sono state inserite all'interno del sistema nazionale d'istruzione, in forza del servizio pubblico che è stato

la scuola paritaria ha tratto molto giovamento sul fronte della qualità dell'offerta proprio dal riconoscimento della parità scolastica,

- che per il sistema dei nidi. E, quindi, riguarda tutto il sistema, ma ancor di più riguarda il sistema

Ora, noi lo diciamo con chiarezza: siamo piuttosto scettici - per la verità lo siamo sempre stati - rispetto alla defiscalizzazione delle rette,

ma anche vigilanza da parte di tutte le istituzioni sulle risorse e sui sistemi di garanzia, di trasparenza di accesso al sistema, che a nostro avviso fanno bene alla scuola paritaria. Nell'annunciare per quanto ci riguarda il voto favorevole sulla mozione a prima firma della

molto importante per tutti noi, per la società, per i milioni di docenti, di famiglie e di ragazzi e ragazze coinvolti.

di crescita collettiva e di scambio tra insegnanti e ragazzi, è la scuola in presenza. Su questo dobbiamo continuare a mobilitarci

Signor Presidente, colleghi, per il Partito Democratico le scuole paritarie sono un elemento essenziale nel sistema di istruzione del nostro Paese.

di scelta educativa dei genitori per i figli e vi sono ancora disparità nel sostegno alle due opzioni del sistema. Esistono ostacoli per cui le famiglie non sempre hanno la possibilità di scegliere liberamente la strada formativa per i propri ragazzi. Purtroppo questo tema è stato terreno di scontro ideologico nella società e in Parlamento, uno scontro che ha impedito di guardare alla questione in modo sufficientemente corretto. Berlinguer, nel 2000, con la legge n. 62, ha riconosciuto un principio costituzionale, inserendo le scuole paritarie nel sistema di istruzione nazionale. Non dimentichiamolo: quello delle scuole paritarie è un servizio che passa dal riconoscimento della libertà di scelta per le famiglie e un riconoscimento che la spesa fatta per l'istruzione per l'istruzione dei figli ha un valore pubblico, sempre. È bene inoltre ricordare che il sistema delle scuole paritarie è scuola a tutti gli effetti, ponendosi come obiettivo prioritario proprio l'espansione dell'offerta formativa, e conseguentemente è risposta alla domanda di istruzione dell'infanzia e lungo tutto l'arco della vita. Per troppi anni queste scuole sono state considerate scuole di serie B, non qualificate, o troppo spesso scuole facilitatrici; ma non è così. Può esserlo in qualche caso; ma non è così in tutti i casi, anzi, ci sono casi di vera eccellenza. Oggi il sistema italiano senza le scuole paritarie sarebbe più povero di qualità e di pluralismo, soprattutto per quanto riguarda il sistema 0-6. È un dato oggettivo che le scuole dell'infanzia paritarie spesso sopperiscono alla carenza dei servizi offerti in diversi Comuni. Se è evidente che la scuola paritaria è fondamentale nel nostro sistema di istruzione, abbiamo certamente la necessità di affermare sempre di più il principio di qualità, che vale per ogni scuola, distinguendo ciò che funziona da ciò che non funziona, il servizio svolto da chi si impegna per il continuo miglioramento dell'offerta formativa e chi non investe abbastanza nel rinnovamento dei servizi educativi. Ma nel frattempo, in questo momento, dobbiamo impedire che il sistema delle scuole paritarie collassi sotto i colpi della crisi. In questo senso l'aumento a 300 milioni di euro nel decreto rilancio per il sostegno alle scuole paritarie, messe a dura prova dall'emergenza Covid, è stata una scelta lungimirante da parte del Parlamento. Ora è necessario che questi fondi arrivino in tempi rapidi alle istituzioni scolastiche, perché molte rischiano davvero di non riaprire noi non possiamo procrastinare i finanziamenti stanziati nel decreto rilancio. La pandemia infatti ha avuto effetti molto duri su questo settore, soprattutto sul segmento dei servizi nella fascia 0-6, come nidi e materne, che da quattro mesi non ricevono più rette dalle famiglie. Sono già 70 le scuole paritarie che hanno dichiarato fallimento l'ultima ieri a Roma - e 3.082 gli alunni ai quali dovrà essere trovata una nuova collocazione nelle scuole statali per la ripresa di settembre, con un nuovo costo a carico della collettività di oltre 26 milioni di euro. Anche a sostenere queste situazioni dovranno essere dedicati i 300 milioni del decreto rilancio, di cui 180 per l'infanzia e gli asili e 120 per le scuole della primaria e secondaria di secondo grado fino a diciotto È chiaro che, proprio perché è necessario che le scuole paritarie siano riconosciute finalmente come una parte integrante e significativa del sistema scolastico, occorre la necessaria trasparenza in virtù del ruolo che svolgono. Con la legge n. 107 del 2015, infatti, sono già stati fatti necessari passi avanti grazie al piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il pieno riconoscimento della parità scolastica: un'attività diretta a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Abbiamo cioè iniziato a individuare la cosiddetta piramide rovesciata, che alcuni conoscono bene: gli alunni che iniziano nel primo anno di corso aumentano progressivamente fino a esplodere nell'ultimo anno. Stanno facendo questo controllo perché noi crediamo nel sistema di istruzione pubblico, che si compone di scuole statali e non statali, ma allo stesso modo non vogliamo diplomifici. Si utilizzino le norme della parità scolastica per effettuare vera scuola e istruzione di qualità. Per questo, grazie a quella legge, sono già aumentati i controlli nelle scuole; per esempio tutte le paritarie, anche ai sensi della legge n. 62 del 2000, hanno già l'obbligo di redigere il bilancio con la relativa nota illustrativa, cioè la riclassificazione del bilancio fiscale, dove si dà evidenza ai contributi pubblici ricevuti, alle rette e ai costi. Se i controlli accertassero che ci sono scuole che non presentano tale bilancio, andrebbe revocata la parità. Questo è solo un esempio per dire che le norme ci sono e vanno applicate. Nel frattempo però è fondamentale dare tutto il sostegno necessario alle scuole paritarie soprattutto ora che patiscono in modo drammatico gli effetti della crisi, ricordando che in Italia ci sono 880.000 studenti che frequentano più di 12.000 scuole paritarie e che eventuali chiusure comporterebbero, oltre all'impoverimento dell'offerta formativa e alla limitazione della libertà di scelta, cui accennavo prima, un impatto negativo sui conti della scuola statale, che avrà minori risorse a disposizione. Riassorbire questi studenti costerebbe migliaia di euro per la scuola statale e renderebbe ancora più difficoltosa la già complessa riapertura di settembre. per cento dell'offerta è rappresentato dai nidi, dalle scuole dell'infanzia paritarie private del terzo settore, riconosciuti dal decreto Si tratta di realtà che offrono un servizio integrativo fondamentale senza il quale bambini e famiglie non potrebbero beneficiare del diritto all'educazione precoce, che tutti sappiamo quanto sia importante. Non solo, ma parliamo di cooperative sociali e imprese, spesso al femminile, che impiegano migliaia di educatori, educatrici e altro personale, e il sistema deve proseguire sulla via dell'integrazione e del riconoscimento. Noi crediamo nella necessità di ampliare l'offerta formativa, di tutelare la libertà di scelta, di dare lavoro a migliaia di educatori e docenti. In questo senso ben vengano le operazioni di trasparenza che servono a isolare le realtà che non fanno il loro lavoro, consentendo invece a chi svolge il servizio pubblico essenziale con competenza, qualità e risultati risultati anche eccellenti, di ottenere risorse e sostegno. In conclusione, la nostra Costituzione, all'articolo 33, garantisce in modo fondamentale il diritto all'istruzione pubblica, quindi statale e paritaria. È evidente dunque come il tema dell'attuazione della Costituzione riguardo al pluralismo scolastico sia un elemento chiave e che la politica debba offrire una risposta adeguata nel rispetto della normativa vigente per costruire ed arricchire ogni comunità educante.

Signor Presidente, Governo, colleghi, vorrei che fossimo tutti profondamente consapevoli dell'importanza dell'argomento che stiamo trattando, *in primis* il Ministro dell'istruzione, che oggi, ovviamente, non è presente. Legge 10 marzo 2000, n. 62, ministro dell'istruzione Luigi Berlinguer, per capirci; sono passati venti anni dal momento in cui si è sancita per legge l'appartenenza delle scuole paritarie al sistema nazionale di istruzione che ne ha riconosciuto il ruolo all'interno del servizio pubblico. Eppure ancora oggi, anche dopo che il sistema dell'istruzione statale paritario ha retto allo *tsunami* di una pandemia, si fanno ingiuste distinzioni all'interno del sistema pubblico integrato dell'istruzione. all'interno del primo decreto di sostegno alla fase due, il cosiddetto decreto cura Italia, poco o nulla era stato previsto per le scuole paritarie, se non poche risorse destinate alla pulizia dei locali, all'acquisto di dispositivi di protezione e igiene personali, a riprova del completo disinteresse di una parte, a quanto pare determinante e condizionante, per la prima e seconda maggioranza al Governo con il *premier* Conte. La voce di Forza Italia si è alzata fin dal primo giorno affiancata poi dall'intero centrodestra e, a seguire, anche dai Gruppi di maggioranza, ad eccezione del MoVimento 5 Stelle che, al contrario, non ha mai perso occasione, non solo per non fare nulla, ma per essere il primo detrattore di una gamba essenziale del sistema scolastico italiano. La voce dei Gruppi di maggioranza si è sentita, ma lo sforzo è stato immane anche per loro - PD, Italia Viva - per riuscire a far passare almeno un trasferimento di risorse dignitoso contro le barricate alzate dal MoVimento 5 Stelle. La scuola italiana non merita questo, soprattutto in un momento come questo. La scuola non merita un Governo sostenuto da una maggioranza che ha perso tempo con dissidi interni, tenuta in scacco da una voce sola fuori dal coro, piuttosto che compattarsi e creare un'alleanza *bipartisan* anche con la minoranza per il per il bene supremo del sistema dell'istruzione nella sua interezza, che rappresenta l'ossatura di un Paese. Ma noi non ci arrendiamo e con questa mozione desideriamo provare ancora ad avviare, siglare e consolidare l'alleanza virtuosa tra scuola pubblica statale e scuola pubblica paritaria. Desideriamo provare ancora a dare la spallata definitiva, una volta per tutte, tutti insieme, allo steccato ideologico sulla libertà di scelta educativa che fino ad oggi si è levato altissimo, facendo prevalere sempre all'interno della stessa maggioranza l'ala statalista che ha schiacciato sotto i piedi i concetti di libertà espressi in Costituzione e che ancora mette a rischio collasso la stessa scuola statale. Se il suono della prima campanella non vedrà aperti prima di tutto i cancelli del buonsenso, dando la possibilità alle famiglie di accedere alla scuola statale o paritaria senza preclusioni reddituali, la scuola statale si ridurrà a peggiorare sempre di più, perché oltre a precludere una sana e virtuosa competizione, stimolo al miglioramento, verrà precluso il regolare avvio delle lezioni e allora sì Le scuole paritarie (non private, ovvero il cui valore legale del titolo è il medesimo della scuola statale e i cui docenti devono essere in possesso di regolare abilitazione) vivono oggi del pagamento delle rette, quelle rette che molte famiglie, in tempo di emergenza Covid non sono riuscite e non riusciranno più a pagare e per le quali abbiamo chiesto tra l'altro a più riprese, presentando emendamenti a ogni decreto utile, almeno la detrazione fiscale totale, visto che le famiglie i cui figli frequentano la scuola paritaria pagano anche le tasse per la scuola statale. Ma rigidi e intransigenti, a costo di far pagare agli studenti il prezzo di un principio statalista oltre ogni senso logico. Vorrei chiedere con tutto il cuore alla senatrice Granato, sempre così agitata e pronta a scattare quando solo si nomina la scuola paritaria qui in Senato, da cosa le deriva tutta questa preoccupazione, che cosa è successo nella sua vita scolastica, come in quella di molti colleghi del MoVimento 5 Stelle, un moto di repulsione così viscerale verso scuole che hanno la sola colpa di avere metodi o indirizzi pedagogici diversi, ma soprattutto sistemi di gestione non statali, tanto da presentare una mozione che da un lato apre al riconoscimento della funzione pubblica della scuola paritaria e anche alla libertà di scelta educativa - questo ci fa molto piacere ed è un momento storico, probabilmente - mentre dall'altro chiede verifiche e controlli in maniera, a nostro avviso, pleonastica, perché i controlli esistono già, pena la revoca della parità. Questo dovrebbe saperlo, perché non dobbiamo dimenticare anche l'enorme patrimonio umano e di strutture delle scuole paritarie - è stato ripetuto da tutti - nelle quali lavorano 180.000 tra docenti e operatori scolastici, in 12.000 sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, patrimonio umano e strutturale che potrebbe rivelarsi utilissimo per agevolare la ripresa della scuola tutta. Come suggerito da CISM e USMI, le scuole paritarie, con la loro maggiore flessibilità, potrebbero cominciare ad accogliere almeno una parte degli alunni più piccoli durante le settimane iniziali della ripartenza, quando i genitori al lavoro saranno in difficoltà con la gestione dei figli, per garantire quel distanziamento sociale che comporterebbe magari per alcune strutture statali lavori anche di edilizia e l'impossibilità di accogliere tutti gli studenti. Si chiama patto educativo, si chiama patto civico, si chiama sussidiarietà ed è la grande alleanza che noi sogniamo. In caso contrario, difficilmente il sistema dell'istruzione potrà assolvere ai propri compiti, perché se le scuole paritarie non saranno messe in condizione di superare questa crisi e di continuare

continuare a sostenere costi fissi che lieviteranno a causa delle nuove regole del distanziamento sociale. Peraltro mi fa sorridere pensare a tutto questo gran da fare per tenere i ragazzi separati a scuola, anche perché, come ho già detto, scuola e distanziamento sociale

(quasi 100) scuole paritarie sono chiuse, che le statali sono piene: dove andranno questi studenti? Dove andranno questi bambini con la scuola paritaria chiusa e la scuola statale piena? Apro una parentesi a questo punto per mandare un messaggio da donna di scuola meno giovane, con una sola laurea, con una sola abilitazione, al ministro Azzolina, donna giovane di scuola con due lauree, per darle il mio parere su cosa fa di un Ministro un buon Ministro, cosa fa di una persona, la persona giusta al posto giusto: essere umili e assumersi le proprie responsabilità. L'umiltà soprattutto salverà il mondo: ascoltare, studiare ed essere presenti. Personalmente, dopo tanti anni di esperienza scolastica, politica, amministrativa, mi tremerebbero le vene ai polsi se mi venisse affidato un incarico di incredibile responsabilità come il suo, sapendo bene che non si viene giudicati per il genere, per l'età i titoli, ma per l'adeguatezza o meno al ruolo e alla funzione. *(Applausi)*. Per questo forse oggi io sarei stata presente in quest'Aula ad ascoltare un dibattito così importante. Le do un consiglio a distanza, signor Ministro. Dica al commissario Arcuri di trovare strade più semplici e più economiche per far ripartire la scuola: la strada della fiducia in chi sa come si fa; gli dica di usare i soldi pubblici per lasciar fare ai dirigenti, agli insegnanti, agli operatori della scuola. La scuola ha bisogno di spazi, di docenti stabilizzati, di sostegno per i servizi di trasporto, non di banchi assurdi. Non c'è bisogno di complicare ulteriormente le cose, di sprecare risorse, visto che sono

Non si possono prendere in giro i luoghi sacri dell'educazione che oggi sono ancora chiusi; chiediamo di smetterla di rimpallare le responsabilità ai dirigenti e al territorio, quindi ai Comuni. È una guerra tra poveri, mancano meno di due mesi alla riapertura della scuola e uno di questi mesi è agosto, quindi settembre è domani. Chiedo a tutta l'Assemblea di sostenere questa mozione e tutte quelle a sostegno delle scuole paritarie. Lo chiedo a tutti e mi rivolgo al PD in particolare; ricordo infatti che proprio il ministro Fedeli aprì per prima il tavolo sul costo *standard* e che fu il ministro Berlinguer l'estensore della legge sulla parità. Vorrei infatti che in nome della libertà di pensiero, che sta alla base di ogni rivoluzione culturale, noi facessimo la vera rivoluzione e la vera riforma della scuola, con l'introduzione del costo *standard* per studente: occorre dare i soldi direttamente alle famiglie perché possano scegliere, senza differenza di casta, di censo, di reddito, di patrimonio, senza preclusioni, innescando un sistema di reale equità sociale, senza contare il risparmio per le casse dello Stato. Nel frattempo, occorre introdurre la detrazione fiscale totale delle rette, almeno quelle in attesa, per non far scappare le famiglie dalla scuola paritaria. Se il primo rilancio non partirà dalla scuola, a cascata fallirà tutto il resto. Dimostriamo di avere le teste ben fatte, come voleva Montaigne, e non solo ben piene. Facciamo diventare questa mozione la mozione di tutti e, per una volta, rendiamo una riforma della scuola veramente rivoluzionaria: una riforma vera, moderna, definitiva, concreta. Rovesciamoli, i tavoli! Grazie, suor Anna Monia per tutto il lavoro che ha fatto per noi. nei provvedimenti del Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica non erano state inserite adeguate misure di sostegno per le scuole paritarie, né per le famiglie degli studenti che le frequentano. La conseguente chiusura di parte degli istituti paritari avrebbe comportato, oltre alla perdita del diritto di scelta educativa (e di posti di lavoro), un notevole aggravio per i conti pubblici, per l'inevitabile passaggio degli studenti dagli istituti paritari a quelli statali, rendendo, tra l'altro, ancora più problematico il reperimento degli spazi necessari per applicare le misure di distanziamento sociale. Solo da poco una maggioranza trasversale, concretizzatasi in Commissione bilancio alla Camera sul decreto rilancio, ha portato ad aumentare i fondi per aiutare le famiglie colpite economicamente dal Covid-19, che si vedono impossibilitate a proseguire nel pagamento della retta delle scuole paritarie: 300 milioni di euro, che permetteranno di aiutare 12.000 istituti, 900.000 famiglie, 180.000 dipendenti, tra docenti e operatori. L'iniziativa è nata per l'impegno delle forze di opposizione e dei cittadini, che si sono spesi in prima persona nel chiedere l'intervento dello Stato. Opposizione e società civile hanno trainato parte della maggioranza fino ad approvare una modifica al decreto rilancio. È così che, per una volta, la quasi totalità delle forze politiche ha sostenuto la libertà di scelta educativa delle famiglie, ribadendo che la scuola paritaria è pubblica, al pari della scuola statale, ed entrambe sono fondamentali per il sistema scolastico nazionale che è, appunto, plurale. Perdere il 30 per cento delle scuole paritarie - questo era il rischio - avrebbe significato lasciare scoperti 300.000 studenti, con conseguenze devastanti per lo Stato, visto il costo aggiuntivo prossimo ai 2,5 miliardi di euro. In piena emergenza Covid-19, le 40.000 scuole statali non avrebbero potuto accogliere l'utenza delle 13.000 paritarie e la mancata ripartenza della scuola avrebbe voluto dire consegnare i ragazzi delle aree disagiate alla criminalità, mentre la mancata riattivazione nel comparto da zero a sei anni avrebbe costretto molte mamme a rinunciare al lavoro. A livello internazionale è ampiamente dimostrato che una sana concorrenza delle scuole alza il livello qualitativo dell'intero sistema dell'istruzione. Devono perciò essere attivati i costi *standard*, statale costa non meno di 5.500 euro l'anno, ma lo Stato ne destina solo 500 per gli alunni delle scuole paritarie. E sono destinati esclusivamente alle scuole statali 29 milioni di euro di risorse europee per istituire le *smart-class* alle superiori, ovvero la fornitura di dispositivi elettronici per l'*e-learning*. In questo modo sono stati esclusi 110.000 studenti delle scuole paritarie di secondo grado, sebbene l'avviso pubblicato sul sito ministeriale reciti di voler garantire le pari opportunità e il diritto allo studio. Va anche segnalata la grave discriminazione che investe gli alunni disabili, che, a fronte della spesa di 20.000 euro che lo Stato sostiene per loro nella scuola statale, per quelli che frequentano la paritaria prevede solo 1.700 euro, di fatto lasciando l'onere a carico della famiglia o della scuola, con conseguenze particolarmente pesanti per le famiglie meno agiate. Considerato che, per una soluzione adeguata alla necessità di maggiori spazi ove ubicare nuove classi che occorrerà formare per rispondere alle esigenze di distanziamento, le scuole paritarie hanno dato disponibilità all'utilizzo dei propri spazi in disuso per accogliere oltre un milione di alunni che non potranno essere accolti negli istituti pubblici, sollecitiamo chi di dovere a non ignorare tali proposte. Con la nostra mozione impegniamo, inoltre, il Governo a prevedere la detraibilità integrale del costo delle rette versate dalle famiglie alle scuole pubbliche paritarie nei mesi di sospensione della didattica, fino a 5.500 euro, che è il costo *standard* di sostenibilità per allievo, a valutare l'opportunità di attribuire alla famiglia una quota pari al costo *standard* di sostenibilità per allievo, consentendo così la libera scelta educativa delle famiglie. a promuovere una concertazione tra Stato e Regioni, per trovare la piena copertura del docente di sostegno, sull'esempio di quanto fatto dalla Regione Lombardia che destina 3.000 euro per ogni allievo disabile che frequenta la scuola paritaria; Per quanto riguarda le mozioni delle altre forze politiche, mi pare esse confermino la convergenza emersa alla Camera dei deputati e di questo non possiamo che compiacerci. In controtendenza, come al solito, è il MoVimento 5 Stelle, che nel suo documento chiede di estendere alle scuole paritarie le norme inerenti agli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni, in particolare per quanto concerne l'organizzazione interna (articolazione uffici e organigramma); la titolarità di incarichi di collaborazione o consulenza (con estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, *curriculum vitae* e compenso erogato); il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute (con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo); i tassi di assenza; i dati relativi al personale non a tempo indeterminato; i provvedimenti adottati (quale, ad esempio, quello di assegnazione dei docenti alle classi); i dati sulla contrattazione collettiva integrativa; i documenti allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; i beni immobili, oltre alla gestione del patrimonio. In sostanza, i grillini chiedono di impegnare il Governo a richiedere a soggetti che restano privati, pur erogando un servizio di pubblica utilità, tutta una serie di adempimenti tipici degli organi pubblici e degli enti che vedono la massiccia partecipazione dello Stato, delle Regioni o degli enti locali in termini sia di finanziamento, che di gestione ordinaria, come avviene per esempio nelle municipalizzate. In base al principio della libertà di insegnamento, invece, le scuole paritarie possono ricevere sussidi quando ne ricorrono le condizioni, ma sono autonome nella loro organizzazione,

Signor Presidente, colleghe e colleghi, con la mozione che abbiamo presentato intendiamo perseguire due obiettivi. Il primo riguarda l'equiparazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza tra scuole paritarie e scuole statali. al secondo, si chiede al Governo un impegno a verificare che il fondo di 300 milioni di euro conferito con il cosiddetto decreto rilancio a beneficio delle paritarie, a titolo di indennizzo delle rette non riscosse, vada effettivamente a colmare questa perdita subita. I soldi pubblici utilizzati per le misure di ristoro sono a debito e le istituzioni hanno il compito di vigilare sul buon fine di quest'operazione, che deve risultare meramente risarcitoria, posto che il finanziamento diretto e indiretto delle scuole paritarie private per i segmenti obbligatori è costituzionalmente inammissibile, diversamente da quanto propongono altre mozioni, come ad esempio quella a prima firma della senatrice Bernini, con cui addirittura si chiede uno sgravio contributivo pari al 100 delle rette versate per le famiglie degli studenti iscritti alle paritarie. Al primo punto della nostra mozione si chiede alle scuole paritarie pubbliche e private l'osservanza rigorosa delle prescrizioni in merito agli obblighi di pubblicità e trasparenza valevoli per le scuole statali, essendo queste abilitate a rilasciare punteggio agli insegnanti valevole nelle graduatorie pubbliche e titoli di studio aventi valore legale agli studenti. Siccome, nonostante le regole apparentemente stringenti e i requisiti previsti dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, che regolamenta la parità scolastica, la vigilanza ai suddetti enti da parte degli uffici scolastici regionali, per endemica carenza di personale ispettivo, è difficoltosa tanto da risultare quasi impossibile, si rende indispensabile estendere gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per le pubbliche amministrazioni anche alle paritarie private e pubbliche, onde consentire a chiunque di verificare, anche da remoto, il possesso e il mantenimento dei requisiti previsti per la parità scolastica da parte di questi enti, fermi restando ovviamente gli obblighi di verifica da parte dell'amministrazione, come da normativa vigente. Molte di queste scuole - certamente le pubbliche paritarie, ma anche le paritarie private per il segmento infanzia e nidi, per esempio ricevono finanziamenti da parte degli enti locali sulla quota loro spettante dei trasferimenti statali. È dunque indispensabile che ciascuna di esse si doti di sito *web* in cui siano resi noti - come avviene per la scuola statale - organigramma, bilancio, decreti di nomina del personale a tempo determinato e indeterminato, assegnazione dei docenti alle classi, orario didattico, piano triennale dell'offerta formativa, organi collegiali e loro delibere, regolamento d'istituto, patto educativo di corresponsabilità, registro elettronico delle presenze e delle attività. Tutto questo ai fini di tutelare famiglie e studenti, garantendo loro una effettiva equiparazione del servizio e per tutelare i docenti dal lavoro sommerso, addirittura nero, che la legge n. 62 del 2000 non è riuscita a scongiurare. Infatti, fatta la legge, trovato l'inganno: gli obblighi retributivi conformi al contratto collettivo nazionale vengono in alcuni casi elusi con vari espedienti che ci sono stati da più parti segnalati anonimamente. Siamo venuti a conoscenza di episodi in cui la retribuzione effettuata ai docenti a mezzo di conto corrente bancario viene seguita da restituzione in contanti di parte o di tutto lo stipendio trasferito. Questa condizione viene posta all'accettazione dell'incarico al docente, pena il licenziamento, con conseguente perdita del punteggio. Oltre a ciò, ci è stata segnalata la pratica di attribuire ai docenti un *surplus* di lavoro che arriva anche fino al 40 per cento dell'orario settimanale extra non retribuito, con mansioni anche fuori contratto. Si parla di docenti addetti anche alla pulizia degli ambienti di lavoro, per fare un esempio. Se ciò avviene è perché lo Stato non riesce a esercitare la vigilanza che dovrebbe su questi enti, e i docenti non denunciano gli abusi, perché l'erogazione del punteggio stimola la connivenza tra datore di lavoro e sottoposto, e poiché sanno che, se vengono licenziati, dietro di loro, sempre per il punteggio - nel miraggio di farlo valere per un posto nelle scuole statali - c'è la fila. Troppe opacità sul sistema scolastico privato paritario, del quale alcuni fanno l'elogio ignorando o fingendo di ignorare ciò che spesso si cela dietro. *Fiat lux*: c'è bisogno di mettere a sistema un regime di trasparenza che consente a chiunque, a tutti i cittadini, di verificare gli atti ed eventualmente segnalare incongruenze nella gestione di queste scuole. Solo estendendo gli obblighi di pubblicità e trasparenza a questi enti vi si può riuscire, nel pieno rispetto del principio di trasparenza che deve essere esteso a tutti gli enti facenti parte del sistema nazionale di istruzione. Noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo deciso di non mettere la testa sotto la sabbia; siamo qui, per conto dei cittadini, a invitare tutti i parlamentari di maggioranza e opposizione a partecipare a questa battaglia di civiltà per la qualità della formazione di migliaia di bambine e bambini e per i diritti di migliaia di lavoratori del mondo della scuola. Vogliamo valorizzare gli istituti virtuosi e obbligare quelli che non lo sono a diventarlo, nel rispetto della funzione pubblica cui assolvono, a beneficio di tutti gli studenti che non possono essere collocati in queste scuole solo perché le famiglie hanno bisogno di un tempo-scuola più adatto alle proprie esigenze, ma per assolvere al loro diritto-dovere all'istruzione riconosciuto dalla Costituzione. Annuncio pertanto il voto a favore della mozione di cui sono prima firmataria per conto del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

imprenditrice lombarda, ma soprattutto fondatrice e prima presidente per lungo tempo del Fondo ambiente italiano (FAI). Credo che il suo impegno, la sua figura e la sua determinazione nel far sì che anche nel nostro Paese, come nei Paesi anglosassoni, i privati potessero e possano farsi carico, attraverso raccolte fondi specifiche, della valorizzazione, della salvaguardia, del recupero e del restauro dei beni culturali e ambientali siano stati un successo straordinario, del quale bisogna rendergliene merito e per il quale credo il nostro Paese debba dirle grazie. Se in Italia, infatti, si è riusciti a sviluppare una maggiore sensibilità sui temi dei beni culturali e ambientali, lo si deve anche grazie al lavoro del FAI e della presidente Crespi. Penso alle giornate di primavera del FAI e ai censimenti dei luoghi del cuore, iniziative che hanno mobilitato migliaia di persone nel desiderio di conoscere meglio il nostro patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale e nel desiderio anche di poter recuperare e valorizzare alcuni beni specifici. Mi piace poter ricordare questa insigne figura

per tanti anni del «Corriere della Sera». Non è stata solo imprenditrice nell'ambito dell'editoria, ma anche, ereditando la tradizione della sua famiglia, imprenditrice nel mondo del cotone. Ha poi dedicato tempo ed energie all'agricoltura con una tenuta che ha fatto un po' scuola.

Signor Presidente, prendo la parola per esprimere, a nome dell'intero Gruppo MoVimento 5 Stelle, le nostre più sentite condoglianze alla famiglia del collaboratore ONU Mario Paciolla. trovato morto il 15 luglio scorso nel suo appartamento a San Vicente del Caguán in Colombia. Ci vorrà qualche giorno per conoscere i primi risultati dell'autopsia, ma vorrei ringraziare l'ambasciatore Gherardo Amaduzzi e il nostro ministro degli affari esteri Luigi Di Maio che si sono subito attivati per sostenere la famiglia in questo difficile momento e per far luce sulle circostanze che hanno portato alla morte di Mario. Al Ministro ho anticipato che presenterò un'interrogazione per aggiornare il Parlamento su questo caso. Del resto l'ipotesi del suicidio, avanzata in un primo momento dalla polizia colombiana, sembra sempre meno attendibile. Ci sono infatti troppe incongruenze che potrebbero far presagire un nuovo caso Regeni; in particolare un biglietto aereo, prenotato per il 20 luglio, giorno in cui il nostro cooperante sarebbe dovuto rientrare a Napoli. A diversi amici Paciolla aveva poi confidato di sentirsi in pericolo; sul corpo, inoltre, sono stati trovati dei tagli incompatibili con l'ipotesi del suicidio. Presidente, auspico inoltre che la missione ONU in Colombia presti la massima collaborazione alle autorità, fornendo tutte le informazioni in suo possesso. C'è infine un contesto politico, quello dell'accordo di pace tra FARC e Governo colombiano, che non ha portato alla stabilità auspicata. In tutta la Colombia si susseguono omicidi mirati di sindacalisti, ambientalisti e attivisti per i diritti sociali ed economici. Sono già 348 i *leader* sociali assassinati sotto il Governo Duque, 234 dei quali soltanto nel 2019: numeri altissimi su cui è calato il silenzio della comunità internazionale, particolarmente attiva invece in altri contesti. Concludo, Presidente, ricordando che il lavoro di Paciolla e di molti suoi colleghi, che in tante parti del mondo si prodigano in prima persona per la pace e la giustizia, è un valore prezioso per il nostro Paese e la sua politica estera. Purtroppo molte volte questi ragazzi rischiano la propria vita per perseguire alti ideali di giustizia. A loro va tutto il nostro riconoscimento. Presidente, ho chiesto di intervenire per portare a conoscenza dell'Assemblea quanto è accaduto in queste ore in Umbria, a Gualdo Cattaneo, che è lo specchio di quanto sta avvenendo a Taranto, in Basilicata e in Veneto e che è la diretta conseguenza delle politiche di questo Governo, che già solo annunciando la volontà di voler cancellare i decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini ha visto moltiplicare per tre gli sbarchi nel primo semestre: da 2.500 a 7.000. Succede allora che persone che arrivano in Italia

per correttezza istituzionale dalla prefettura, con decisioni che vengono prese sopra la loro testa, e che venticinque di questi clandestini siano arrivati, appunto, a Gualdo Cattaneo, provenienti dalla Tunisia. Non ci risulta che in Tunisia ci siano guerre. Sono arrivati il giovedì pomeriggio; ebbene, già il sabato pomeriggio 23 su 25 si erano dileguati indisturbati, visto che non c'era stato nessun controllo da parte dei gestori.

se un libro non l'avesse già scritto Mario Giordano che si intitola «Profugopoli». Ebbene, non è accettabile che i gestori non garantiscano una presenza fisica, continua e costante nelle strutture.

predisposto una mozione - e non semplicemente un'interrogazione per sapere che cosa non abbia funzionato - che preveda regole più stringenti e sanzioni

i propri errori, soprattutto quando, come sta avvenendo in queste ore, si mette a rischio, ancor prima della sicurezza, la salute dei cittadini italiani.

migliaia di cittadini, se non decine di migliaia (ripeto, a pochi chilometri da Roma), stanno subendo una vicenda che ha dell'incredibile: odori nauseabondi che si sentono da svariati mesi in questo territorio. Sabato scorso è stata fatta una manifestazione a San Cesareo, organizzata dal comitato «Aria pulita», cui hanno partecipato numerosi cittadini che non possono più respirare. In particolare nelle prime ore del giorno, le ultime della notte, si sentono degli odori nauseabondi dei quali non si riesce a capire la provenienza. L'ARPA Lazio sta svolgendo le sue indagini, ma purtroppo le sue centraline non sono tarate per gli odori nauseabondi, ma soltanto per l'inquinamento atmosferico. Pertanto, sono in

Sono qui perché i sindaci dei Comuni di Colonna, San Cesareo, Monte Compatri e Rocca Priora hanno scritto alle procure della Repubblica, quindi mi aspetto che le procure della Repubblica di Tivoli e di Velletri, che sono state interessate, svolgano presto il loro lavoro. Il gruppo dei Carabinieri di Frascati sta indagando tramite i carabinieri forestali ed è stato interessato anche il Nucleo operativo ecologico. Stanno controllando a tappeto tutti gli impianti. Credo che sia una situazione che colpisce la salute e che ha dell'inverosimile, quindi auspico che l'Assemblea del Senato e i Ministri interessati possano svolgere immediatamente il loro compito. Questi cittadini e i loro figli non possono più vivere in questa situazione, quindi al più presto l'autorità giudiziaria, la polizia giudiziaria e l'intervento normativo debbono porre rimedio a questa situazione di incredibile disagio.

ed erano in gravi difficoltà. In particolare, uno di essi non era più in grado di nuotare perché afflitto dai crampi nel tentativo, inutile, di contrastare la corrente. Entrambi erano in immediato pericolo di vita.

avendo la presenza di spirito di portare con sé un attrezzo galleggiante. Ha raggiunto i due ragazzi, è riuscito a farli aggrappare al galleggiante e poi, con non poca fatica, a riportarli a riva salvando loro la vita. Quel quarantenne è il senatore Marco Siclari, che ha compiuto questo atto ovviamente senza qualificarsi da senatore ma qualificando la propria carica con un atto davvero rischioso, perché due ragazzi di quattordici-quindici anni - lo dico da maestro di salvamento a nuoto al soccorritore presi dal panico, mettono davvero in pericolo la sua vita. Invece la vicenda è finita bene: si sono salvati i ragazzi e anche il senatore Siclari è potuto tornare ed ora essere con noi in Aula.